decreto ristori e le sue integrazioni con i decreti *bis*, *ter* e *quater* hanno introdotto nuove disposizioni in materia fiscale e contributiva per il sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro, oltre che ulteriori misure urgenti. L'approvazione di nuovi emendamenti da parte delle Commissioni riunite 5a e 6a ha introdotto diverse novità a sostegno delle famiglie e dei lavoratori penalizzati dall'emergenza. È giusto rimarcare che queste sono frutto di un lavoro congiunto fra maggioranza e opposizioni. Queste ultime, per alcune modifiche condivise, hanno proposto emendamenti per circa 380 milioni di euro rispetto ai 600 a disposizione del Parlamento su questo provvedimento. È la prima volta, in questa fase difficile e tormentata della vita del Paese, che maggioranza e opposizione riescono a instaurare un dialogo e un confronto produttivo, consentendo di trovare punti di condivisione e valorizzazione di alcune proposte migliorative. una cosa positiva che ci auguriamo possa ripetersi. Italia Viva-PSI ha contribuito a migliorare e arricchire con i propri emendamenti questo corposo e variegato decreto. Dopo aver proposto questa misura in vari provvedimenti, questa volta le Commissioni riunite hanno ridotto, per l'anno 2021, la spesa sostenuta per le utenze elettriche diverse dall'uso domestico nei confronti delle attività già attive dal 25 ottobre 2020 e dotate di partita IVA attiva rientranti nei codici Ateco che il provvedimento tutela, per un costo complessivo di riduzione delle bollette nei confronti dei soggetti considerati pari a 180 milioni di euro per il 2021. Molto si è detto in passato per criticare misure come il *jobs act*, che, attraverso lo sgravio contributivo, ha comunque assicurato un aumento dell'occupazione. Oggi quella stessa *ratio* sta alla base dell'approvazione dell'emendamento che, al fine di promuovere in modo specifico l'occupazione giovanile, che si riconosca uno sgravio contributivo integrale per i contratti stipulati nel 2021 ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello. Italia Viva-PSI è impegnata sui temi della parità di genere. Un nostro emendamento, approvato dalle Commissioni riunite 5a e 6a, assicura che tra i componenti dei consigli nazionali degli ordini professionali ci sia equilibrio tra i generi. A tal fine, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato. Inoltre, l'emendamento prevede che presso i consigli nazionali sia istituito un comitato a tutela delle pari opportunità. un altro emendamento si prevede l'attribuzione di un contributo in favore delle cooperative sociali con riferimento alle assunzioni di donne vittime di violenza di genere e inserite nei relativi percorsi di protezione con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Da settimane esprimiamo la nostra preoccupazione per la sorte dei pescatori italiani fermati in Libia. Con un nostro emendamento viene garantito un adeguato supporto economico in favore dei loro familiari e delle stesse aziende. A tal fine si prevede che, con un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, siano determinate le modalità per l'erogazione dei contributi. Le Commissioni riunite 5a e 6a hanno approvato un emendamento che, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, esonera gli esercizi di ristorazione e quelli dediti alla somministrazione di pasti e bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. La disposizione mira a favorire la ripresa delle attività turistiche. Vengono esonerati inoltre dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche o del relativo canone i titolari di concessioni e autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Ci siamo occupati anche di territorio. Al fine di favorire e potenziare l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte della cittadinanza dei piccoli centri urbani, un emendamento riconosce, per l'anno 2021, alle farmacie che operano nei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti un credito di imposta per un importo massimo di 3.000 euro per l'acquisto e il noleggio di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina. In modo più puntuale, poi, un emendamento è volto a favore dei lavoratori appartenenti al bacino Pip, cosiddetto Emergenza Palermo. La Regione Siciliana è autorizzata, al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro atipico, a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società per il transito del personale. Un ulteriore emendamento è volto a consentire al responsabile unico del procedimento relativo al progetto Mantova di apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, sempre nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee, al fine di consentire il completamento dei lavori e, al contempo, la valorizzazione del territorio. In tema di studio e formazione, un emendamento è volto ad ampliare, attraverso l'operatività di Studiare Sviluppo Srl e di INDIRE, l'offerta di assistenza e supporto alle amministrazioni centrali, alle Regioni e agli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza. Il secondo emendamento prevede, quindi, un contributo di tre milioni per i collegi universitari di merito. Infine, in ambito sociale, un emendamento è volto a modificare le norme attuali ed equiparare le imprese sociali alla stregua delle cooperative sociali, a loro volta considerate imprese sociali, ai fini degli obblighi della legge n. 68 del 1999. Ciò per sostenere quelle imprese che intendono promuovere l'inserimento di lavoratori in condizioni di svantaggio sociale e, nel contempo, assolvere agli obblighi previsti dalla legge n. 68 del 1999. Presidente, crediamo che il lavoro fatto per questo decreto sia complessivamente positivo. Ringrazio i presidenti D'Alfonso e Pesco, i relatori Marino e Presutto, insieme ai sottosegretari Guerra e Castaldi, per la conduzione dei lavori e l'attività di coordinamento e analisi delle diverse proposte. Mi sia, però, consentito esprimere una preoccupazione, che credo ampiamente condivisa, circa il sempre più ingessato *iter* cui siamo costretti a sottostare nell'esame dei diversi provvedimenti. Ancora una volta, signor Presidente, un provvedimento del Governo viene vagliato solo da una delle due Camere di cui si compone il Parlamento italiano. Siamo ormai ad una modifica *de facto* della Costituzione materiale del nostro Paese, con un surrettizio monocameralismo alternato. Credo che nessuna forza politica in quest'Aula possa apprezzare la stabilizzazione di una modalità operativa impropria e problematica. Faccio, quindi, appello a tutti, alla Presidenza, ai Gruppi, al Governo, perché, con responsabilità, si metta mano alle norme regolamentari e costituzionali per tornare a dare piena dignità al Parlamento, detentore del potere legislativo a norma di Costituzione, ma che, purtroppo, nella prassi è sempre più spesso relegato ad un ruolo marginale.

tanti emendamenti. Emendamenti importanti, indispensabili e di buon senso. Richieste arrivate dal pianeta Terra, da artigiani, commercianti, professionisti, partite IVA, associazioni di categoria, semplici cittadini. Scostamento di bilancio per oltre 100 miliardi di euro. Abbiamo iniziato con il decreto cura Italia e con le dichiarazioni del presidente Conte: siamo un modello. L'Europa ci segua. Meno male che l'Europa non ci ha seguito. Il decreto rilancio, sempre il presidente Conte: un testo complesso, pari a due manovre, un lavoro incredibile per orientare l'economia a una pronta ripartenza. Una ripartenza che non c'è stata. Per arrivare, poi, al decreto agosto. Intervento di portata storica e il *premier* Conte che ribadisce: non vogliamo lasciare indietro nessuno. E tanti, troppi, sono stati lasciati indietro. mesi e mesi di mancata programmazione e di mancato ascolto del territorio, siamo arrivati ad oggi, con quattro decreti ristori.

ha presentato un pacchetto di emendamenti, che avrebbero dato respiro e dignità alla categoria dei lavoratori fragili. Con un emendamento avevamo chiesto la possibilità di equiparare l'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, per le persone immunodepresse, per i malati oncologici, per chi sta

per i genitori lavoratori che hanno figli con gravi disabilità e di poterne usufruire fino al 31 dicembre. Anche questo emendamento è stato bocciato. Non ci venite a dire che è una questione trasversale, che interessa tutti i partiti, perché altrimenti le nostre proposte e i nostri emendamenti non sarebbe finiti nel cestino. Come avete trovato le risorse per i monopattini, e tanti altri soldi che avete rimesso nella legge di bilancio, come avete trovato le risorse per i banchi a rotelle, come avete pagato i 72 milioni di euro di provvigioni per l'acquisto di mascherine,

nei centri storici dei piccoli Comuni a vocazione turistica, che avete abbandonato, considerando solamente i capoluoghi di Provincia. Ne ricordo uno fra tutte, San Gimignano,

state completamente dimenticate. Vorrei soffermarmi ora sull'articolo 633 del codice penale, secondo cui «Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito,

con una norma, autorizzano chi occupa senza titolo un immobile ad autocertificare la residenza nell'immobile stesso, per ottenere così il riconoscimento del reddito d'emergenza. Ovviamente anche l'emendamento presentato dalla Lega, che metteva fino a questa vergognosa norma, è stato bocciato. Quindi il Governo e la maggioranza non solo incitano all'illegalità, ma fanno di più: dicono ai delinquenti di occupare abusivamente gli immobili, perché, se li occupano, li paghiamo. È questa l'Italia che vogliamo? Noi non la vogliamo così! Vi siete resi conto che questa norma vanifica il complesso e difficile lavoro, che svolgono le amministrazioni locali, per la lotta contro l'abusivismo?

Vorrei ricordare ai colleghi che le scuole dovevano aprire a settembre: i nostri ragazzi hanno perso mesi di scuola e l'incapacità e l'incompetenza di questo Ministro la pagheranno i nostri e i vostri figli. Concludo davvero, signor Presidente, mi scusi. Il ministro Bonafede, con l'avallo del Governo e dei partiti di maggioranza ha portato avanti un vero e proprio svuota carceri, perché saranno messi in libertà, tra arresti domiciliari e braccialetti elettronici, 5.000 detenuti, dimenticandosi ancora una volta della polizia penitenziaria, che è priva di mascherine

gentili colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, siamo qui per mettere l'ultima parola alla conversione del decreto-legge n. 137 del 2020. In realtà, siamo qui a convertire quattro decreti-legge, i nn. 137, 149, 154 e 157. Il fatto stesso che siamo qui a convertire quattro decreti in un decreto solo credo sia sufficiente a fornirci una fotografia della complessità

le conseguenze dell'epidemia Covid lasciano alla nostra comunità civile. Questi quattro decreti-legge contengono proroghe di versamenti, rinvio di scadenze fiscali, esenzione da versamenti, indennità, contributi a fondo perduto, fondi di sostegno per i settori in particolari situazioni di drammaticità a causa dell'emergenza, crediti di imposta, prolungamenti di cassa integrazione, bonus per settori particolari, finanziamenti a cittadini e imprese per il rilancio dell'economia, sostegno alle Regioni e ai Comuni, bonus, congedi parentali, redditi di emergenza, sostegni particolari al settore agricolo, al terzo settore (lo sport, lo spettacolo, la cultura) e un po' a tutti i settori colpiti dalla situazione che stiamo vivendo. vivendo. Come già è stato detto da molti dei colleghi che mi hanno preceduto, sono tanti gli interventi messi in campo, perché si è cercato di affrontare tutti i risvolti della situazione di emergenza nella quale ci troviamo a navigare.

che, dei 600 milioni messi a disposizione per le misure di integrazione da parte del Parlamento, ben 380 siano stati destinati a provvedimenti segnalati

consapevolezza della necessità di un Paese più semplice. Leggendo moltissimi degli emendamenti presentati, alcuni dei quali poi sono stati anche approvati, ci siamo resi conto di quanto ci sia da lavorare per semplificare la vita dei cittadini e delle imprese, che nella quotidianità si trovano ad affrontare mille complessità. dovremo tornare e che dovremo lavorare tutti insieme, perché questa è una sfida fondamentale per guardare con maggiore serenità al futuro. La seconda grande consapevolezza è che, passata questa emergenza (che speriamo finisca presto), dovremo tutti insieme lavorare per una visione più strategica e progettuale per il futuro del Paese. Quanto successo ci consegna sicuramente la necessità di affrontare e di risolvere le questioni quotidiane, ma ci consegna soprattutto la consapevolezza che dobbiamo disegnare, da adesso in poi, un Paese futuro che tragga dalle vicende che abbiamo vissuto le indicazioni per modellarsi in modo nuovo. Credo che questo sia un dato assolutamente fondamentale per i passaggi ulteriori che andremo a fare, a partire dal cosiddetto decreto ristori cinque, che già si palesa all'orizzonte. La terza consapevolezza è che tutti insieme dobbiamo lavorare alla ricostruzione di un nuovo modello di coesione sociale. di coesione sociale. Il fatto di dover ragionare su come andare incontro a coloro che non sono inquadrabili nelle figure ordinarie di lavoro e di impresa

in qualche modo evidenziavano settori di elusione, di evasione o comunque di marginalità economica che richiedono di essere ripensate.

Dicevo prima della consapevolezza che le vicende che abbiamo vissuto ci consegnano. Credo che, nel momento in cui guardiamo al decreto-legge ristori 5

E dovremmo avere chiaro che, a partire dalle misure prossime che dovremo affrontare, i tasselli che caleremo sul campo dovranno andare nella direzione di quell'idea di Italia e di comunità civile che abbiamo in mente. Siamo chiamati a risolvere le emergenze e a fare misure di programmazione per il bilancio del 2021, ma siamo chiamati soprattutto a immaginare l'Italia che vorremmo consegnare ai nostri figli. Gli investimenti fatti durante quest'anno e che ci apprestiamo a fare per gli anni a venire sono sicuramente necessari e importanti, ma sono in qualche misura a debito, e li consegneremo come tali ai nostri figli. Pertanto, dobbiamo fare in modo che questo debito, questo investimento che faremo sia assolutamente in linea con quelli che pensiamo siano le aspettative e le attese dei nostri figli. Concludo con una citazione che in tanti momenti mi è venuta in mente,

sapere che con le nostre scelte camminiamo sui sogni dei nostri figli e dei cittadini che guardano a noi. Se sapremo fare questo e sapremo calarlo nella modalità concreta in cui quotidianamente ci muoveremo in quest'Aula sui prossimi provvedimenti, credo faremo qualcosa di buono per questa nostra nostra Patria, che molto si aspetta dalle scelte che noi dovremo fare.

questa non è collaborazione. State distruggendo il Paese e ne siete responsabili voi.

il decreto ristori si aggiunge alla lista dei provvedimenti messi in campo dal Governo per far fronte alla situazione emergenziale dovuta al Covid-19. La pandemia è entrata nel nostro quotidiano con una violenza inaudita, stravolgendo le nostre abitudini e soprattutto le nostre certezze. Il 2020 è stato un anno che ci ha fatto scoprire fragili, fisicamente e psicologicamente, rendendo necessari plurimi interventi in diversi ambiti: sanità, scuola, famiglia e organizzazione del lavoro a distanza nei settori economici e commerciali. La prima ondata Covid è stata affrontata con una serie di decreti i quali, seppur con qualche difficoltà organizzativa dovuta all'inaspettato carico di lavoro, hanno cercato di arginare al meglio le più disparate problematiche. al decreto rilancio, al decreto agosto - o rilancio-*bis* - e a tutti gli aiuti economici che con essi sono stati disciplinati per un totale di 100 miliardi di euro che sono stati stanziati per aiutare il nostro Paese. Tutti noi abbiamo sperato che i tempi difficili non si ripresentassero più nel corso dei mesi, cercando di riconquistare piccoli spazi e di ricominciare con le piccole azioni quotidiane, quelle azioni di cui spesso ci siamo lamentati, definendole banali *routine*, ma di cui abbiamo imparato ad apprezzare l'essenzialità. La calma è stata solo apparente e la seconda ondata che ci ha colpiti ha reso necessari nuovi provvedimenti. Il Governo ha pertanto varato, ad ottobre, il decreto ristori che ha previsto il riutilizzo dei fondi non impiegati con i precedenti provvedimenti. Questa non è una mancanza del Governo, un errore, ma è la naturale conseguenza della necessità - unica a causa della pandemia - di attivare con la massima celerità gli strumenti in grado di aggiungere il maggior numero di imprese e cittadini nel minor tempo possibile. E così è stato. D'altro canto, talvolta, l'ottimo è nemico del bene e allungare i tempi per scrivere un decreto perfetto avrebbe reso gli strumenti stessi poco efficaci. Pareto insegna, a questo punto. Così succede anche per lo stesso decreto ristori di ottobre che, se da un lato ha avuto la possibilità di raggiungere subito le imprese di 73 categorie di codice Ateco e di pagare entro i primi giorni di dicembre già 2,4 miliardi di euro, dall'altro era insufficiente nella sua portata risolutiva. Ecco che quindi è nato il ristori-*bis,* che ha ampliato a 130 le categorie di imprese beneficiarie degli indennizzi, ha definito proroghe di termini per gli acconti fiscali, sospensione del versamento dei contributi previdenziali, cancellazione della rata IMU di dicembre e ancora congedo straordinario per i genitori dovuto alle chiusure delle scuole secondarie di primo grado, *bonus baby sitting*, fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore e potenziamento del trasporto pubblico locale. Poi nello scenario hanno fatto ingresso altri due provvedimenti: il ristori-*ter*, che ha previsto 2 miliardi a favore dell'estensione dei contributi a fondo perduto per le Regioni passate in zona arancione o rossa, ma anche ulteriori 400 milioni a beneficio dei Comuni per l'emergenza alimentare, e il ristori-*quater*, che ha aggiunto 9 miliardi per coprire una vasta serie di proroghe fiscali (versamento Irpef, Ires, IVA, contributi, rate della rottamazione-*ter*) che serviranno a dare maggiore solidità alle nostre imprese e partita IVA, e indennità per le Forze dell'ordine e i Vigili del fuoco. Numerosi sono stati gli emendamenti approvati nel corso dell'*iter* parlamentare, tra i tanti ne cito due fortemente voluti dal MoVimento 5 Stelle. Il primo, a mia prima firma e condiviso con le altre forze di maggioranza, riguarda l'esonero dal pagamento TOSAP/COSAP per il primo trimestre 2021

dovute al rispetto di tutte le norme anti-Covid, tra cui il distanziamento dei tavoli e la conseguente necessità di acquisire ulteriori spazi per i tavoli all'esterno, l'eliminazione di questo ulteriore costo concede respiro alle attività economiche in difficoltà.

Detto emendamento permetterà un maggiore utilizzo di questo strumento, utilissimo nell'attuale fase per la ripartenza e la nascita di nuove imprese. Complessivamente il pacchetto dei quattro decreti ristori conta su una dote superiore ai 19 miliardi di euro per potenziare ed estendere la rete di protezione intorno al nostro tessuto economico-produttivo. Nella notte tra venerdì e sabato nelle Commissioni riunite bilancio e finanze abbiamo approvato una settantina circa di emendamenti che valgono poco più di 600 milioni di euro, che hanno contribuito a interessare ulteriori settori del nostro Paese, ma abbiamo chiuso - e questo non va dimenticato e va detto agli italiani - perché la maggioranza ha concesso alla minoranza il 60 per cento circa di tale importo, in quanto l'atteggiamento ostruzionistico di parte delle opposizioni era tale da far rischiare di non chiudere il provvedimento. Avrei potuto dire che abbiamo chiuso perché, nonostante il confronto serrato fra maggioranza e opposizione, alla fine ha prevalso il buonsenso. Ma la realtà è che le opposizioni - o parte di esse - hanno deciso di fare ostruzionismo parlamentare in un momento in cui si dovrebbe invece viaggiare tutti uniti a supporto dell'Italia, così come ha richiesto anche il Presidente della Repubblica. Queste cose, signor Presidente, vanno dette al Paese e a chi ci ascolta e dobbiamo soprattutto ricordarle noi, perché la dialettica parlamentare è una cosa, fare ostruzionismo in una situazione pandemica è altra cosa, perché non si deve giocare con la vita degli italiani. A tale proposito, faccio una digressione e ricordo a chi mi ha preceduto che si è vantato di aver presentato 1.500 emendamenti, che è esattamente questo il problema, se dobbiamo pensare all'Italia. sempre a chi ci ha preceduto che le misure per gli agenti di commercio sono all'interno dell'articolato del ristori-*quater*, per cui parlarne come una cosa che non è passata non ha senso. Ciò detto, signor Presidente, la situazione emergenziale dovuta al Covid-19 è unica della storia della nostra Repubblica; non si è mai verificata una situazione così complessa e, a causa della sua natura mutevole giorno dopo giorno, può essere approcciata non con gli schemi classici, ma con provvedimenti che vanno tarati di volta in volta. Siamo consapevoli che quello che abbiamo fatto fino ad ora non è sufficiente: sono ancora tanti gli ambiti di cui il Governo e noi come forze di maggioranza dobbiamo occuparci. Ma di una cosa siamo certi: nessuno di noi si è tirato indietro; abbiamo sempre lavorato; questo Parlamento non si è mai fermato e tantomeno le Commissioni, anche in mezzo alle tante difficoltà organizzative che ci accompagnano. Mi auguro solo che, così come abbiamo cercato di coinvolgere tutti, perché i provvedimenti riguardanti il Covid-19 non possono e non devono avere colore, le opposizioni - o meglio, parte di esse - decidano per i futuri provvedimenti di collaborare davvero per il bene del Paese con i fatti e non solo con le parole.

sono due i sentimenti che provo di più: rabbia e impotenza. Provo rabbia per come state gestendo la crisi economica del nostro Paese in modo approssimativo, con una comunicazione incomprensibile e senza visione strategica; rabbia nel leggere i quattro decreti oggi in discussione, ironicamente chiamati ristori. Provo poi impotenza davanti a provvedimenti lontani dal mondo lavorativo, dal mondo delle partite IVA e degli imprenditori, dal mondo reale. Dopo averci snobbati per mesi, ora vi riempite la bocca di parole quali collaborazione solo perché siete con l'acqua alla gola e, con la vostra incompetenza, state trascinando nel baratro l'Italia intera. In questi mesi ci siamo battuti per tutte le categorie che hanno subito dei danni, per vederle risarcite e sostenute. Che senso ha poter restare aperti, ma non poter lavorare perché il mio committente è chiuso? La logica doveva essere quella dell'intera filiera ma, siccome la proposta arrivava da noi, siete rimasti sordi continuando con il caos dei codici Ateco. Vi state comportando come nemici degli italiani. Voglio invece ringraziare gli imprenditori che hanno anticipato addirittura di tasca loro la cassa integrazione: loro sì che hanno a cuore il bene dei lavoratori e vi danno lezioni di civiltà ogni giorno. Siamo stanchi dei vostri trattamenti differenziati tra dipendenti garantiti e imprenditori e professionisti, solo tartassati. Chi lavora nel pubblico, compresi noi, è stipendiato da coloro che pagano le tasse, fanno girare questo Paese, rischiando personalmente e dando lavoro ad altri, e voi li avete lasciati soli soli e senza tutele. Siamo stanchi di un Governo nemico di chi fa veramente girare l'economia nel nostro Paese. Senza imprese non c'è lavoro. Fate così fatica a capirlo? Smettetela di trattare le partite IVA come evasori, delinquenti, cittadini di serie B, da ostacolare in ogni modo. Vogliamo che i giovani possano scegliere liberamente se intraprendere, oppure lavorare da dipendenti e possano farlo con gli stessi diritti, gli stessi doveri e le stesse condizioni, anzi, addirittura con maggiore sostegno se, grazie alla loro iniziativa imprenditoriale, daranno lavoro anche ad altri. Molti di voi però non hanno nemmeno idea di che cosa io stia dicendo. Avete autorità senza autorevolezza. Non siete credibili. State ignorando quel mondo di persone che si alzano ogni mattina all'alba. Non sapete che cosa vuol dire fare dei sacrifici e far quadrare i conti a fine mese, come un buon padre di famiglia.

Parlate invece di come sanare le mostruose inefficienze e ridurre le voragini di sprechi. *(Applausi).* State raccontando agli italiani che arriveranno fiumi di denaro, ma perché non dite che sono delle ricevute di pegno che le generazioni future dovranno restituire a una Europa che ci imporrà un altro avvocato del popolo? Avete fatto scempio del Parlamento, costituito ridicole *task force* con centinaia di persone pagate con denaro pubblico, generando solo una confusione indecorosa. Lo scostamento complessivo di 108 miliardi è stato buttato in mance e *bonus* di ogni tipo, dai monopattini alle biciclette, dalle vacanze alle lotterie.

Non so quanto tutto ciò sia incompetenza e quanto volontà di distruggere in modo scientifico il nostro Paese. Stiamo andando verso la più grande crisi economica e sociale dopo la Seconda guerra mondiale, con il peggior Governo che ci potesse capitare. State minando le radici e le tradizioni del popolo italiano. Ogni santo giorno puntate ad aumentare la paura degli italiani tramite un'informazione scandalosa. Dopo quasi un anno mancano ancora un piano pandemico e dei protocolli chiari per le cure a domicilio. Dopo aver abolito la messa di Pasqua e ora la millenaria tradizione della messa di mezzanotte, schierate 70.000 uomini armati per controllare passeggiate e spostamenti. Immaginate se lo avesse fatto il pericoloso sovranista Salvini? Vi sentite legittimati a decidere chi gli Italiani devono vedere all'interno della propria sfera familiare e intima. Vergognatevi! Gli italiani hanno già visto chi siete. Non potete più nascondervi. Il re è già nudo e la libertà di decidere da chi essere governati è ancora valida. Preparatevi.

Signor Presidente, ci troviamo nel mezzo della seconda ondata di questa grave pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero. Stando alle dichiarazioni dei virologi e dei medici che sono in prima linea, a cui va sempre rinnovato il nostro ringraziamento, anche a nome di tutti gli italiani, per il commovente impegno che hanno profuso e che stanno continuando a profondere per cercare di salvare quante più vite umane possibili, si prospetta una terza ondata per l'inizio del nuovo anno, a meno che non arrivi quanto prima il tanto atteso via libera dell'EMA per la somministrazione dei vaccini che hanno già superato positivamente la sperimentazione.

IVA, albergatori, lavoratori stagionali e potrei continuare a lungo: ognuna di queste categorie ha subito perdite importanti, che per alcune di loro hanno già significato la morte economica. Ebbene, in una situazione di tal genere un Governo responsabile avrebbe messo in campo azioni strutturali tese - da una parte - a consentire a tutte queste attività una sopravvivenza economica e - dall'altra - a mettere in campo azioni di garanzia per le famiglie. Fratelli d'Italia sin da subito si è resa disponibile, con spirito collaborativo e nell'interesse esclusivo di tutti gli italiani, ad avanzare proposte in tal senso, contemperando la giusta tutela della salute pubblica con l'innegabile tutela dell'economia e della produttività. Purtroppo però il Governo si è dimostrato, almeno sino a questo momento, sordo a qualsiasi nostra proposta. Ciò è dimostrato dal fatto che il decreto-legge in discussione è stato immediatamente sconfessato dallo stesso Governo, che è dovuto ricorrere ai ripari con i decreti-legge ristori-*bis, ter* e *quater,* gettando l'intero Paese in un grado di insofferenza e di incertezza. tale provvedimento si è dimostrato di corto respiro e alla lunga ha scontentato un po' tutte le categorie, per l'irrisorietà dei ristori riconosciuti a fronte delle perdite subite. Infatti, pensare di dover ristorare solo le attività costrette alla chiusura, dimenticandosi completamente di quelle facenti parte del loro indotto che, seppur non chiuse per decreto, hanno subito nei fatti la medesima sorte, è stata una scelta sbagliata. Penso - ad esempio - alle aziende del settore delle mense scolastiche, che sono state escluse dal provvedimento, nonostante alcune Regioni in zona rossa hanno chiuso le scuole e, di conseguenza, le mense scolastiche. a quelle attività di servizi correlati ai poli museali che, in ragione delle chiusure imposte a quest'ultimi, hanno di fatto sospeso tutte le loro attività; o alle imprese all'ingrosso nel settore della ristorazione che, a causa della chiusura dei ristoranti, delle pizzerie e dei bar, hanno compresso il loro fatturato e sono stati lasciati fuori. Per questo Fratelli d'Italia aveva avanzato proposte di buonsenso, come il ristoro di tutte le attività che hanno avuto una contrazione del fatturato superiore al 33 rispetto all'anno precedente, oppure l'applicazione di un regime IVA e fiscale agevolato fino al 2022 per le aziende che garantiscono la continuità societaria, continuando con il riconoscimento di un sistema unico di ammortizzatori sociali, perché tutti i lavoratori sono uguali e non devono esserci discriminazioni fra autonomi e dipendenti. dipendenti. Nessuna di queste proposte è stata recepita dal Governo che, anzi, ha continuato a mettere in campo azioni che, piuttosto che essere risolutive e strutturali, tendono a spostare il problema in avanti. Ribadiamo il

L'inevitabile conseguenza sarà che, entro alla fine di quest'anno, sono a rischio di chiusura 350.000 piccole attività, che lasceranno senza lavoro un milione di addetti. Dall'inizio della crisi pandemica le risorse che sono state stanziate direttamente a sostegno delle imprese italiane ammontano a circa 35 miliardi di euro.

la situazione economica in questo periodo natalizio è poi destinata a peggiorare ulteriormente. Ci saremmo aspettati più coraggio, quel coraggio che avrebbe dato un po' di fiducia in più a tutti gli italiani, che oggi si sentono sopraffare da un senso di insicurezza e sfiducia per il futuro. Sarebbe auspicabile, infatti, un sostegno maggiore per quelle imprese che continueranno a restare aperte, con un netto cambio di passando dalla logica dei ristori a quella dei rimborsi, indennizzando fino al 70 per cento i mancati incassi e, in secondo luogo, abbattendo i costi fissi, così come ha stabilito la Commissione europea. Voglio comunque sottolineare che, nel corso dell'esame di questo provvedimento, per la prima volta sono stati accolti alcuni emendamenti presentati dal centrodestra. Ciò dimostra che le nostre proposte sono aderenti alla realtà. Mi auguro che questo percorso continui nell'esclusivo interesse degli italiani.

il blocco delle attività sociali ed economiche anche attraverso quello che è stato nel primo periodo un *lockdown* generale; poi, nella seconda ondata, da settembre in poi, anche attraverso l'aiuto, il sostegno e la condivisione con le Regioni, vi è stato un *lockdown* più selettivo. È chiaro che una scelta di questo genere è penalizzante per l'economia del Paese. Ma, se serve per tutelare quello che è un bene primario e costituzionalmente garantito, come la salute, allora va bene. Ma deve essere chiaro che, per attuare una strategia di questo genere, serve una premessa necessaria, e cioè che lo Stato garantisca e indennizzi tutte quelle categorie alle quali ha imposto la chiusura forzata; una chiusura che ha di fatto generato delle perdite di bilancio e una situazione drammatica che l'economia e le aziende coinvolte si trovano addosso in questo momento. Farsene carico vuol dire anche avere la capacità da parte del Governo di intervenire tempestivamente, o meglio, anche di intervenire in anticipo rispetto alla situazione; in anticipo proprio per aiutare a sostenere le imprese, i liberi professionisti, gli artigiani e le famiglie e in modo tale - come dicevamo - da garantire quelle che sono le perdite. È questa la *ratio* oggi del cosiddetto decreto ristori, cioè la possibilità di garantire immediatamente delle misure urgenti. Sono quattro i decreti-legge ristori che sono stati emanati, ma nessuno di questi oggi

che oggi ha il Governo nell'avere una visione di lunga gittata rispetto al problema dell'economia, e continua a varare soltanto dei provvedimenti tampone. Se aggiungiamo poi che in questi provvedimenti ci sono anche delle lungaggini burocratiche, allora sicuramente il danno è fatto. Ecco perché le associazioni di categoria, le associazioni dei professionisti, le partite IVA, i commercianti e i liberi professionisti criticano il Governo, che è stato rapido nel chiudere le attività economiche, dalla sera alla mattina, ma che in questo momento non è capace di trovare delle soluzioni di ristoro e di indennizzo in maniera così veloce per quelle stesse attività che oggi stanno subendo perdite economiche. Non parliamo poi della questione che si è aperta con i decreti ristori sui codici Ateco, che hanno discriminato ancora di più le attività. Non vorrei aprire un capitolo, in

dalla parte del Paese. Fin dall'inizio di questa drammatica pandemia, la nostra scelta è stata unica: l'interesse del Paese. Per questo abbiamo sostenuto anche la settimana scorsa il voto sullo scostamento di bilancio di altri 8 miliardi e lo abbiamo votato per responsabilità nei confronti del Paese.

richiede una verifica di Governo. I problemi sono più che altro dall'altra parte. Ma noi continueremo con un atteggiamento di responsabilità, perché abbiamo interesse che il Paese torni torni a navigare in acque più sicure e, soprattutto, a guardare con fiducia al futuro. Non ci interessano e non siamo interessati, pertanto, alle tattiche parlamentari, come saggiamente il presidente Berlusconi ieri ci ha ricordato sulle pagine del «Corriere della sera». *(Applausi)*. Noi abbiamo una visione del Paese; l'abbiamo per il futuro e, quindi, a noi le tecniche e le tattiche parlamentari non ci interessano. Noi siamo sempre per lo sviluppo e la tutela delle categorie oggi meno garantite e, cioè, quelle del lavoro autonomo, dei professionisti, del commercio, dell'artigianato e della piccola impresa. Non siamo soddisfatti del lavoro del Governo, ma continueremo a portare le nostre proposte. Lo continueremo a fare - lo stiamo facendo già nell'altro ramo del Parlamento, alla Camera - con le nostre proposte alla legge di bilancio: lavoro e giovani sono le priorità da aiutare con degli sgravi fiscali. Il semestre bianco fiscale serve per dare ossigeno alle imprese. Bisogna cercare tutte le soluzioni che garantiscono la ripresa del Paese. Per ottenere questo bisogna cambiare assolutamente rotta: basta assistenzialismo. Oggi bisogna puntare esclusivamente sugli investimenti. Noi abbiamo le proposte concrete. Se ci cercate, sapete dove trovarci perché noi, di sicuro, saremo sempre schierati dalla parte del Paese.

senatori, quando - nei mesi estivi - si discuteva del possibile secondo frangente, la comunità scientifica era divisa e questo ha sicuramente creato confusione. Ora, la seconda ondata c'è stata, nonostante la beata ingenuità di alcuni sommi professori che ci hanno raccontato, a rullo di tamburi, che il virus sarebbe sfumato con i primi tramonti estivi. E così, in un Paese come l'Italia, che vive soprattutto di servizi, di scambi, di contatti e di piccole imprese, i nostri Ministri partorivano machiavelliche strategie a due o quattro ruote e, anziché organizzare un efficace servizio territoriale e coinvolgere le Regioni in un intervento mirato, hanno pensato di alleggerire le tensioni trattando argomenti ben distanti dal tema Covid. Dispensavano buoni vacanze e intanto il picco di agosto gridava vendetta. A novembre, in ricaduta pandemica, si è capito che la mutazione di questo virus ha una caratteristica molto antipatica: non ha una mortalità elevatissima, ma non ha mezze misure, e pertanto, se non gli piaci, ti spedisce direttamente in terapia intensiva, e le terapie intensive - si sa - sono ancora oggi un lusso che appartiene a quelle poche Regioni che durante l'estate, anziché pensare se essere uomo o donna, hanno potenziato gli ospedali.

e con il Covid, al Nord siamo anche finiti di nuovo sott'acqua: l'ennesima mazzata per gli imprenditori. Cito tutti coloro che non sono capaci di imparare e si sono messi a insegnare, e ogni consiglio esperito sui territori ed espresso a gran voce dai governatori è stato scartato come come un vuoto a perdere. Con l'ordine del giorno che avevo proposto si chiedeva di istituire una zona logistica semplificata sulla fascia confinaria del Friuli-Venezia Giulia. Sapete, durante la chiusura dei confini con Austria e Slovenia, gli incassi in IVA e accise sono più che raddoppiati: numeri, signori, sono numeri; IVA e accise sono numeri per lo Stato, e non del solo Friuli-Venezia Giulia e del presidente Fedriga.

per le aree portuali, benefici fiscali per le aziende locali, ma soprattutto essere uno strumento attrattivo per i nuovi investitori, anche stranieri. A questo punto, è evidente che non solo la sanità non rientra nei vostri potenziali, ma neanche i "conticini". Essere sani, signori, è una fatica fisica e mentale, ed essere sani e anche imprenditori, in questo momento, è una *via crucis.* Il pessimismo verso il futuro innesca fobie, panico collettivo, disubbidienza e perdita di controllo sulle masse. È per questo che la gente è scesa in piazza per protestare, da Nord a Sud; sono scesi tutti: da destra ai sindacati alla sinistra più rossa, e questo dovrebbe farvi riflettere.

Siete degli incantatori di serpenti! Ma gli italiani, signori, non sono serpenti. No, signori, il flauto magico non può essere il solo strumento che avete a disposizione per dare vero ristoro a un Paese millenario e orgoglioso come l'Italia. Che Dio ci protegga, perché voi non l'avete fatto e non lo state facendo.

completare l'*iter* di esame di questi quattro decreti in uno non è stato semplice, ma questo Parlamento ha utilizzato anche quest'occasione per inserire delle norme che potessero far progredire il nostro Paese nella strada verso la modernizzazione. In questa strada un faro deve essere la ricerca scientifica che, nella tragedia che stiamo vivendo, ha rappresentato per noi la luce in fondo al *tunnel*.

per permettere ai dottorandi dell'ultimo anno di completare gli esperimenti necessari per chiudere i propri lavori di tesi. Il nostro prossimo obiettivo deve però delle borse di dottorato al minimo contributivo INPS, perché oggi i dottorandi italiani lavorano per trentasei mesi, ma ottengono soltanto trentatré mesi di contributi previdenziali. Per adeguare le borse al minimale contributivo è necessario incrementare ogni borsa di 540 euro all'anno. Pertanto, servono 16 milioni di euro per coprire i 27.000 dottorandi in corso. Questo adeguamento a fini contributivi non colmerebbe certamente il *gap* che oggi esiste tra la retribuzione dei dottorandi italiani e quella degli altri Paesi, ma sarebbe un importante passo verso il riconoscimento del valore delle dottorande e dei dottorandi italiani, che contribuiscono a far funzionare il sistema delle università e dei centri di ricerca italiani. Il secondo emendamento approvato, a mia prima firma, istituisce un fondo di 5 milioni di euro dedicato alla diagnostica molecolare per l'utilizzo di test di profilazione genomica attraverso *next generation sequencing*. La profilazione genica rappresenta una delle più importanti innovazioni per personalizzare le terapie per i pazienti oncologici, perché permette di analizzare molteplici biomarcatori su piccoli campioni e individuare alterazioni genetiche che, se presenti, rappresentano dei bersagli

invece, grazie a questo fondo dedicato, garantiamo equità di accesso per i pazienti oncologici su tutto il territorio nazionale. Questa emergenza ci ha mostrato quanto sia importante tutelare i pazienti fragili. L'aumentata mortalità per patologie oncologiche dovute a ritardi di diagnosi o mancati controlli, l'assenza di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali uniformi, la carenza di strumenti di telemedicina e la non accessibilità ai farmaci innovativi ci spingono a procedere con urgenza al necessario ammodernamento strutturale e di processo del Servizio sanitario nazionale, promuovendo le reti oncologiche regionali con un coordinamento nazionale e l'assistenza oncologica domiciliare territoriale, nonché rinnovando e modernizzando la dotazione strumentale tecnologica per la diagnostica tumorale. Ed è proprio in questa direzione che il provvedimento oggi in esame segna un traguardo importante.

di chiedere la solita ipocrita collaborazione, se poi mostra questo atteggiamento di arroganza e, soprattutto, di inefficienza. Tante, troppe, categorie e professioni - su tutti, i lavoratori fragili e il mondo delle disabilità sono state né tutelate né ristorate e nemmeno rincuorate. Briciole o poco più per realtà artigianali e agricole, per i bar, per i ristoranti, per i benzinai, per gli ambulanti, per il mondo della moda, per le piccole e medie imprese nate proprio durante il periodo del Covid-19; per le spa, per le terme, per le palestre e per chi ha speso, come loro, soldi per mettersi in regola, ma cui poi avete cambiato, voi stessi, le stesse regole. Ancora, penso alle imprese turistiche e alberghiere,

pur non avendo mai pagato la tassa di soggiorno, per due milioni di euro, dal 2014

al rispetto delle regole, non si è nemmeno interessato a scongiurare un'iscrizione alla Crif per chi non può pagare un debito: Mentre si chiudono locali di scommesse sportive e si lasciano aperte quelli per l'estrazione del Lotto in presenza, avete trovato pure il tempo di inventare la lotteria degli scontrini. L'intento per lo Stato è di incassare, ma anche di incassare, ma anche di far arrabbiare i commercianti che, nei tre quarti dei casi, devono adeguarsi con 150 o 600 euro, ovviamente senza ristoro. Per Per la CGIA di Mestre, la riffa di Stato regalerà soldi ai ricchi, perché sono loro ad avere maggior capacità di spesa, come ha già dimostrato qualche senatrice del MoVimento 5 Stelle. Io, poi, mi chiedo sempre se sia difficile far scaricare tutti gli scontrini, dando maggior valore ai prodotti italiani, tra le altre cose. Avete litigato e vi siete rinfacciati anche le briciole. Come per l'emendamento che proponeva di prorogare il versamento delle accise dei tabaccai da gennaio-febbraio 2021 a entro luglio 2021, con debenza degli interessi, lo avete bocciato perché a firma Lega, ma trasformato in ordine del giorno quello a firma del Partito Per bramosie e personalismi, questa suddetta briciola - per voi motivo solo di vanto - per i tabaccai, che sono circa 50.000, con 120.000 addetti, era ristoro vero. Nel decreto, la manina ha scelto poi, a rappresentare i vari emendamenti al ristoro per i pescatori, il testo 2 di un subemendamento del senatore Faraone, con il quale si ristorano sia le famiglie sia le imprese. E lo volete fare con 500 milioni? La Lega aveva avanzato un ristoro di 4,8 milioni, spalmato in tre anni,

in Libia! Perché non si imbarca ora? Perché non porta con sé anche il ministro Bonafede, che è di Mazara del Vallo? *(Applausi)*. Piuttosto, vediamo se l'articolo 7 del *memorandum* Italia-Libia possa essere applicato. Signori senatori, se Erdogan, in cinque giorni, ottiene la liberazione di sette suoi cittadini e Putin, in poche ore, di due cittadini russi, non credete che il Ministro degli esteri debba dare spiegazioni e, magari, le dimissioni? Abbiamo un Governo fifone, senza la capacità di compiere scelte e formulare strategie, come quando ha votato con fermezza la scelta di far entrare nei Tribunali chi, come il ministro Salvini, a testa alta, difeso con onore e fermezza gli uomini e le donne, che orgogliosamente ha rappresentato. Avete bocciato anche un emendamento di ristoro alle professioni sanitarie, perché ovviamente nemmeno questo fa parte del vostro programma. Concludo dicendo della maggioranza che state aprendo il salvadanaio dei nostri figli e state gestendo i soldi in maniera confusa, inopportuna e condizionata. Cercate di avere rispetto, orgoglio e capacità, per il bene degli italiani, ma abbiate soprattutto l'umiltà di capire che non siete all'altezza dell'incarico. Dovreste alzarvi dalle poltrone!

i temi più vari. È al nostro esame un provvedimento veramente molto complesso e complicato, perché raccoglie una serie di provvedimenti d'urgenza, con l'obiettivo di andare a ristorare tanti e tanti settori, che sono stati colpiti da questa necessità e da questo bisogno a causa della pandemia, che ci costringe ad impedire molte attività economiche, in una variazione continua delle delle aree chiuse. Una delle difficoltà maggiori delle scelte che innanzitutto il Governo - poi parlerò del Parlamento - ha dovuto portare avanti è proprio quella di non emanare dei provvedimenti che, banalmente, andassero ad interessare tutti. Ascolto sempre con attenzione i colleghi, ma

in un momento di crisi come questo. Allora, andare ad individuare puntualmente, con le dovute misure e con le variazioni legate alla chiusura e all'apertura delle diverse aree, chi ristorare e come è un tema maledettamente complesso. Su questo esercizio si sono

di coprire tutte queste persone, tutti questi lavoratori. Non dobbiamo pensare tanto e solo agli artisti e men che meno agli artisti famosi, che certamente non sono il problema; il problema sono quelle migliaia di tecnici e di operatori che lavorano, ad esempio, nel campo della grafica o della promozione. Mi riferisco cioè all'ecosistema dei lavori della cultura, che è un ecosistema complesso, articolato, variegato e che contiene in sé un elemento di disordine non riordinabile. E tuttavia a tutte queste persone, a tutte queste donne e a tutti questi uomini per la prima volta è stato riconosciuto appieno il loro essere lavoratori e non persone che si divertono a fare qualche cosa nella vita. Si è cercato e si è riuscito non

Su tutto ciò si è intervenuto e noi oggi lo dobbiamo riconoscere, così come sono stati potenziati dei fondi che sono nella disposizione del Ministero e che stanno andando puntualmente a coprire questo e quel settore che veniva escluso. Siamo soddisfatti? Ho sentito esattamente nei discorsi precedenti. È chiaro che non siamo soddisfatti. Anzitutto la soddisfazione è un sentimento che non ha niente a che vedere con la situazione in cui siamo, perché questa non è una situazione in cui si può essere soddisfatti.

dei lavoratori del settore. Però non possiamo non riconoscere che, rispetto al punto in cui eravamo, alle normative vigenti e alla fatica anche economica, ma non solo economica, c'è una sensibilità e un'attenzione da parte di questo Governo

venire. Penso agli amici che lavorano nel campo dello spettacolo viaggiante, che sono tra le categorie più in difficoltà e per i quali abbiamo previsto degli interventi economici, ma che hanno bisogno di molto altro, perché sono in una situazione particolarissima; si tratta infatti di persone che vivono vivono lungo le strade del loro mestiere e che hanno i bambini e le bambine che vanno a scuola in posti diversi. Penso inoltre agli ambulanti e a chi lavora nelle fiere. Insomma, ci sono tante persone preoccupate e in difficoltà; a tutte queste persone noi dobbiamo scegliere che messaggio dare e lo dobbiamo scegliere in maniera corale. Dobbiamo dire loro che il Parlamento italiano sta lavorando insieme; infatti molte delle misure che avevo proposto sono state approvate attraverso emendamenti a prima firma di colleghi dell'opposizione.

o vogliamo ogni volta spaventarli, allarmarli e dire che qui nessuno si sta occupando di loro? Io credo che questa seconda scelta non faccia il bene né della maggioranza, né dell'opposizione, ma faccia danno alla politica

Abbiamo approvato la riduzione del numero dei parlamentari, ma se le cose dovessero continuare così, probabilmente avremmo potuto anche esagerare:

di affidarsi a una politica seria, a una politica dibattuta anche duramente. Stiamo parlando di un decreto-legge ristori che dovrebbe fare gli interessi della comunità imprenditoriale e delle famiglie. Ho sentito i relatori che con grande buona fede si sono espressi in quest'Aula, ma comprendo la loro difficoltà. Ringrazio il Sottosegretario, che è qui presente in pianta stabile, ma il Governo è totalmente assente. C'è un rapporto di supponenza nei confronti del Parlamento, che è l'origine del Governo. Invece qui si ragiona completamente alla rovescia, della serie, come dico spesso: siamo un orpello che dà anche un po' fastidio. Tutte queste persone che si alzano e parlano: una noia mortale per il Presidente del Consiglio e per i suoi Ministri. Del resto, quello che dico è provato dai numeri: dei circa 18 miliardi che è la somma dei ristori, il Parlamento si è accapigliato per un tozzo di pane,

tre quarti non ci sono; poi interrompono in maniera garbata. Ho sentito delle sciocchezze, ma sono stato zitto tutta la mattina. Si ragiona in questo modo e voi siete tutti felici e contenti: una cosa meravigliosa. Addirittura ci si preoccupa dell'ostruzionismo e qualcuno ha definito «becera» almeno fateci dire qualcosa. Voi vi date tutte le mattine delle martellate sulle dita per stare zitti e per non dire cosa pensate realmente di questa maggioranza e di questo Governo; almeno fatelo dire a noi. Forse vi siete

Da fine gennaio, quando salterà il blocco dei licenziamenti, ci sarà un milione e mezzo di disoccupati in più, che si vanno a sommare banalmente a quei 15 milioni di disoccupati che già ci sono nel nostro Paese. L'altra notizia è che le imprese che resteranno aperte hanno perso due terzi del fatturato. Per chi non ha mai lavorato un minuto, probabilmente quella che dico è una cosa banale; ma per chi nella vita deve fare i conti con il fine mese, con gli stipendi da pagare e con le responsabilità nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, mi sembra una cosa seria. Però voi avete fatto veramente un'azione importante: vi siete addirittura spesi per una bella marchetta da 5 milioni per i bus scoperti di qualche amico vostro. Ora io dico che bisogna anche essere bravi. Vi devo fare i complimenti perché andare a scovare 150 autobus sui 25.000 bus turistici e schioccargli una bella *fiche* da 5 milioni

l'ho già detto più volte in quest'Aula - che, per quanto riguarda gli stagionali, chi lavorava nove mesi ne ha lavorati quattro, chi ne lavorava quattro ne ha lavorati due

Ristoranti, bar, hotel, negozi, la questione dei balneari è una vergogna assoluta e il Governo fa finta di nulla. Quando gli parli dei balneari si gira dall'altra parte.

Vorrei dare dei numeri, anche se qualcuno penserà che li abbia dati fino adesso, ma credetemi ho cercato sempre di essere aderente alla realtà. Ho sentito nel dibattito dell'altro giorno, di fronte al Presidente del Consiglio, illustri esponenti della maggioranza

che è un bel numero. Sono i numeri che avrebbe un Governo di centrodestra con qualcuno di quelli della maggioranza che probabilmente ha detto: «Perché io farò ...». Noi ci siamo. Siamo pronti. Se volete mandare a casa questo Governo ci sono tutte le condizioni per poterlo fare. E se sono arrivato io a contare fino a 163 ho la sensazione che qualcuno di voi sia in grado, allo stesso modo, di farlo. Prima mandiamo a casa questo Governo e prima, probabilmente, risolveremo i problemi del Paese. Auguri a tutti.

ristori-*quater* del 30 novembre, sono stati messi in campo circa 20 miliardi. Ripassando la storia, di 100 miliardi si è parlato con i decreti cura Italia, rilancio e agosto, il tutto con ben quattro scostamenti di bilancio votati anche da noi delle opposizioni. Ebbene, la prima domanda che vorrei porre è se qualcuno del Governo mi volesse spiegare se qui stiamo facendo sul serio o se stiamo giocando a Monopoli. Lo chiedo perché questa è una domanda che mi viene rivolta tutti i giorni da chi il ristoro lo sta ancora aspettando e da chi non ha ancora visto un euro di cassa integrazione. Parlo di padri e madri di famiglia che, se non fosse per la solidarietà che si è mossa e si muove autonomamente in molte nostre realtà territoriali, a quest'ora non saprebbero come fare per mettere insieme il pranzo con la cena. Non parliamo poi delle partite IVA, costrette a chiudere perché se anche qualcosa è stato fatto, è chiaro che con 600 o 1.000 euro non si possono pagare le spese e in più vivere e noi su questo fronte abbiamo fatto ben più di una proposta. E se anche solo una di queste fosse stata ascoltata, forse molti avrebbero evitato la chiusura dell'attività. Parlo, ad esempio, della moratoria sui mutui bancari, sul rendere immediatamente spendibile il credito di imposta, sulla conversione dei crediti in contributi a fondo perduto, sul cancellare i contributi fissi per gli autonomi, sul rinviare le scadenze di novembre, ma non di dieci giorni, sul tagliare le aliquote IVA, sull'indennizzare i costi fissi delle piccole e medie imprese. Passiamo alla seconda domanda che vorrei porre che riguarda la tanto richiesta collaborazione che voi chiedete alle opposizioni in questo difficile momento. Ecco, io vorrei che voi chiariste cosa significa per voi collaborazione: forse intendete l'accettazione di ogni vostra decisione senza alcuna osservazione o proposta alternativa? assolutamente non può essere, perché collaborare significa ragionare insieme sulle decisioni da prendere, ascoltare la voce dei cittadini e da lì partire per portare avanti delle proposte. Vorrei farvi notare che questo noi della Lega lo abbiamo sempre fatto con molta meticolosità e responsabilità, traducendo poi in emendamenti quelle richieste di salvataggio che ci arrivano dalle famiglie, dai lavoratori, dalle imprese, dai liberi professionisti, dai commercianti, dagli artigiani, da tutti coloro che con molta dignità e determinazione hanno mandato avanti il nostro Paese e ora, con molta vergogna, sono quasi costretti a chiedere la carità allo Stato di cui sono cittadini. Ebbene, le nostre richieste e proposte si sono ridotte in questo decreto a 380 milioni sugli 8 milioni complessivi stanziati con l'ultimo scostamento di bilancio, una briciola in fin dei conti. Non potete certo dire che noi non abbiamo avuto spirito collaborativo e lo dimostrano i fatti. Posso portarvi l'esempio della Commissione di cui faccio parte, la Commissione cultura, in cui come opposizione abbiamo condiviso e votato a favore delle osservazioni e delle raccomandazioni contenute nel parere stilato dai membri della maggioranza, prendendoci l'impegno di trasformarle una ad una in emendamenti. Poco o niente è stato accolto e avete deluso così anche la vostra maggioranza che siede sui banchi di quest'Assemblea e sono sicura che buona parte di essa sia rimasta amareggiata da questo atteggiamento di chiusura alle proposte di tutto il Parlamento, anche quella parte che vi sostiene e non solo quella formata dalle opposizioni. Sempre parlando di collaborazione davanti alla vostra richiesta di segnalare emendamenti che non prevedessero oneri, abbiamo per esempio proposto di derogare alla chiusura di tutte quelle librerie collocate nei centri commerciali, chiaramente svantaggiate rispetto alle altre. No, non si può fare, non si può derogare perché va contro quanto previsto dal DPCM, che in questo modo va a generare discriminazioni tra esercenti della stessa tipologia di prodotti, in questo caso i libri, proprio in un momento in cui poteva esserci un certo guadagno per le librerie.

alle aperture dei luoghi della cultura perché siamo fermamente convinti che con la prenotazione e il contingentamento degli ingressi si poteva evitare la chiusura di musei, biblioteche, cinema e teatri. Neanche questo. Sono questi solo esempi per dirvi che quando parlate di collaborazione, dovete poi specificare di che tipo di collaborazione state parlando, se poi le nostre proposte, onerose o non onerose che siano, vengono sempre puntualmente cassate e dichiarate inammissibili o senza copertura. Non so sinceramente con questo atteggiamento di chiusura nei confronti delle opposizioni dove vogliate arrivare e cosa vogliate far credere agli italiani. So però una cosa: i cittadini italiani non ce la fanno più e hanno bisogno in questo momento di supporto economico, ma ma soprattutto di provvedimenti strutturali che consentano loro di continuare a lavorare perché il lavoro dà dignità e non li rende sudditi del potere. *(Applausi)*.

che si sarebbe presentato dinanzi a noi così aggressivo e senza scrupoli. Il coronavirus ha ribaltato le nostre vite, sconvolgendo abitudini, usi, costumi, consapevolezze, umori,

per contrastare e contenere il contagio. Come abbiamo constatato, il virus corre veloce, ma fortunatamente abbiamo visto all'opera un Governo che ha cercato di rispondere con altrettanta rapidità. velocità certificata dai dati del 7 dicembre del 2020; i contributi a fondo perduto e i ristori erogati dall'Agenzia delle entrate ammontano a più di 9 miliardi, con una platea di beneficiari enorme pari a 2,4 milioni di partite IVA. che il decreto ristori di cui discutiamo vale ben 18 miliardi complessivamente. Si tratta in sostanza di quattro decreti in uno, visto e considerato che dal primo testo varato si sono registrate purtroppo nuove chiusure. Il provvedimento arriva a toccare addirittura 173 tipologie di attività diverse, a riprova di quanto sia deflagrante il coronavirus per il nostro tessuto produttivo. C'è però un comparto tra quelli colpiti sul quale voglio soffermarmi ed è quello del turismo. Un segmento colpito in maniera devastante dal Covid-19; secondo l'Agenzia nazionale del turismo a fine 2020 si registrerà un calo spaventoso di turisti italiani e stranieri pari al 49 per cento rispetto al 2019, con 57 milioni di visitatori in meno e con un tracollo di 186 milioni per quanto riguarda i pernottamenti. Una flessione di spesa turistica nell'ordine di 71 miliardi. Non esiste un ristoro, non esiste una copertura per questi numeri. È inutile continuare a soffiare sul fuoco su un tema del genere. Si sta cercando di affrontarlo. Sono numeri che fanno tremare i polsi e ci danno la misura della catastrofe in cui è stato scaraventato uno dei comparti che negli ultimi anni aveva registrato un segno positivo. *(Applausi).* Per questo, con tutti i limiti del caso, il Governo e la maggioranza hanno prodotto il massimo dello sforzo per dare modo di vivere e proteggersi dall'onda d'urto così violenta che ha investito il turismo. Tra le principali manovre che sono state inserite nel decreto ristori-*quater* vi è l'indennità di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, che si sono visti costretti involontariamente a cessare il rapporto di lavoro in questo periodo. Inoltre, si è voluto dare un'attenzione specifica al segmento relativo alle agenzie viaggi a ai *tour operator,* per i quali si prevedono stanziamenti suppletivi per 400 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi a quelli già stanziati. Vi è poi il bando di 20 milioni destinato destinato al segmento delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici e sono stanziati oltre 100 milioni già destinati al sostegno del settore alberghiero e termale.

Si è tentato di fare il possibile. Questo 2020 nero per il turismo deve però portarci a riflettere sulla necessità di congegnare progetti a lunga gittata con una visione di questo settore così importante, che è troppo spesso trascurato dalla politica nonostante l'espansione e il suo lungo percorso di rinnovamento ancora tutto da completare. Se la riconversione *green* e gli investimenti per la competitività e l'innovazione faranno la parte da leone nel *recovery fund,* il turismo dovrebbe essere messo all'interno di questo grande dibattito per la volontà del percorso da tracciare per i prossimi dieci, venti anni. Personalmente, resto convinto che un'agevolazione epocale come quella del superbonus al 110 per cento per l'efficientamento energetico e il miglioramento antisismico degli edifici vada estesa anche al settore ricettivo e alberghiero, proprio per proiettare definitivamente queste strutture nel terzo millennio. Sarebbe un'opportunità senza pari, ad alto moltiplicatore e spero che il Governo lavori con il massimo sforzo per realizzarla. Oggi però ribadiamo la necessità di portare a casa questo composito decreto-legge come ammortizzatore per reggere l'urto di questo durissimo 2020. Alle chiacchiere abbiamo preferito i fatti e il testo che ci accingiamo licenziare ne è il miglior certificato

cercate di moderare la vostra tirannia, altrimenti, dovessi anche rimetterci la vita, tornerete nella polvere; nel popolo la pazienza comincia a mancare. Queste sono le parole di un magistrato sardo, Francesco Ignazio Mannu, che rappresentò in maniera accorata la ribellione del popolo sardo nel 1794 guidato da altro magistrato, Giovanni Maria Angioy, quando i feudatari sabaudi vennero cacciati dalla Sardegna. Questi versi, che costituiscono l'inno della Sardegna, rappresentano anche un accorato appello in difesa del popolo sardo, perché troppo spesso è stato ed è dimenticato dai governi centrali.

ma lo ha fatto grazie all'apporto che è stato dato dal relatore, dai componenti delle Commissioni e dalla Sottosegretaria che ha seguito tutti i lavori, a cui non posso non rinnovare la mia stima personale ed il ringraziamento per quello che è stato fatto. Tuttavia non posso non sottolineare che, dopo i disastri che ci sono stati in Sardegna a seguito degli eventi che si sono aggiunti ad una situazione già gravissima, con un'economia ormai assolutamente

Noi senatori sardi abbiamo presentato un emendamento, giusto per far fronte in maniera almeno temporanea o comunque emergenziale alla situazione che si è venuta a creare dopo i disastri del 28 novembre. Ci sono state belle parole e cordoglio per le vittime, tanta solidarietà a chiacchiere, ma fatti concreti ancora non se ne sono visti, come peraltro avevo puntualmente previsto nel mio intervento in quest'Aula. Spero non mi si dica che questo provvedimento è destinato ai ristori per fatti legati alla pandemia, perché, come ho detto, i disastri sardi si sono aggiunti alla situazione tragica

Spero che non mi si dica che l'emendamento presentato era inconferente, perché purtroppo devo sottolineare che è questo il disagio nel quale mi trovo quando parlo di questo provvedimento. Infatti, sono stati introdotti emendamenti che di fatto con la pandemia non c'entrano nulla; basti pensare all'emendamento che è stato approvato per consentire a chi aveva già sostenuto due volte l'esame per la nomina a procuratore dello Stato di poterlo sostenere per la terza volta. Si è tentato poi di introdurre, ancora una volta, la possibilità di portare l'età pensionabile dei magistrati da settanta a settantadue anni, mascherandolo con un emendamento analogo, correttissimo e giustissimo, che era destinato ai medici.

sostanzialmente marginalizzato e ad esso sia stata rivolta poca attenzione, con l'approvazione di una serie di emendamenti che, guarda caso, provenivano da una sola forza politica, mentre quelli di buon senso che avevamo proposto noi, che effettivamente avrebbero potuto accorciare e in qualche maniera dare un buon apporto per il miglior funzionamento della giustizia, sono stati tutti disattesi. Mi farò ancora portatore degli interessi e dei bisogni della mia terra. Mi farò ancora

la dovuta attenzione alla Sardegna, che oggettivamente - lo ribadisco - si trova in una situazione di disagio economico mai vista prima di oggi. Mi auguro che il Governo voglia cogliere l'occasione per dare la dimostrazione che noi facciamo ancora parte dell'Italia, ma per quello che ho visto e da quello che è stato annunciato fino ad oggi oggettivamente non mi pare che siamo sulla strada giusta. Quindi, rinnovando rinnovando ancora una volta la stima verso il Sottosegretario che conosco da tempo e so quanto impegno mette nelle cose che fa, chiedo di badare un po' di più alla Sardegna e ai sardi, perché davvero in questo momento ne hanno bisogno, altrimenti sarà difficile continuare a guardare - l'ho già detto in quest'Aula detto in quest'Aula - a un Governo che disattende e si dimentica regolarmente che la Sardegna fa ancora parte dell'Italia. colleghe senatrici, colleghi senatori, rappresentante del Governo, in questi difficili giorni, prossimi alle festività natalizie, siamo chiamati ad esprimerci in merito alle misure adottate da questo Governo nei confronti del sistema produttivo italiano. Per farlo, colleghi, vorrei dare una doppia analisi: una prima che analizzi il problema del breve e medio termine, mentre una seconda che guardi più al futuro. Voglio essere chiaro sin dall'inizio che il tema dei ristori è particolarmente complesso e difficile e in alcun modo non deve rischiare di essere affrontato con la sola finalità di polemica. L'attività imprenditoriale e manifatturiera del nostro Paese è un patrimonio di cui l'Italia deve essere orgogliosa. Siamo una delle economie più importanti al mondo e le nostre capacità manifatturiere ci vengono riconosciute in ogni angolo del globo. Dobbiamo essere altrettanto chiari, gentili colleghi, che l'unico modo che abbiamo per uscire da questa crisi, che peraltro ancora oggi non ha una data certa di scadenza, è il sostegno al mondo imprenditoriale. Un sostegno che non deve trovare differenza tra le grandi aziende e la piccola azienda, tra un settore chimico e un settore agricolo, tra l'artigiano e il commerciante, tra il ristoratore e il parrucchiere: tutte queste categorie oggi, come non mai, hanno la necessità, ma soprattutto il diritto, di essere ascoltate, sostenute ed aiutate. medio termine - e qui affronto il primo punto - non deve significare distribuzione a pioggia di denari, come spesso nei mesi scorsi è accaduto, con inutili, se non pessimi, risultati. Serve un piano immediato, ponderato e ben costruito. Siamo giunti, infatti, a un momento in cui il Paese dev'essere sostenuto sia dal lato dell'offerta sia da quello della domanda dei prodotti. A tal proposito, non posso esimermi dal dire che alcuni provvedimenti adottati dalla vostra agenda politica sono stati pensati andando in quella direzione. Riconosco, infatti, che alcune delle associazioni di categoria del mondo produttivo - non tutte per la verità - hanno accolto anche positivamente quanto da voi proposto. Tuttavia - e qui affronto il secondo punto - ci sono ancora molti aspetti che devono essere chiariti e il Paese, oggi come non mai, ha bisogno di un progetto lungimirante, che guardi ai prossimi anni e alle prossime sfide. L'impressione, talvolta, è che siate troppo impegnati a cercare il modo per arrivare a fine legislatura e non per rilanciare il sistema produttivo per i prossimi anni. proprio oggi, in questi minuti, sta per iniziare nella mia città l'annuale assemblea generale degli industriali bresciani. un appuntamento di primaria importanza, vista anche la vocazione manifatturiera della provincia che ho l'orgoglio di rappresentare in questo Parlamento. L'incontro, cui parteciperanno, tra gli altri, il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli e il ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola, è stato presentato dal presidente Pasini, che parlerà di tre temi che ritiene fondamentali per il mondo imprenditoriale, e cioè la solidarietà, l'impegno e l'orgoglio. mi permetto di rubare questi temi agli amici imprenditori bresciani, perché da qui bisogna ripartire e concentrare la prossima attività economica del Governo. Questa dev'essere l'agenda politica del Paese per i prossimi mesi. Le nostre aziende che oggi non sono in estrema difficoltà negli anni scorsi hanno investito in tecnologia e scommesso sull'innovazione e la ricerca e lo sono ancor meno quelle che hanno avuto la capacità di internazionalizzare la propria attività. Da qui dobbiamo ripartire: dobbiamo pensare alla necessità di sostenere le politiche in grado di proiettare le nostre attività e scommettere sul futuro. Il comparto produttivo chiede sostegni mirati, che permettano alle aziende di continuare a produrre e lavorare con fiducia. Non so a voi, colleghi, ma ciò che tanti imprenditori che frequento mi continuano a chiedere non sono soldi, ma scelte e decisioni coraggiose, che consentano a ogni imprenditore di continuare la propria attività. Nessuno nega l'emergenza sanitaria, ma è ovvio che oggi dobbiamo pensare anche a quella economica e sociale. Come farlo? Per il futuro pensiamo a ristori che abbiano la capacità di sostenere tutte le filiere industriali e non soltanto alcuni particolari settori. Abbiamo visto, infatti, nelle scorse settimane l'esclusione di tante piccole attività commerciali al dettaglio, che in futuro resisteranno sicuramente con estrema difficoltà. È innegabile, infatti, che proprio le realtà più piccole sono oggi le più sofferenti rispetto a un quadro di tutta l'intera economia italiana Queste attività sono quelle che hanno fatto uso massiccio di cassa integrazione, che spesso - anzi, quasi sempre - viene anticipata dalle stesse imprese. È quindi necessario, colleghi, non tralasciare alcun settore, perché un piccolo tassello dimenticato all'interno della filiera manifatturiera potrebbe avere un effetto domino dalle conseguenze devastanti. È necessario avere il coraggio di adottare politiche che stimolino l'attività produttiva e, al contempo, l'incrocio tra domanda e offerta. Solo con scelte coraggiose avremo la possibilità di salvare il mondo produttivo italiano. Non ne va solo della loro sopravvivenza, ma di quella dell'intero nostro Paese Italia.

non per colpa del sottosegretario Guerra qui presente, che stimo da anni, ma perché, sotto il profilo dei ristori, vi sono deficienze enormi. Non c'è alcuna iniziativa specifica sulle imprese che possa contribuire alla crescita economica del nostro Paese. Vi sono poi intere categorie di lavoratori abbandonate, distrutte. Mi riferisco, tanto per fare un esempio,

in Aula. È questa la logica, altrimenti vi è la perdita di dignità non solo dell'Assemblea, non solo di un ramo del Parlamento, ma di ciascuno di noi,

per quanto riguarda specificamente la giustizia e le norme contenute nel provvedimento, grazie ad alcuni emendamenti della maggioranza, si sono serbati alcuni aspetti del processo d'appello,

Vi riporto solo un aspetto. All'inizio della pandemia si è pensato che il giudice dovesse restare presso l'ufficio giudiziario,

Che cosa avviene? Quando c'era soltanto lo scambio di memorie, su questa interpretazione molte volte diventava difficile che ci fosse l'unanimità del collegio.

il Presidente del tribunale a decidere se fare o meno il processo da remoto, oppure che sarà il Parlamento a stabilire se ci sarà o meno la possibilità di fare il processo da remoto. No: dev'esserci la possibilità per il cittadino, in quanto è una libertà fondamentale. Ricordate che il processo si basa sulla disponibilità delle parti, quindi occorre che vi sia una necessità.

in questo nefasto 2020, dominato da un nemico invisibile, il coronavirus o Covid-19, con gravi impatti, a livello sanitario, economico e sociale. Tali provvedimenti, se gestiti con lungimiranza, avrebbero gettato le basi per una radicale, profonda, vera e possibile ripartenza per il nostro Paese, slegata da un altro virus, quello della burocrazia, della lentezza e della mancanza di una visione strategica. Solo per citarne alcuni: sono stati votati un decreto rilancio, ma il rilancio non c'è stato,

qui, che ci osserva, composto da italiani, persone, lavoratori e imprenditori. Ora siamo qui a discutere e votare il decreto ristori, inesorabilmente inefficace, perché lascerà ancora fuori molte categorie, segnalate dalla Lega e dal centrodestra, ma non prese in considerazione da un presuntuoso e vanitoso Capo del Governo, deciso ad annientare i provvedimenti fortemente voluti dalla allora componente di Governo, la Lega, con il suo uomo più potente e forte, Matteo Salvini.

La forte volontà di affondare Matteo Salvini, con ogni strumento e ogni mezzo, è poi sotto gli occhi di tutti, ma non ce la farete: non ve lo permetteremo. Basti pensare che, nel corso delle audizioni, le categorie alle quali ho chiesto personalmente se fossero favorevoli all'anno bianco fiscale hanno risposto tutte di sì. Sarebbe stato un modello di semplificazione, nessuno avrebbe dovuto fare richiesta. Sarebbe stato un modello di ristoro, perché avrebbe coinvolto tutti. Avrebbe avuto le coperture, se non fossero state scialacquate in quelle che alcuni chiamano marchette, ma che io, per non offendere nessuno, chiamerò "pacchette", quelle sulle spalle. L'anno bianco fiscale però arriva dalla Lega, da Matteo Salvini, e il presuntuoso e vanitoso l'ha stroncato sul nascere.

sentito l'intervento del collega Comincini in merito alle misure contenute nel decreto ristori relativamente alle donne vittime di violenza, vi faccio un esempio dell'efficacia e della rapidità di questo Governo. Nel corso dell'esame della scorsa

della Lega e del MoVimento 5 Stelle e introduceva l'obbligo di esposizione del numero antiviolenza 1522. Inserito in legge di bilancio, votato e approvato,

siamo fermi qui, dopo un anno, per definire un cartello, quello del numero antiviolenza 1522, che avrebbe potuto essere preparato anche dall'ultimo dei funzionari della Presidenza del Consiglio

penso che tutti ricordiamo la legge di bilancio del 2018. Fu una grande battaglia, nel corso della quale la Lega *in primis*, insieme all'allora alleato di Governo, cercò in tutti i modi

nel nostro contratto di Governo. Era evidente infatti che per la Germania, la Francia e per altri Paesi dell'Unione europea la linea di galleggiamento entro la quale doveva stare l'Italia era posizionata esattamente un centimetro sotto il nostro

(come stanno dimostrando alcuni in modo particolare), avrebbero dato la possibilità di mettere in sicurezza l'economia nella fase iniziale della pandemia

Di Maio ha detto di voler proporre un anno bianco per le tasse nel 2021. Qua ci vorrebbe un applauso generale, perché noi l'abbiamo detto circa otto mesi fa che andava fatto un anno bianco, che non andavano riscosse le tasse e che prima bisognava mettere in sicurezza il Paese. Vivaddio, ci è arrivato: facciamogli un grande applauso! *(Applausi)*. Mi auguro che il Governo e, in modo particolare, il Ministro dell'economia prendano atto di questa grande intuizione.

Un'altra cosa: il *cashback*. Ieri qualcuno ha fatto una citazione della frase di Osho, straordinaria, perché ve la siete presa con la gente,

Signor Presidente, per la prima volta siamo chiamati a discutere e approvare quattro decreti in uno; un aspetto, questo, che dimostra l'eccezionalità del periodo che stiamo vivendo e che dobbiamo affrontare con determinazione e serietà, in risposta all'emergenza Covid. Il decreto ristori introduce un'ulteriore serie di misure volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali dell'epidemia. Nelle ultime settimane, i colleghi delle Commissioni bilancio e finanze, i relatori, i Presidenti e i Sottosegretari hanno impiegato una parte importante delle loro energie nel tentativo di raggiungere un accordo sulle modifiche da apportare ai testi originari dei decreti-legge.

Negli ultimi mesi sono più volte risuonate le parole del Presidente della Repubblica, che vanno nel senso di una maggiore unità e compattezza in questo momento così complicato e doloroso della nostra storia. Quelle parole del Presidente della Repubblica devono essere un monito per tutti noi, soprattutto per coloro che nelle ultime settimane sono stati tentati dalla via della strumentalizzazione delle difficoltà del Paese per finalità che - ormai è evidente - esulano dalla reale volontà di portare un contributo al lavoro del Governo e del Parlamento. *(Applausi)*. La definizione di questo provvedimento deve invece costituire l'avvio di un nuovo percorso di condivisione nelle scelte politiche per il superamento delle difficoltà dei tanti. Le misure introdotte dal decreto-legge in discussione, a partire dai ristori, sono rivolte proprio ai settori maggiormente colpiti dalle restrizioni governative. L'urgenza di ristorare le imprese che hanno subito le restrizioni pandemiche ha determinato purtroppo l'esclusione di tante altre imprese con diversi codici Ateco. Per queste imprese il Governo ha pensato, per il prossimo decreto-legge ristori, a un fondo di perequazione che superi il sistema dei codici Ateco, per ricomprendere tutti coloro che hanno registrato un calo del fatturato nell'anno 2020, anche e soprattutto quelle imprese rimaste fuori dai ristori previsti da questo provvedimento. Il collega che è intervenuto poco fa ha parlato dell'idea dell'anno bianco. Vorrei dire che l'anno bianco fiscale è nei fatti. Il problema delle imprese nel 2020 non sono state le imposte, ma la sopravvivenza. Per questo, anche il Governo

La crisi ha fatto emergere ancora di più il divario tra coloro che possono contare su un reddito fisso e sicuro e quei soggetti, come le imprese o le partite IVA, che invece vivono dell'incasso giornaliero e non hanno le stesse garanzie e tutele dei primi. Questa situazione ci impone scelte ben precise: dobbiamo prevedere forme di *welfare* strutturali anche per le nostre partite IVA e nella manovra in corso di esame alla Camera, grazie anche all'impegno del MoVimento 5 Stelle, si sta delineando un'importante soluzione in tal senso, sia per garantire un po' di più le nostre partite IVA, sia per alleggerire il carico dei versamenti a cui sono tenute. Non dobbiamo più permettere che proprio coloro che da sempre hanno contribuito allo sviluppo del Paese e al sostegno dello Stato possano restare privi di protezione economica in caso di crisi o di assenza di reddito. È altresì necessario ristabilire un principio di giustizia fiscale, prevedendo nuove forme di prelievo nei confronti di quei colossi digitali che si fanno scudo dell'extraterritorialità delle loro sedi per celare i redditi conseguiti nel nostro Paese. Sulla *digital tax* non possiamo restare appesi all'attesa di incerti accordi internazionali, come quelli che si attendono in sede OCSE, sotto il ricatto di ritorsione nei confronti delle nostre imprese esportatrici. Dobbiamo agire comunque e subito per salvare le nostre imprese, certi che, insieme agli altri Stati europei a noi più vicini e simili, possiamo opporre alle minacce di ritorsione una forza contrattuale enorme data anche dal valore dei profitti conseguiti da questi colossi nel nostro territorio e dal valore economico enorme dei nostri dati digitali. Dobbiamo insomma sfruttare la contingenza della pandemia per creare una società moderna, più giusta e inclusiva. Il raggiungimento di questo risultato, però, passa anche dall'unità e dalla serietà che la politica deve saper dimostrare. Per questo, credo e ribadisco che l'accordo sulla conversione del decreto-legge ristori deve costituire l'avvio di un nuovo percorso politico di unità, come ci ha ricordato il Presidente della Repubblica, per il rispetto dei diritti dei cittadini e per il superamento dei divari sociali. *(Applausi)*.

sui ristori, a nome di Fratelli d'Italia, sono già intervenuti i colleghi Nastri, Maffoni e Petrenga, quindi, come componente della Commissione giustizia, voglio intrattenermi sul capitolo degli interventi in tale ambito contenuti all'interno dei quattro decreti-legge che oggi esaminiamo per la conversione.

le categorie interessate, e finalmente il Governo si è svegliato e ha introdotto questa semplice possibilità, che non si capisce perché non fosse prevista in precedenza, per il deposito degli atti penali. Siamo invece contrari e particolarmente preoccupati per il trattamento cartolare dell'appello penale che viene introdotto con questa misura e non parliamo poi della discussione della causa in sede di Cassazione. Praticamente quello che era un cardine da sempre fondamentale del processo penale, cioè l'oralità, viene trasformato in un criterio residuale, soltanto in casi particolari e su richiesta di parte. Questo, secondo noi, è molto preoccupante e siamo assai contrari.

la condizione prevista dalla norma generale che viene derogata, è stato semplicemente ignorato, come tantissimi altri di quelli che abbiamo presentato. presentato. Risultato: gli unici che restano davvero condannati nel sistema carcerario italiano sono gli agenti di custodia, che vengono tartassati, mandati allo sbaraglio, costretti a turni massacranti (perché sappiamo che l'organico è deficitario di quasi diecimila agenti), senza strumenti e a volte senza nemmeno le mascherine. Ecco, i veri condannati nel nostro sistema carcerario sono gli agenti di custodia, cui va tutta la nostra solidarietà. Quello che più manca in questi quattro decreti-legge, però, è qualsiasi misura a favore della magistratura onoraria. Avete ignorato un mio emendamento relativo ai magistrati onorari, che, come tutti sappiamo, sono privi di qualsiasi tutela, vengono pagati a cottimo e quindi con il rinvio delle udienze chiaramente sono in grosse difficoltà, perché non percepiscono emolumenti. Avevamo proposto di riconoscere loro almeno un indennizzo di 1.500 euro al mese per tutta la durata dell'emergenza. Anche questo nostro emendamento è stato ignorato. È proprio sulla magistratura onoraria che vorrei richiamare l'attenzione di quest'Assemblea, perché, come tutti leggiamo sui giornali, è in corso una protesta molto molto forte da parte dei magistrati onorari, che lamentano - giustamente di lavorare senza alcuna tutela. Per loro non ci sono ferie né diritti, non c'è il riconoscimento della maternità

non riconosciamo la malattia professionale, come avviene anche per le altre malattie, perché il magistrato onorario non ha alcuna tutela nel nostro ordinamento giuridico. Sono dei paria, Sono dei paria, servitori dello Stato che si sacrificano e tengono sulle loro spalle il 50 per cento e più di tutti gli affari che vengono trattati di fronte ai nostri uffici giudiziari, ma non hanno diritti per il nostro Stato e per il Governo. Questo è veramente vergognoso. Credo che questi cinquemila servitori dello Stato meriterebbero ben altro, come ha del resto riconosciuto la Corte di giustizia europea e come sta riconoscendo finalmente la stessa Associazione nazionale dei magistrati che in questi giorni sta facendo uscire comunicati su comunicati in cui riconosce finalmente che senza i magistrati onorari la giustizia semplicemente si blocca. Sappiamo tutti benissimo che il 90 dei processi penali davanti al giudice monocratico del tribunale si tengono grazie ai vice procuratori onorari, perché altrimenti si bloccherebbe tutto, tant'è vero che in alcune procure i procuratori hanno deciso di andare in udienza proprio come forma di solidarietà nei confronti dei magistrati onorari. Ebbene, di fronte a questa situazione drammatica come risponde il ministro Bonafede? Risponde dicendo che questo trattamento vergognoso dei magistrati onorari è necessario, perché altrimenti la magistratura professionale subirebbe la perdita di prestigio e la riduzione della retribuzione. Lo ha detto il ministro Bonafede non a «Porta a porta», ma in un atto ufficiale, rispondendo a un'interrogazione alla Camera del mio collega di partito, l'onorevole Delmastro di Fratelli d'Italia. È una risposta vergognosa, dalla quale hanno preso le distanze persino gli stessi magistrati professionali, perché badate bene, questa non è una delle tante *gaffe* del ministro a «Porta a porta», ma è un'affermazione contenuta in un atto ufficiale del Governo di fronte al Parlamento.

Scusate la sintassi, non è mia, è del Ministro, che ho citato testualmente. Questa non è una *gaffe*, è un atto ufficiale di fronte al Parlamento e credo che da questo punto di vista sia davvero inaccettabile che in ben quattro decreti-legge si sia totalmente ignorata la situazione dei magistrati onorari. Credo che non ci rendiamo davvero conto che se non risolviamo, anche con un decreto-legge,

i pubblici ministeri in udienza e quindi con la paralisi totale delle indagini da parte dei pubblici ministeri. Non ci rendiamo conto che oggi l'ufficio del giudice di pace non è più quello che una volta era il conciliatore, ma è diventato di fatto una vera e propria sezione del tribunale, che tratta affari anche importanti, soprattutto in materia civile, ma anche in materia penale. Tratta, ad esempio, tutta la materia relativa all'espulsione degli immigrati, tratta questioni importanti e fondamentali, perché quelli che vengono definiti i reati bagatellari, reati di seconda importanza, in realtà per chi li subisce sono reati importanti e il giudice onorario di pace aiuta la giustizia a dare risposta alla domanda di giustizia del cittadino, che altrimenti non la vedrebbe soddisfatta. Per tutte queste ragioni, caro Presidente, credo sia importante che questa Assemblea oggi prenda atto dell'importanza di rispondere il più presto possibile alla domanda di giustizia di questi servitori dello Stato che sono stati troppo a lungo mortificati e invito il Governo, tramite il Sottosegretario, a dare finalmente e al più presto nel prossimo decreto-legge ristori o con un decreto-legge *ad hoc* la risposta che stanno aspettando da troppo tempo. *(Applausi)*.

ragione, la legge di bilancio, che arriverà a fine anno in Senato. Sono tutti provvedimenti connotati e caratterizzati dalla data certa. Di fatto, però, cosa si dimostra con il decreto ristori e gli altri provvedimenti? Si dimostra che il sistema bicamerale paritario è stato in realtà trasformato di fatto in un monocameralismo a senso unico alternato.

allo stesso modo, ma in senso inverso, ci è arrivato il decreto sicurezza; sostanzialmente bloccato, inemendabile e prossimo alla scadenza. Così arriverà anche la legge di bilancio. Ciò comporta un vero e proprio svuotamento del ruolo del Parlamento e del mandato stesso del parlamentare. In pratica, a questo punto, è vera ipocrisia continuare a fare menzione della centralità del Parlamento. Noi stiamo assistendo, in realtà, *apertis verbis*, ad una vera e propria esternalizzazione del procedimento democratico attraverso *task-force* e cabine di regia. A ciò si aggiunge l'ulteriore abitudine di "invagonare" - mi sia consentito questo termine - dietro un decreto-legge, caratterizzato da requisiti specifici di necessità e urgenza, norme ad esso del tutto estranee.

professori universitari, avvocati dello Stato e magistrati. L'emergenza sanitaria può giustificare ovviamente il richiamo in servizio dei medici, ma per quanto riguarda i professori universitari e i magistrati, le norme ordinamentali, per evitare di interferire nelle legittime aspettative esistenti, dovrebbero essere il più possibile stabili e disciplinare un futuro non immediato. Per quanto riguarda i magistrati, inoltre, è chiaro che, trattandosi di un altro potere dello Stato, bisognerebbe smetterla di giocare con l'asticella del limite d'età. Ricordo che il Governo Berlusconi ha innalzato il

perché è fin troppo evidente che si tratta di una selezione dei capi degli uffici giudiziari. È uno strumento con cui si violenta l'indipendenza della magistratura con un controllo politico inaccettabile.

noi dobbiamo ricordare due cose. Primo: il citato emendamento era stato annunciato a dicembre del 2018, quando del Covid non se ne parlava, ed è stato presentato varie volte, anche in assenza di Covid. Tutto questo, mentre - come ha ben detto il collega ed io eviterò di ripetere

di esigenze insopprimibili di tutela del lavoro. Non c'è invece alcuna urgenza di selezionare politicamente i capi degli uffici giudiziari. Il contenuto dell'emendamento è del tutto estraneo agli indennizzi, ai ristori, alle necessità della gente.

che la prassi di far seguire emendamenti impertinenti rispetto al testo deve cessare. Il riferimento al Covid non basta

problema. Quando prendete il tempo e lo dividete in cinque minuti, non è poi possibile andare oltre il settimo minuto, altrimenti è un'ingiustizia verso i Gruppi che

le tasse per chi è stato più colpito da questa pandemia. Noi ristoriamo chi ha perso il lavoro, però vorrei anche gli interventi che riguardano le persone più deboli, gli invisibili, chi in questi anni ha più subito e rischia di subire ancora di più da questa crisi i danni di un aumento delle distanze e delle differenze sociali. 400 milioni per i Comuni, per il fondo per gli incapienti e la proroga del reddito di emergenza sono provvedimenti importanti che credo vadano sottolineati: ci si deve occupare di tutti e abbiamo tentato di occuparci di tutti, perché lo *slogan* che nessuno deve essere lasciato solo non può restare soltanto sulla carta. Signor Presidente, concentrerò brevemente il mio intervento su un tema che riguarda anche in

chiaro a tutti che qualunque istituzione in cui le persone sono concentrate presta di più il fianco alla diffusione del *virus* e del contagio.

140 hanno sintomi. Quindi, la situazione è seria ma non è fuori controllo, anche grazie al lavoro fatto in in questi mesi dai direttori, dalle maestranze, dagli operatori sanitari, dagli operatori delle carceri e soprattutto dagli agenti di custodia. Grazie a quel lavoro si è contenuto il contagio, ma grazie anche ai provvedimenti presi dal Governo all'inizio della pandemia e oggi riproposti. Li ricordo perché sento cose assolutamente non vere: non c'è stato alcuno svuota-carceri, non c'è stata alcuna persona ci sono stati gli arresti domiciliari per molti; si è intervenuto e si deve intervenire meglio e di più per ridurre le pressioni e le presenze Ci vuole un'attenzione maggiore per tutelare la salute dei carcerati. Abbiamo detto in questi mesi, insieme a tanti operatori, insieme ai ai garanti regionali e al Garante nazionale, insieme a tante associazioni, che si deve e si può fare di più, anche rispetto a quello che già il Governo ha fatto e che è contenuto in questo decreto. decreto. La popolazione carceraria è ancora troppo alta rispetto alla ricettività; non ci sono spazi per il distanziamento all'interno degli istituti di pena; non ci sono spazi di isolamento ed è difficile trovare il modo di curare le persone e di metterle in sicurezza. L'approvazione del decreto al nostro esame e di alcuni emendamenti migliora la situazione. Noi avremmo voluto di più, lo dico e lo dirò: avremmo voluto il blocco delle esecuzioni delle condanne che passano in giudicato in questo periodo per non far entrare

ha avuto un percorso positivo e per chi ha vissuto bene e con buona condotta la propria esperienza in carcere. delle condizioni nelle carceri, di chi è recluso e di chi opera nelle carceri penso sia un tema molto serio e la condizione perché si risolva è che ci sia una minore pressione. È bene che nel *recovery fund*, nel programma del Governo, siano già previste risorse per migliorare gli spazi di detenzione e per difendere la salute, così come spazi adeguati per la formazione e il lavoro. Il Governo, il Parlamento e la politica hanno il dovere di rispettare il dettato costituzionale, che è sicuramente quello di garantire la certezza della pena, ma anche il rispetto della salute delle persone detenute. Chi pensa alla pena come alla vendetta e non alla rieducazione e al reinserimento, chi agita le paure - come ho sentito fare oggi - evocando lo svuota-carceri, chi fa propaganda su delle persone evocando la necessità di buttare via le chiavi se qualcuno ha sbagliato, crea le condizioni perché il carcere diventi un moltiplicatore di violenza e di criminalità. modo si mette ancora di più a rischio la sicurezza di tutti. Su questo argomento il provvedimento che stiamo votando non è come l'avremmo voluto, ma fa un passo avanti: non mette in discussione la certezza della pena, né libera nessuno, come state raccontando, ma afferma un principio, quello per cui la politica deve agire per tutelare la salute di chi sta in carcere e perché la detenzione non sia solo sofferenza, ma diventi un'opportunità.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, relatori, un grazie particolare va ai membri della 5a della 6a Commissione,

All'origine erano interventi sui codici Ateco, incrementativi con i vari ristori: congedi, congedi *baby sitter*, stop all'IMU, credito d'imposta per tre mesi d'affitto ottobre-novembre-dicembre, ma anche 300 milioni per il sistema dei trasporti e 250 milioni per le Regioni. Peraltro, stiamo parlando di decreti

invece in considerazione altri criteri. Forza Italia e il centrodestra hanno contribuito con loro proposte particolari e con

l'avvio di un processo di accompagnamento del cambiamento del sistema dei trasporti e di risposta sul sistema dei trasporti. Gli indicatori

La realtà della Calabria non è la stessa dell'Umbria o del Piemonte, per cui dovrà essere dato uno spazio, regolato e non disordinato, a interventi puntuali da parte del sistema regionale.

gravissima situazione è anche l'occasione per intervenire sulle procedure e per regolare i troppi poteri che immobilizzano il sistema. Dobbiamo stare certamente attenti ai ladri, ma mi mi permetto di citare il TAR, il caso della Puglia, che, con due decisioni su due Province diverse sulla questione del *lockdown*, è significativo. Corte dei conti, timbri, monitoraggi, tribunali civili: ieri il collega Dal Mas ci ha ricordato che da noi i processi civili durano mediamente più del doppio della media degli altri Paesi europei. Monitoraggi, statistiche, ordinaria burocrazia, di cui noi siamo parte, da cui non possiamo tirarci fuori e a cui molte volte abbiamo contribuito. Un esempio del noi, citato ieri dalla collega Toffanin, è quello del microcredito. Nel decreto liquidità

il dovere di passare dalla bombola dell'ossigeno all'ossigeno respirato direttamente dalla nostra società a seguito della situazione che si è creata,

Servono riforme per farci diventare un Paese moderno. D'altra parte, nel diventare Paese moderno, chiaramente la mia parte politica dice che non possiamo risolvere tutte le crisi con la statalizzazione. Dobbiamo produrre margini. L'indagine di Banca d'Italia, che mette alcune città in testa alla classifica per risparmi,

significa anche che le imprese non investono; e, se non si investe, non si coglie lo snodo che ci sarà con il *recovery fund* e che dovrà permettere all'Italia

È un impegno che noi chiediamo al Governo ed è un impegno importante per far uscire il Paese da questa condizione. *(Applausi)*. Signor Presidente, è possibile fare una sintesi di due giorni di intervento? Sì, con toni e accenti diversi riferiti al provvedimento, almeno su un punto siamo tutti d'accordo:

Sia chiaro: questo non toglie nulla all'impegno positivo sul singolo emendamento, che magari ci ha visto tutti impegnarci insieme. Potrei citare l'emendamento che ha portato ad escludere dal pignoramento, i contributi per la ricostruzione; emendamento che, senza un impegno di tutti, non sarebbe passato. Non è però un singolo

gli spesometri e gli studi di settore, e poi, quando c'è da dare i contributi, a qualcuno si danno le elemosine, tipo i 600 euro. È questo che non va bene.

tutte le categorie definite da quei famigerati i codici Ateco, che sono state escluse. Dietro ognuna di quelle siglette, però, ci sono migliaia di aziende e centinaia di migliaia di persone. Senatore Rampi, è difficile? No, è facilissimo, perché il criterio è di considerare chi ha avuto un danno, diretto o indiretto, dal Covid. Non possiamo ristorare i ristoratori - scusate il bisticcio di parole - e magari non i grossisti del comparto Horeca che ai ristoratori vendono. Si tratta di un danno indiretto, ma assolutamente evidente e molti

le attività economiche dei centri storici delle città d'arte a vocazione turistica. Chi ha un'attività economica e magari vende prodotti artistici e non cineserie ha un danno economico, perché mancano i turisti, tanto che il suo Comune sia un capoluogo di Provincia quanto che sia un Comune normale, che magari ospita centinaia di migliaia o milioni di turisti. Vi sembra normale che Comuni come Assisi o Sorrento - ma potrei citarne per tutta l'Italia e non mi basterebbe il pomeriggio - siano esclusi per il solo fatto di non essere capoluogo di Provincia? Questa è un'ingiustizia all'interno di un'indicazione valida e positiva - perché non riconoscerlo? - da parte del ministro Franceschini, ma che esclude, a fronte di 29 città comprese, migliaia di Comuni italiani, comunque turistici. Allo stesso modo va benissimo aver dato un contributo alle città delle grotte, che magari hanno avuto meno turisti: per 20 Comuni sono

evidenti nel provvedimento in esame. Si dirà che mancavano i fondi, ma noi - come abbiamo detto - siamo disponibili a un ulteriore scostamento di bilancio, purché le risorse siano impegnate costruttivamente e senza distinzioni. Avete preferito utilizzare i fondi avanzati dai decreti-legge precedenti e questo già la dice lunga su come sono andate le misure, se ci sono addirittura miliardi di euro non utilizzati che vengono reimpiegati. Concludo con un ultimo esempio: avete dato qualche volta il necessario, qualche volta il superfluo, ma ad alcuni non è stato dato l'indispensabile. Penso alle persone che andavano ristorate per la distanza dagli affetti e ai lavoratori fragili. Avete prorogato le licenze premio e non avete trovato il modo di equiparare l'assenza dal lavoro per i lavoratori fragili, che rischiano la vita, se sono a contatto con persone contagiate, per andare a lavorare. degli abbracci. Il senatore Santillo ha mandato un abbraccio a distanza ai nostri anziani, ma noi avremmo voluto darglielo fisicamente. Troviamo allora le risorse per intervenire in questa direzione. Non a noi, ma a quelle persone dovete chiedere scusa,

lo spera tanto. Ci sono delle volte in cui il tempo fa la differenza: c'è la legge di bilancio: troviamo insieme il modo di ristorare emotivamente quelle persone e non lasciamole sole. Qualche volta quello che per noi è poco è per altri tutto. Facciamolo con il prossimo provvedimento.

sono veramente felice del lavoro che è stato fatto sul provvedimento in esame. Sono state fatte molte riunioni, telefonate e *videocall* giornaliere per non lasciare indietro nessuno e, alla fine, ce l'abbiamo fatta. Ciò che provo è un sentimento di fatica positiva, quella che si prova alla fine di una gara molto dura, ma che conferma il fatto di avercela messa tutta. Purtroppo non tutti in quest'Aula possono dire lo stesso: c'è chi ha lavorato instancabilmente e chi invece troppo spesso utilizza provvedimenti emergenziali come questo per alimentare la propria voglia di propaganda elettorale continua. Possiamo pensare ad alcuni *leader* politici come agli studenti di una scuola. Penso che la metafora calzi a pennello in riferimento alla situazione contingente che si sta delineando nello scenario politico italiano. Assegnate voi i ruoli, io non farò i nomi. Abbiamo l'arrogante con la sua cricca, più avvezzo a gonfiarsi il petto a parole che per fatti concreti. Abbiamo l'alunno bravino, ma che si impegna poco; il professore crede in lui, ma deve rincorrerlo sempre. Abbiamo purtroppo anche quello capace, ma molto insolente, che crede di sapere più dello stesso professore, cosa che lo porta poi sulla strada sbagliata e a compiere scelte figlie dell'errato dimensionamento delle proprie capacità. Tutti questi ragazzi - metaforicamente parlando ovviamente - nelle ultime settimane stanno mettendo in scena una gazzarra politica futile per il Paese e sinceramente anche incomprensibile. Sembra ogni giorno un'urlante assemblea d'istituto, per continuare con metafore sempre prese dall'ambito scolastico. Solo che qui non sono in gioco solo le dinamiche interne della scuola: qui è in gioco l'intero futuro del nostro Paese. venissero a dire che è il gioco delle parti, perché questo non è il momento. Non ci sto! *(Applausi)*. Abbiamo oltre 65.000 morti, famiglie distrutte, imprese in difficoltà. Ora basta, dico basta: occorre responsabilità. Torniamo però alla realtà e ai problemi evidenti e tangibili che questa emergenza ha portato con sé. Il testo di cui stiamo discutendo oggi supporta economicamente decine di settori economici, lavorativi e produttivi che altrimenti non avrebbero trovato la forza di resistere e che sarebbero finiti in un baratro. Ovviamente noi abbiamo fatto e stiamo facendo di tutto, ma chi da quei banchi - e mi rivolgo a chi è seduto verso la mia sinistra - ogni giorno urla contro il buon lavoro di questo Governo spinge sempre di più le nostre aziende e i nostri cittadini proprio verso quel baratro. Ci sono stati appelli a una trasversalità parlamentare nei lavori di questi mesi; appelli a un senso dello Stato che chi occupa questi scranni in Parlamento dovrebbe avere; richieste tutte cadute nel vuoto, tutte diventate parole al vento. Il testo che voteremo è il frutto di un intenso lavoro sinergico tra il Governo, le imprese, i lavoratori e le parti sociali. Abbiamo rafforzato la rete di protezione predisposta con i precedenti provvedimenti a favore delle categorie più vulnerabili e penalizzate dalle necessarie restrizioni; un sostegno questa volta mirato ai settori economici più colpiti, mediante un contributo a fondo perduto diretto incrementato fino al 400 per cento rispetto al passato. Non abbiamo lasciato indietro nessuno, disponendo misure specifiche a favore delle aziende operanti nelle filiere agricole e della pesca, senza dimenticare però, in una prospettiva di lungo corso, di sostenere l'*export* e l'internalizzazione delle nostre imprese mediante l'erogazione di crediti agevolati. Il fulcro del provvedimento, in particolare del cosiddetto ristori-*quater*, consta poi di una serie di proroghe fiscali finalizzate a dare ossigeno al nostro tessuto economico-produttivo; tra le altre, la proroga dei termini di versamento dell'Ires, Abbiamo inoltre cancellato la rata IMU e introdotto un fondo perequativo volto a concedere un esonero totale o parziale dei versamenti contributivi e fiscali attivo a favore di quelle attività che hanno subito una significativa perdita di fatturato. Tra le tante proroghe disposte, meritano un cenno quelle della cassa integrazione e il differimento del termine del blocco dei licenziamenti che, unitamente al reddito di emergenza, si inseriscono nell'ambito delle misure disposte a sostegno delle famiglie e delle fasce più fragili. Ricordate? Nessuno verrà lasciato indietro. Non era solo uno slogan *(Applausi)*, ma stiamo cercando costantemente di tradurlo in fatti concreti. Per tornare alla scuola, abbiamo messo in campo ulteriori risorse per l'innovazione digitale e la didattica a distanza, al fine di consentire a tutti gli studenti di proseguire il proprio percorso formativo, garantendo al contempo ai genitori strumenti per conciliare il lavoro alle rinnovate esigenze familiari mediante strumenti quali lo *smart working* e il congedo. Attenzione: questi interventi per sostenere le famiglie italiane sono solo il preambolo ad interventi via via più incisivi. Ricordo che l'assegno unico partirà proprio il prossimo anno. Infine, voglio soffermarmi anche sullo sforzo straordinario delle nostre Forze dell'ordine, chiamate a garantire l'incolumità pubblica in questa delicata fase di contenimento del contagio. Abbiamo messo in campo ulteriori risorse volte a retribuire il loro encomiabile lavoro. Ho esordito in questo discorso plaudendo al lavoro lungo e molto duro portato a termine. Chi è mancato in questo interlocuzione è solo che ha scelto scientemente di non farne parte.

Concludo ringraziando tutti gli uffici che ci hanno supportato e ci supportano durante i lavori, i colleghi delle Commissioni bilancio e finanze, i relatori, i sottosegretari Castaldi e Guerra per la costanza, la pazienza e la dedizione mostrate durante l'esame del provvedimento, il cui testo arriva oggi in Aula arricchito e migliorato rispetto a quello di partenza. Ciò che abbiamo fatto non solo negli ultimi mesi, ma in tutto questo ultimo anno, il modo in cui stiamo affrontando la più grande crisi economica del dopoguerra, sarà il più prezioso dei tesori che potremo lasciare alle nuove generazioni, nella speranza che - ne sono sicura - i prossimi due anni della XVIII legislatura saranno la base per costruire un Paese più inclusivo, tecnologicamente avanzato e votato all'equità sociale e di genere.

interessanti, ma devo dire in alcuni casi fuori luogo, e fuori luogo perché dobbiamo ricordarci che ci stiamo muovendo in un contesto di pandemia mondiale; una pandemia che ha generato un'emergenza sanitaria e una economica rispetto alla quale non vi è una soluzione, non c'è una bacchetta magica con la quale intervenire e risolvere i problemi che stanno mettendo a dura prova l'Italia, e non solo. Il

un'idea, una genialata del Governo: è stata la necessità di rispondere a una seconda ondata di contagio che ha determinato due DPCM con misure restrittive necessarie per tutelare la salute degli italiani. Da queste misure restrittive sono generate delle conseguenze di natura economica, e non solo: anche organizzative di alcuni apparati dello Stato come la giustizia e la scuola. Si tratta di argomenti che stiamo affrontando

Dobbiamo tenere conto anche di un'altra cosa: le risposte che sono state date e che bisogna dare ai cittadini devono essere veloci ed efficaci, e questo all'interno di un'attività ordinaria dello Stato che, soprattutto in questo periodo, sta vedendo alla Camera la discussione del bilancio.

aventi una importanza strategica fondamentale. È vero: ci sarà il decreto ristori cinque ma - lo ripeto - è un'esigenza governativa, e del Parlamento in questo caso, tenere conto di variabili economiche che mutano in conseguenza di aspetti sanitari che stanno condizionando l'attività politica dello Stato in funzione delle esigenze del territorio. Ritengo però che non sia giusto dire che il Governo non abbia o non abbia avuto una visione. La visione c'è stata fin dal primo momento e continuerà ad esserci. ad esserci. Aggiungo che abbiamo lavorato, insieme al collega Marino, in tutte le varie fasi di questa trattativa che è stata soprattutto accompagnata, prima di entrare in Commissione, da un continuo confronto con le opposizioni. La collaborazione c'è stata, altrimenti questo provvedimento, che non serve alla maggioranza ma al Paese, oggi avrebbe avuto difficoltà nella sua discussione.

di unità nazionale rispetto un'emergenza che non ha colore politico, che non ha differenza geografica. *(Applausi)*. Oggi il Parlamento sta dando una risposta univoca alla Nazione ed è anche merito vostro.

sono tutti emendamenti che hanno una legittimità nazionale condivisibile. Oggi quest'Aula sta dando una risposta all'Italia veramente onorevole per tutti

e dopo ci sarà il *recovery plan*. Per il rilancio del Paese gli italiani vogliono certezze. Non vogliono contrapposizioni politiche. *(Applausi)*. Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, signor Ministro, dispiace avere cinque minuti di replica di fronte a un dibattito lungo e articolato, anche perché lo abbiamo seguito e, quindi, sarebbe una forma di rispetto poter replicare ai colleghi. Vorrei che questi quindici secondi non mi venissero computati, ma chiedo che nella prossima Conferenza dei Capigruppo si tenesse conto anche della divaricazione dei ruoli proprio in funzione del rispetto che si porta ai colleghi quando si ascoltano e si ritiene che, magari, si debba anche replicare. Dispiace che elementi di polemica, alcuni anche non proprio civili, abbiano travalicato quel necessario senso di comunità di cui ha bisogno il nostro Paese in questo momento e cui accennava molto bene collega il collega Presutto. Dispiace - come dissi in Commissione - che vi siano momenti in cui ci si dà del "tu" e momenti in cui ci si dà del "lei". Scherzando in maniera umoristica il collega di Bertoldi dice che ci sono anche momenti in cui ci si dà del "voi". Pensavo che l'accordo potesse farci ritornare a quel "tu" in maniera costruttiva, e invece alcuni hanno impostato il dialogo con un "lei" talora altezzoso, scostante e non proprio molto disponente.

ma di una di tripartizione che non è quella dello spirito delle leggi di Montesquieu, ma che è quella del rapporto fra Governo, maggioranza e minoranza. Pensavo ad una narrazione positiva cui dare seguito anche nel ristori cinque, perché questa è stata parte del dibattito che abbiamo sviluppato. In alcuni casi, invece, c'è stata una *summa* di critiche un po' ingenerose, nonostante i milioni fossero passati da 600 a 620 a 620 e in questa ripartizione vi fosse stata la divisione di 380 per l'opposizione e 240 per la maggioranza, che si capisce proprio nella logica della tripartizione e non nella logica complessiva, perché il Parlamento è una cosa e il Governo - che pur è appoggiato da una maggioranza - è una cosa diversa. una cosa diversa. Su quelle risorse a disposizione si sono dovute fare delle scelte che sono state dettate dalla velocità e dall'importanza, e cioè per una volta si è tenuto in considerazione insieme sia ciò che è urgente, sia ciò che è importante, che di solito sono due categorie dello spirito su cui si tende un po' a confondersi. Personalmente ho molto apprezzato la proposta avanzata nel dibattito generale del senatore Bergesio di 100 milioni per le filiere alimentari, come ho apprezzato quella della senatrice Cantù di 100 milioni per sostenere i bisogni dei sanitari o quella non quantificata della senatrice Nisini sui lavoratori fragili. Bisogna però fare delle scelte: la politica è anche assumersi la responsabilità delle scelte fatte e devo dire che anche noi della maggioranza avremmo potuto avanzare delle proposte su come spendere bene quei 380 milioni.

rispetto ai Comuni montani, quelli più abbandonati e più difficili da gestire. Ma ce ne sono alcune di importanza e rilievo come quelle per le abitazioni, e le cifre sono significative e importanti. Ribadisco che questo è l'inizio di un percorso che dovrà approdare a qualcosa di diverso. Va tutto bene? No, voglio essere

C'è un problema strutturale, però, che voglio denunciare in conclusione, che merita una riflessione autonoma: come legislatori abbiamo posto in essere una normativa emergenziale a cui non sempre è stata data dalla burocrazia sottostante una risposta all'altezza delle nostre aspettative, perché in alcuni casi c'era una *forma mentis* non adeguata.

portandoci a un livello di sistematizzazione, di organicità della trattazione di tutte queste materie di cui c'è assolutamente bisogno e di cui sono convinto saremo all'altezza.

ho ascoltato attentamente i vostri interventi e soprattutto quelli di maggioranza - a me piace ascoltare - e ho colto tante lodi a questo provvedimento, tanta autocelebrazione e poche critiche devo dire -a parte qualche caso. caso. Vi ricordo, colleghi, che l'opposizione ha assunto un atteggiamento costruttivo, non ostruzionistico, senatore Dell'Olio.

il ricorso al calcolo del contributo a fondo perduto con il rapporto aprile 2020 su aprile 2019. Contestiamo il ricorso ai codici Ateco, che ha escluso ingiustamente tante categorie fortemente colpite dalle chiusure. Per noi era giusta una logica di filiera, era quella la logica da adottare. Contestiamo le proroghe arrivate troppo tardi, oppure non arrivate. Contestiamo le tante, troppe anomalie e contraddizioni,

Conoscete anche voi queste distorsioni. Perché non avete accolto - ad esempio - il nostro emendamento sull'armonizzazione dell'IVA per l'asporto? Non voglio pensare che si voglia far cassa sulla pelle dei ristoratori e sugli ignari cittadini.

anche le forze di maggioranza hanno votato contrariamente al loro stesso emendamento. Si trattava di un emendamento che non costava niente e avrebbe sollevato i nostri commercianti già in grave crisi da un'ulteriore incombenza. Evidentemente però l'avvocato degli italiani aveva già pronta la pubblicità ministeriale per incitare gli italiani al gioco, a tentare la fortuna. Permettetemi, signori: questa mi sembra davvero una vergogna. È dall'inizio della crisi che noi chiediamo a gran voce un anno bianco fiscale e solo ora la maggioranza sembra ascoltarci. Cito le parole pronunciate ieri dal capo politico del MoVimento 5 Stelle: «È una misura fondamentale a cui stiamo lavorando anche grazie a una seria collaborazione istituzionale con le opposizioni». Colleghi, per carità, va tutto bene, ma ormai è tardi: dovevate darci retta magari qualche mese fa. Non ci vuole Non ci vuole tanto a capire che, prima di elargire le mancette e l'elemosina agli italiani, bisogna *in primis* non farli pagare; è una misura di buon senso.

mi dispiace contraddire il collega Presutto, ma collaborazione vuol dire non utilizzare logiche distributive dei fondi, a mio parere assurde. Se noi pensiamo che, su 18 miliardi impegnati, ai parlamentari si sono lasciati da gestire 601 milioni,

il Governo ci ha trattato come se ci avesse dato un lascito ridicolo, inesistente. Questa dovrebbe rappresentare la nostra attività di legislatori, di eletti, e invece, veniamo mortificati da provvedimenti governativi quasi per niente modificabili dal Parlamento. al netto del nostro giudizio negativo sul provvedimento in sé, è ancora una volta quello che avevo fatto qualche mese fa in quest'Aula. Ascoltateci, ascoltate le nostre proposte perché l'Italia ha bisogno di interventi seri

dalla discussione in Aula è emerso che molteplici sono le criticità del decreto-legge in esame, a partire dai codici Ateco, dalla loro applicazione, dalla proroga delle scadenze fiscali così come è stata declinata, dal fatto che temi importanti come quello della giustizia siamo entrati in un provvedimento sui ristori per le attività economiche. Quattro decreti-legge sono stati emanati, uno dopo l'altro, non per la complessità del momento che stiamo vivendo, ma per il modo tardivo di operare di questo Esecutivo. Si è parlato di scuola, ma non si può dire che l'eventuale riapertura delle scuole a gennaio - se riapriranno - sarà un successo, perché il vero successo sarebbe stato continuare con la didattica in presenza sin dall'inizio, così come è avvenuto in altri Paesi europei. Il fatto poi che lo sgravio dei costi fissi delle bollette elettriche sia stata una misura già presentata in un precedente provvedimento dal Governo e dalla maggioranza significa che le misure adottate da questo Esecutivo non sono sempre distanti dalla sensibilità delle opposizioni. Il problema è che i provvedimenti sono sempre adottati a *spot,* con risorse limitate, senza continuità e senza una progettualità su cui noi invece riteniamo sia necessario puntare. Alcune proposte del centrodestra hanno riguardato temi corrispondenti a quelli della maggioranza, come dimostra una serie di emendamenti che sono stati approvati: ad esempio in materia di attenzione alle esigenze alle RSA, di agevolazioni alle assunzioni giovanili, di considerazione per l'editoria. Noi dell'opposizione abbiamo ritenuto doveroso puntare su tre aree di intervento per concentrare l'azione in maniera efficace. Ci auguriamo ora che tali interventi trovino la necessaria continuità nei prossimi provvedimenti. Noi ci mettiamo a disposizione del Paese con le nostre proposte, non senza lo spirito critico necessario nel merito.

ha sollecitato le autorità ad agire urgentemente, perché in molti Paesi ci si trova sull'orlo di una crisi di solvibilità, più di quanto non sembri, specialmente per le piccole e medie imprese, considerando che i programmi di sostegno sono in scadenza e che le massicce iniezioni di liquidità hanno contribuito a schermare la situazione. Tutte le nostre azioni sono ispirate a quest'obiettivo. Bisogna investire per far girare l'economia e far crescere il PIL con incentivi e riforme che favoriscano il mantenimento e la creazione di veri posti di lavoro. intervento ringraziando i colleghi relatori, il Governo, i Presidenti di Commissione e tutti i commissari per il lavoro che è stato svolto nelle scorse giornate

l'importanza che anche per il Governo hanno avuto il dibattito e il lavoro svolto in Senato sugli importanti provvedimenti in esame. Ci sono due aspetti che credo sia necessario sottolineare: qualunque sia la valutazione che viene data - e abbiamo avuto valutazioni difformi rispetto ai provvedimenti originari - è indubbio che l'intervento e il lavoro fatto in Senato ne abbiano aumentato sia l'efficacia che la portata, con un contributo rilevante che è venuto - va riconosciuto come dato aggettivo - sia dalla maggioranza che dalla minoranza. Questo è un aspetto che reputo positivo che va assolutamente sottolineato.

e - ahimè - del mondo, sarà necessario dare continuità ed essere vicini all'economia e alla società in ogni momento, cercando di affinare, completare e migliorare gli interventi, che pure dal punto di vista del Governo pensiamo siano stati già validamente messi in atto. Quindi, ci sono aspetti positivi anche nel dibattito, nelle critiche e nei limiti evidenziati e nelle tante proposte - vorrei sottolinearlo sono largamente contenute negli emendamenti, che non è stato neppure possibile esaminare perché i tempi sono stati stretti, e soprattutto negli ordini del giorno che li hanno recepiti e che devono essere valutati e considerati, perché sono ricchi di spunti. Penso che potrà essere messo a frutto anche nel proseguimento dei lavori parlamentari. Vorrei in particolare ringraziare, anche a nome del sottosegretario Castaldi

i relatori, che molto pazientemente ci hanno accompagnato passo per passo, e ovviamente - dico «ovviamente», ma non sempre li ricordiamo con la dovuta attenzione tutti i dipendenti degli uffici a cui abbiamo chiesto sforzi notevoli, sia festivi che notturni, cosa che non è proprio sempre da dare per scontata. Con questi ringraziamenti e con questo auspicio chiudo il mio intervento.

Su disposizione del Presidente, sospendo la seduta fino alle ore 16,30. *(La seduta, sospesa

Vi ringrazio. Onorevoli colleghi, la Presidenza ha esaminato gli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione del decreto-legge cosiddetto ristori

alla luce dei precedenti relativi ai provvedimenti d'urgenza, nonché in considerazione delle osservazioni e dei richiami del Presidente della Repubblica, contenuti da ultimo nella lettera dell'11 settembre 2020. In tale occasione, si è richiamata la sentenza n. 247 del 2019, nella quale la Corte costituzionale ha precisato che la legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge ed è caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario. Essa non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto. A pena di essere utilizzate per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso. Questa è parte della sentenza della Corte costituzionale. Nel caso di specie, non si tratta di un unico provvedimento a contenuto plurimo, ma di ben quattro provvedimenti a contenuto plurimo succedutisi nel tempo, tre dei quali confluiscono, attraverso emendamenti governativi, nel decreto-legge originario. Conseguentemente, nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite bilancio e finanze, si è reso necessario emendare i tre decreti successivi, divenuti a loro volta emendamenti al testo principale, attraverso lo strumento dei subemendamenti e di subemendamenti, per così dire, derivati. Solo ed esclusivamente per tale ragione sono stati ammessi subemendamenti aventi natura di veri e propri emendamenti aggiuntivi. Siffatta peculiarità non può tuttavia rappresentare un precedente di carattere generale, applicabile indistintamente per tutti i provvedimenti all'esame dell'Assemblea. Ciò per dire che questa è stata una misura eccezionale, per la difficoltà di lettura che tutti abbiamo avuto di questi provvedimenti. Pertanto la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, in quanto estranei all'oggetto del decreto-legge, gli emendamenti di cui all'elenco distribuito.

Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3*-ter,* del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento che recepisce le modifiche proposte dalle Commissioni in sede referente, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

rilevare, rispetto a quello che è stato inserito dal Governo nel maxiemendamento, quelle che ritengo essere le improponibilità e le stavo per pronunciare.

siano identiche rispetto alle improponibilità che lei ha dichiarato. È evidente che la fiducia il Governo la metterà non sul testo che è stato depositato, ma su quello che verrà sollecitato in senso modificativo da parte della Presidenza, e quindi porrà la fiducia su quel testo e non su quello che è stato depositato. Come ben sa, di solito il Governo presenta un testo che riproduce tutti tutti gli emendamenti che sono stati approvati in Commissione. Rispetto a questo testo, quello che ho distribuito è per completezza, nel senso di dire quello che fa la Commissione. Il giudizio del Presidente è inappellabile, come sa meglio di me. Cosa diversa è il precipitato di quello che è stato stato deciso dalla Commissione e che è entrato in un maxiemendamento, che ho esaminato. Alla luce delle improponibilità che ho posto nel testo fatto distribuire, vado a leggere quello che ritengo improponibile e lo sto facendo ora. Alla luce dell'intervento del Ministro, la Presidenza valuta l'emendamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-*ter* del Regolamento, salvo nelle parti che riproducono gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite dichiarati improponibili dalla Presidenza. Li

27.0.7, 27.0.9, 33.0.25 (testo 4), 1.1000/508,

mi dispiace di averla interrotta e le chiedo scusa. Le chiedo, come forma di cortesia nei confronti dei relatori, se per favore può leggere secondo l'ordine del fascicolo che ci è stato consegnato,

dato la parola. Capisco l'eccezionalità degli eventi e anche del processo normativo, inclusa la difficoltà di far confluire la bellezza di quattro decreti-legge all'interno di un unico provvedimento e quindi il meccanismo dei subemendamenti, così diffuso e complicato. Del resto, l'Italia vive un passaggio molto difficile per l'emergenza sanitaria e altrettanto per quella economica. Tuttavia, signor Presidente, mi sento obbligato a farle presente un tema soprattutto in prospettiva: personalmente, come tutto il mio Gruppo, ma credo forse tutta l'Assemblea, vivo con grande difficoltà un certo tipo di processo normativo, perché le forze politiche, con i loro Gruppi parlamentari, membri delle Commissioni alle quali lei ha assegnato i provvedimenti, discutono e si confrontano. La discussione e il confronto, signor Presidente, sono stati particolarmente delicati delicati e hanno visto un atteggiamento da parte delle opposizioni che mi permetto di definire costruttivo: nei loro confronti va il mio ringraziamento per averci permesso oggi di arrivare in Aula. C'è una fase nella quale la discussione diventa difficile e scopriamo, solo alla fine del processo, che una parte di quelle decisioni

un lavoro, costruirlo e perseguirlo fino in fondo, per poi arrivare alla considerazione finale che tutto il lavoro a monte, spesso su diversi temi, è stato

Senatore Marcucci, prendo atto. La sua difficoltà è anche stata la mia, perché perché su questo testo abbiamo lavorato. Certamente, ci siamo trovati di fronte all'esame di 4.000 emendamenti. emendamenti. Non è stato tanto un problema di quantità, quanto di qualità. Come sa, valuto non il merito, ma l'estraneità di materia e su questo provvedimento è stato davvero difficile: per questo ho detto che è stata un'eccezione che non costituisce un precedente, perché spero che non ci sia più questo modo di lavorare. Signor Presidente, intervengo perché il capogruppo Marcucci ha fatto riferimento a un disagio di tutti i Gruppi parlamentari. Vorrei chiarire che nelle Commissioni 5a e 6a riunite, come Gruppo,

abbiamo anche deciso di non partecipare alla votazione di alcuni emendamenti, perché, al di là del merito, ritenevamo che fossero estranei per materia e che fossero altre le sedi in cui legittimamente potevano essere discussi e approvati,

e la necessità di dare risposta a categorie produttive di lavoratori danneggiate durante i periodi di chiusura delle Regioni e delle attività che sono si sono succeduti.

alla fine abbiamo bisogno di una sola cosa: disporre del tempo adeguato, che è necessario per visionare non tutto l'elenco iniziale, che giustamente ha riportato, ma quello ristretto delle improponibilità legate al secondo elenco di emendamenti, che vanno effettivamente a incidere sul testo sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Speriamo che la Commissione competente abbia un tempo adeguato e sufficiente per approfondire le modifiche, perché

Presidente, ho ascoltato con attenzione quello che ha detto e condivido alcune cose, con molta sincerità.

siamo arrivati a questo punto. Presidente, onorevoli senatori, come Governo accettiamo le indicazioni della Presidenza sulle improponibilità proposte, nel contributo del testo per le improponibilità indicate all'interno del maxiemendamento; quindi, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1994, nel testo ritenuto proponibile dalla Presidenza, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

un evento senza precedenti nella storia del Senato decreti-legge che si succedono sotto forma di emendamenti, subemendamenti e subemendamenti al subemendamento. L'attività dei Gruppi, ma anche degli Uffici e della stessa Presidente è stata resa complicatissima da chi al Governo ha scelto questa strada, pericolosa e confusa. Peraltro voglio ricordare che circa venti giorni fa,

un tema così delicato, dovendo avere a che fare con emendamenti che andavano a toccare il testo originario, mentre venivano toccati e modificati a loro volta da emendamenti successivi, che erano i decreti ristori al Governo di legiferare con più ordine, magari prevedendo due decreti accoppiati e poi un altro, anch'esso accoppiato, ma non siamo stati ascoltati. quindi è davvero incomprensibile che, soprattutto dalle parti della maggioranza, ci si lamenti della confusione in cui siamo costretti a votare questo maxiemendamento.

La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo, così come stralciato.

trattava di testo 2. Per il resto va tutto bene. Nell'elenco di carattere generale va stralciato dall'improponibilità l'emendamento 1.0.52.

Per la discussione sulla fiducia è stata ripartita un'ora e venti minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno le dichiarazioni di voto finale e la chiama. È stato inoltre stabilito che la seduta di domani avrà inizio alle ore 10,30. La Presidenza precisa che l'elenco in distribuzione sulle improponibilità va corretto, nel senso che il riferimento dell'emendamento 23.0.8 va inteso come 23.0.8 (testo 2), identico all'emendamento 23.42. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia. È iscritta a parlare la senatrice Rivolta. Ne ha facoltà.

anomalo. Voglio ricordare come sia la prima volta che a un decreto ne seguano altri tre, che ne diventano poi parte attraverso emendamenti. Quindi si può parlare di un decreto-legge ristori quattro in uno. La rituale verifica delle inammissibilità per l'Aula ha portato poi allo stralcio di ben venti emendamenti, di cui undici con testi 2, 3 e addirittura 4. Ma voglio sottolineare come ci sia stato un altro strappo al Regolamento e alle prassi da parte di questo Governo con la sua maggioranza, sua maggioranza, con altri colpi alla Costituzione. Insomma, già abbiamo dovuto vedere il quasi sistematico superamento del bicameralismo perfetto, ormai abolito, e soprattutto sempre e regolarmente la fiducia posta sui vari decreti-legge. Ricordo - mi piace ricordarlo tutte le volte che dovrebbe esserci un equilibrio sancito dalla Costituzione, che parla appunto di un equilibrio che deve essere sempre mantenuto tra i cinque organi costituzionali. Ripassiamo insieme: Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo, Corte costituzionale e magistratura. Mi sembra che di strappi a questo equilibrio se ne facciano molti e si continui soprattutto a farli. Ed ogni volta

Sono tutti precedenti pericolosi. Molti colleghi della maggioranza hanno contestato la modalità della nostra condotta, definita ostruzionistica.

Ma cosa pretende la maggioranza? *(Applausi)*. Non dovremmo presentare emendamenti e non usare i tempi previsti dal Regolamento? Oppure anche cantare «Viva Conte presidente, noi diciam che grande mente»? Volete che cantiamo le canzoncine? Se una parte della maggioranza ha presentato 1.109 emendamenti, vuol dire che non è soddisfatta

Soprattutto volevo dire che i nostri emendamenti sono volti a migliorare il testo e a dare ristoro a molte realtà completamente dimenticate. Voglio fare un esempio che ritengo molto significativo. In un'epoca così *green*, in cui tutti i giorni si parla di svolta *green* e si dice che bisogna cambiare modalità di vita, di produzione, di attenzione e cultura, noi eravamo tutti convinti che bisognasse salvare il mondo dell'apicoltura.

è stato ignorato. Quindi, anche il vostro essere *green* è fasullo, perché poi, alla prova dei fatti, come questo sono state ignorate tantissime categorie e tantissimi settori dietro i quali ci sono persone vere e famiglie vere. vere. Che fine faranno? L'Istat ha riportato, qualche giorno fa, un dato sconvolgente: su 73.000 aziende in crisi 17.000 non riapriranno. Quante persone, quante famiglie, quante storie, quanta disperazione dietro tutto questo. Però non c'era abbastanza capienza. Si può capire, ma

ai molti colleghi che hanno contestato anche questa cosa - abbiamo certamente contratto un debito. Prima c'è la sopravvivenza ma, se non ci sarà un sostegno per lo sviluppo, non andremo molto lontano.

in una fase di sviluppo e di ripresa. Tale aspetto è veramente di una gravità unica. È per quello che parliamo di lungimiranza.

Noi continuiamo a dirlo, continuiamo a urlarlo. Abbiamo cercato di lavorare al meglio, anche con comportamenti responsabili. Abbiamo avanzato

perché anche voi potevate avere tantissime proposte serie da fare, ma al Governo, di noi, ma anche di voi, sinceramente non importa tanto. *(Applausi)*. Io penso che, al di là di tutto, sia una cosa veramente grave e mi spiace che da parte della maggioranza, tutto sommato, non si dica più di tanto su questo fatto. Stanno cambiando questo Paese non fa niente, ma stiamo parlando della nostra istituzione, della nostra Costituzione, ma è sacra a giorni alterni?

la cifra che si pensava di utilizzare per il *quinquies* nella legge di bilancio, ma c'è stato risposto che probabilmente non avrebbe resistito agli attacchi feroci e famelici di alcune parti.

a fare la nostra parte con serietà. Spero che capiate che è faticoso anche fare opposizione e sinceramente sentirci dire, come addirittura dobbiamo fare opposizione mi sembra una cosa fuori dal mondo. *(Applausi)*. Noi continuiamo a fare quello che riteniamo giusto, in maniera seria e sempre in rappresentanza delle aziende, delle famiglie e dei cittadini, che meritano attenzione anche se sono piccoli e in settori che sembrano insignificanti.

che è un atto generale sull'operato del Governo, appunto prescinde dal merito del provvedimento su cui abbiamo cercato, e soltanto in parte ottenuto, di realizzare un nostro intervento migliorativo, come tutte le forze del centrodestra e dell'opposizione. Si tratta della fiducia e quindi in questo caso non possiamo che esprimere con forza il nostro no. Abbiamo detto no in altre occasioni a questo Governo che esautora il Parlamento e al suo Presidente che esautora il Governo. no a questa maggioranza che, in piena emergenza Covid, si divide - sembra - su questioni di Ministeri e di poltrone (togliti tu che mi ci metto io) ed è qui la prima anomalia che voglio evidenziare a questa

con una verifica di Governo in atto. C'è una verifica sul vostro Governo e nel contempo chiedete al Parlamento la fiducia. È una questione di poltrone? Non è una questione di poltrone, vi credo, perché è peggio: è una questione di cassa, di denaro e di *intelligence*, di Servizi. Lo ha detto uno tra voi, un ex Presidente del Consiglio, quando ha parlato dei Servizi, della delega, dell'Istituto cibernetico del nostro Paese. Ed è un problema di cassa e io direi di banca o di banche. Noi sappiamo bene che voi vi accapigliate sul tesoretto. Io qui in Aula, l'altro giorno, parlando del Presidente del Consiglio, l'ho definito come Gollum nella saga «Il signore degli anelli».

e voi, tutti intorno a questo presunto tesoretto, dite che no, è anche vostro. Non basta la cabina di regia, non è soltanto suo questo tesoretto, ma è anche vostro. Parliamo del *recovery fund*,

che usavano l'immagine dell'apriscatole che apriva le scatole di tonno: ciò che state facendo è la tonnara della democrazia,

Chi li mette questi soldi e perché di soldi, di denaro e di banche si tratta? Un sovranista - che forse tale non è - come Federico Fubini,

Gaia, per lo spazio e l'avio, per il 5G, per il sistema di pagamento. Cosa vogliono questi francesi? Ci dice anche che tra Parigi e L'Aia, tra Parigi e l'Olanda, con la supervisione tedesca, c'è uno strano aggirarsi in Europa. Cosa dice Federico Fubini, e non un sovranista? Dice che si stanno cercando di chiudere tutte le strade aperte dal Governo italiano negli ultimi anni per salvare l'operatività delle banche. banche. Con il MES, l'unione bancaria e con tanti altri, stanno chiudendo tutte le strade di salvataggio delle banche. Non lo dico io, lo dice il «Corriere della sera» e Federico Fubini. Ciò perché in in Italia, qualcuno sospetta, che a Parigi si stia cercando di chiudere la scappatoia per i salvataggi in modo da gettare le basi di una nuova stagione di acquisizione di banche italiane in difficoltà da parte di Paribas,

Perché mentre noi abbiamo proposto e ottenuto - e ringraziamo la Presidenza per aver salvaguardato quell'emendamento - che la *golden power*, che noi stessi chiedemmo al Governo a marzo e poi il Governo ci concesse ad aprile

per altri sei mesi. Avete quindi gli strumenti per tutelare quello che non io, ma il «Corriere della sera» denuncia si stia preparando come il sacco delle banche e del risparmio italiano.

sta accadendo che mentre noi discutiamo e vi forniamo lo strumento per proteggere l'Italia, voi, alla Camera dei deputati, nella manovra di bilancio avete inserito una norma, peraltro senza definire lo stanziamento, che facilita le aggregazioni le fusioni tra le banche per sopperire a quello che sta per capitare, a quello che anche Draghi ha denunciato oggi, una nuova ondata anche di insolvenze, di crediti deteriorati che metterà a rischio il sistema del nostro Paese.

tra primo salvataggio, ricapitalizzazione, ristori agli azionisti e poi l'acquisto da parte di AMCO di 8 miliardi di crediti deteriorati.

la parte internazionale di Unicredit per cederla a francesi e tedeschi in cambio della fusione con Banca Monte dei Paschi di Siena, con la vostra banca. Voi avete stanziato 3 miliardi su quella norma per favorire la fusione e poi altri 2,5 miliardi grazie al cosiddetto decreto agosto

questo si sta facendo la verifica di Governo: se banca Monte dei Paschi di Siena resta in mano ai 5 Stelle, che se ne sono impadroniti pochi mesi fa e che vuole fare una banca pubblica insieme a Carige e alla Banca popolare di Bari, o se la banca del PD torna al PD che si è preso Unicredit con Padoan.

approvato farebbe saltare il Monte Paschi di Siena (o meglio rimarrebbe pubblica), ma consentirebbe a una sola banca, a Crédit Agricole e ai francesi, di fare l'operazione sul Credito Valtellinese con i soldi pubblici. Vale 450 milioni, sarebbero gli unici a farlo. Di conseguenza il sistema italiano sarebbe scoperto.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, io continuo a pensare (e questa è la posizione del Partito Democratico) che il confronto tra la maggioranza e l'opposizione nelle Commissioni riunite sia stato utile e costruttivo, lo ribadisco. In molti In molti casi, lo voglio ripetere ai colleghi intervenuti poc'anzi, a cominciare dal senatore Urso, il voto di fiducia viene dopo aver votato il mandato al relatore, dopo aver approvato in Commissione, in un percorso ordinato, diversi emendamenti, frutto di una collaborazione costruttiva tra maggioranza e opposizione. I relatori hanno svolto un compito complesso e difficile con equilibrio; il Governo ha contribuito a favorire un dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione. Questi sono i fatti. Non serve alzare il tono della voce, anzi in molti casi gli urli nascondono l'assenza di proposte e di contenuti propositivi utili a quest'Assemblea e soprattutto al Paese nella gestione di una fase così difficile come quella della pandemia che stiamo attraversando. Questi sono i fatti che confermano che è utile un confronto tra maggioranza e opposizione e che il confronto tra maggioranza e opposizione si è sviluppato nella pienezza del suo funzionamento. La questione di fiducia viene posta dopo questi voti e dopo questo percorso ordinato e costruttivo. Se molti temi, a cominciare dall'esenzione dalla COSAP e dalla TOSAP, dal tema dei dottorandi, dal sostegno alle residenze sanitarie, così importanti e così in difficoltà in questa gestione pandemica, così come l'intervento per favorire la riduzione dei canoni sugli affitti, insieme alle tante altre proposte che voglio per chiarezza sottolineare, dalla riduzione del peso delle bollette energetiche fino agli interventi utili nei confronti del sistema delle Regioni e del sistema dei trasporti in questo Paese, sono tutti temi che hanno visto un largo consenso all'interno della Commissione e sono il frutto, e dunque l'arricchimento, di una prospettiva legislativa utile complessa. Siamo infatti in presenza di quattro decreti convertiti in uno, che credo debba essere un patrimonio non così poco rilevante, come in molti casi è stato rappresentato in questa sede. Lo dico perché ho grande rispetto per le prerogative dell'opposizione, però il contesto che ho raccontato non è compatibile con le tante affermazioni che ho ascoltato in quest'Aula dai colleghi del centrodestra: attribuire cioè al Governo la responsabilità della seconda ondata pandemica e chiederne ogni tanto (anzi oserei quasi dire spesso) le dimissioni è, credo, il volto peggiore di un'opposizione irresponsabile che non solo mostra la sua contrarietà nei confronti del Governo, ma ostacola il bene comune, cioè le famiglie e le imprese italiane. Questo esercizio credo che rappresenti il volto peggiore delle prerogative così importanti che invece le opposizioni potrebbero rappresentare, perché dentro una pandemia è un'anomalia italiana la richiesta di dimissioni, una critica senza contenuti e in molti casi una critica che trova la non verità delle proposte rispetto agli atti acquisiti da parte del Governo. È un'anomalia italiana. In ogni angolo del Paese questa pandemia ha un volto duro e difficile. La seconda ondata pandemica ha attraversato l'Italia come tutti gli altri Paesi europei e se guardiamo al tasso di mortalità, che oggi anche l'Istat ci mette di fronte, siamo di fronte ad un tasso di mortalità che supera quello di una guerra. E se siamo di fronte ad un percorso (non voglio fare anticipazioni) che probabilmente dovrà vederci protagonisti della gestione di una terza ondata pandemica, che speriamo di evitare e di scongiurare, questo quadro richiede responsabilità. Dovete togliere di mezzo urli e insulti inutili e avanzare proposte costruttive nell'interesse del Paese. *(Applausi)*. Questo per quello che ci riguarda è la sfida che abbiamo di fronte. Siamo perfettamente consapevoli che stiamo parlando di oltre 20 miliardi di euro, 8 miliardi di nuovo indebitamento e 12 miliardi di riutilizzo di risorse che erano già inserite all'interno dei saldi di finanza pubblica. Sono risorse utili perché i codici Ateco hanno sì dei limiti, ma hanno consentito all'Agenzia delle entrate, in tempi celeri, di garantire ristori che in qualche modo fatto un'opera di prevenzione di fronte a conflitti sociali possibili, perché quando si introducono nuove limitazioni il rischio di un conflitto sociale cresce. Allora, colleghi, lo dico con grande chiarezza: dobbiamo toglierci dalla testa l'idea che dentro un'emergenza si possano affrontare temi strutturali irrisolti. Io credo che il Governo abbia prodotto numerosi decreti ristori e ne elaborerà altri nelle prossime settimane anche per il mese di gennaio; non è il frutto di una mancata programmazione, ma è il frutto dell'esigenza di leggere le dinamiche economiche per dare risposte adeguate a dinamiche economiche complesse e inedite che dovremo affrontare. Potrei fare un esempio banale: dobbiamo mettere anche in cantina la dietrologia e il dibattito del passato. Ho sentito parlare da rappresentanti del centrodestra e dell'opposizione di un anno fiscale bianco, di meno tasse per tutti, di sospendere la pressione fiscale e il gettito delle entrate del nostro Paese. Guardate che non c'è lo spazio; è un qualcosa di iniquo e ingiusto. Noi dovremo sempre di più lavorare sull'equità e sulla riduzione delle disuguaglianze perché questa crisi pandemica ci mette di fronte nuove disuguaglianze e non colpisce tutta l'economia allo stesso modo. Sarà necessaria, d'ora in avanti, se vogliamo accompagnare la gestione dell'emergenza, una visione per l'uscita dell'emergenza. Da qui nasce l'esigenza di un quinto decreto ristori a gennaio, dove dovremo fare con grande concretezza un'analisi sulle filiere che sostituisca quella dei codici Ateco, che possono servire in una prima emergenza, ma non sono lo strumento e la risposta compatibile con l'esigenza di individuare le filiere più colpite. Una cosa è la manifattura che esporta nel mondo le macchine automatiche e un'altra sono il turismo e i servizi, che hanno bisogno di coprire l'intera filiera. I nuovi provvedimenti economici dovranno individuare le filiere al posto dei codici Ateco. Chiedo al Governo di tenere conto del lavoro svolto nelle Commissioni. Ci sono tanti emendamenti approvati che vanno verso la trasformazione dei codici Ateco in filiere; vanno nella direzione di esaminare per alcune filiere non il mese su mese, ma il trimestre su trimestre; vanno nel senso di individuare le priorità per salvare le imprese, che non sono tutte uguali. Ciò riguarda anche il tema della riduzione della pressione fiscale. Forse vi siete dimenticati che il decreto

Non c'è lo spazio per la demagogia dell'Ottocento e del Novecento, che continua a dividere maggioranza e opposizione su *slogan* inadeguati nella lettura della crisi pandemica perché le disuguaglianze aumenteranno

da chi, magari, non ha subito gli effetti della crisi o dentro la crisi è stato in grado di reggere la sfida. Per poter uscire dall'emergenza, l'esigenza che abbiamo oggi è di cominciare ad accompagnare nel prossimo decreto delle misure per uscire dall'emergenza. Ciò significa che probabilmente diverse misure economiche dovranno essere equiparate alla trasformazione in chiave energetica dell'economia; diverse misure economiche dovranno essere direttamente collegate allo sviluppo dell'Italia digitale.

Ci accorgeremo sempre di più che la transizione ecologica dell'energia e dell'economia e la transizione digitale richiedono un percorso di formazione universale. Noi avremo bisogno degli ammortizzatori selettivi, di un reddito di formazione e di aiutare le persone deboli e fragili che restano indietro con il reddito di cittadinanza, ma avremo bisogno di un reddito di formazione per accompagnare le dinamiche del lavoro verso il futuro. Le politiche attive richiedono una riforma. Allora, dico con grande chiarezza che questa deve essere l'asticella della sfida. sfida. Con il decreto ristori bisogna cominciare a traguardare un'uscita dell'Italia dalla crisi. Questa non è mancanza di programmazione, ma capacità di lettura delle ricadute pandemiche che dobbiamo affrontare

l'altro come scatole cinesi - in cui davvero non si capisce cosa contenga l'una, ma si capisce quanto sia facile che sia in contraddizione con quella che la precede e con quella che la segue - ciò che, ripeto, mi ha veramente sorpreso sono state tre testimonianze La prima è stata quella del Governo, concretamente nella persona del sottosegretario Guerra, la quale ha voluto giustamente rivendicare la qualità del lavoro fatto anche dal Parlamento, dal Senato, riconoscendo limiti ed errori dei provvedimenti così come erano usciti dalle mani stesse del Governo. È stato un tono molto pacato il suo, direi anche molto umile, ma chiaramente decisamente orientato a sottolineare i limiti strutturali dei documenti che ci sono stati consegnati e la mancata attività di revisione degli stessi documenti, l'uno accanto all'altro, che il Governo per primo avrebbe dovuto fare.

È mancato questo lavoro proprio da parte del Governo; non lo dico io evidentemente, ma l'ha detto il Sottosegretario ed è agli atti. La seconda testimonianza che vorrei sottolineare - anch'essa mi ha colpito molto - si riferisce a quando il collega senatore Faraone, capogruppo di Italia Viva, si è alzato in piedi chiedendo dieci minuti, un quarto d'ora, ovvero il tempo necessario a cercare di capire che diamine avremmo votato. Ora, evidentemente non è un Capogruppo dell'opposizione; è un Capogruppo della maggioranza, ma a questo punto tutti potremmo immaginare che - si sa - quelli di Italia Viva ogni giorno che passa ce ne hanno una per negoziare la loro posizione e il loro ruolo all'interno del Governo e provare a contare di più. Insomma, avremmo potuto pensare che il buon Faraone prendeva quella posizione per evidenziare e denunciare il fatto che

legge, colui che in qualche modo garantisce non solo il prodotto finale, ma anche le procedure alla luce delle premesse,

non so su che cosa ci stanno chiedendo la fiducia. È evidente, colleghi, che chiedere la fiducia su un oggetto che i principali responsabili non sanno cosa contenga è un atto di grande arroganza. È un atto che sta a significare: non importa che cosa ti dico, tu la fiducia me la dai perché io governo, perché tu sei tu e quindi ti devi fidare. È molto difficile, come si dice, affidarsi e fidarsi di qualcuno che non sa che cosa chiede, di qualcuno che ha perso di vista il processo, perché quando il relatore dice di voler leggere cosa c'è scritto vuol dire che egli stesso ha perso di vista il filo di Arianna, che avrebbe dovuto attraversare l'intero procedimento. Signori, tra pochi minuti ci chiederete la fiducia *nominatim*, sappiamo già come finirà: l'opposizione dirà chiaramente no, stando nella verità dei fatti; la maggioranza dirà di sì per qualche misteriosa alchimia, perché lei stessa non sa come stiano davvero i fatti. Maggioranza e opposizione saranno però condannate a un gioco delle parti in cui l'opposizione fungerà da parte che non collabora e non collabora perché non può dare un consenso a condizioni di così grave disinformazione. Il consenso, lo impariamo tutti, è un consenso informato: senza correttezza dell'informazione il consenso è veramente un abuso di fiducia, una mancanza radicale di quella virtù straordinaria per l'arte del buon governo che è la prudenza.

Detto questo, è evidente che, in questa sequenza di decreti ristori, guardiamo con orrore anche al quinto decreto, l'ennesima provocazione.

debba pensare un oggi per l'ora, per l'*hic et nunc*, per questo momento per cui, cambiando le condizioni al contorno, deve cambiare anche la norma data? Questa improvvisazione è veramente lesiva della dignità del Senato. Ciò che è grave, innanzitutto, è il fatto che il Governo ignori sempre, totalmente e sistematicamente le proposte dell'opposizione, come se l'opposizione fosse fatta di persone che vogliono soltanto creare pregiudizio

condizionata e capace di guardare anche oltre lo stretto immediato risultato del consenso popolare in una dialettica che si snoda alla ricerca di un consenso troppo

il nostro vaccino sarebbe arrivato per primo - peccato che forse arriverà per quarto, quinto o penultimo - o che magari i contagi diminuiscono e che, se per caso aumentano, è sempre colpa della gente che sta per strada, o senza mascherina o semplicemente in una relazione troppo stretta. Non ci viene però mai detto perché siamo il Paese in cui in Europa si muore di più:

un tasso altissimo di persone che muoiono, né ci dicono perché Draghi, presidente fino a poco fa della BCE, oggi esce su tutti i giornali per dichiarare che la situazione economica alla quale andiamo incontro sarà di gran lunga più grave di quanto viene detto. C'è dunque un inganno di sistema, che io credo sia frutto anche dell'ignoranza di sistema, dell'incapacità di governare, di prevedere e di assumere le responsabilità per il futuro. Come si può chiedere la fiducia?

avvincente la sua lavorazione, come ben sa il pezzo di Governo qui presente, un pezzo a noi caro e certamente rilevante per il suo incarico, anche se magari qualche Ministro di area economica ci avrebbe confortato con la sua presenza, ma noi tenteremo lo stesso di parlare di numeri e del tema.

l'ultimo decreto era un emendamento del primo, infatti, si è dovuti partire dall'ultimo per risalire al primo. Tutte cose bellissime, che hanno costituito oggetto di avvincenti lezioni per i

Solo sul tema della fiducia mi sento di aprire e chiudere immediatamente la discussione. Alla fine, infatti, noi abbiamo passato tanto tempo, grazie anche al lavoro dei relatori grazie all'eccellente lavoro dei Presidenti di Commissione (che qui non vedo, perché uno adesso è impegnato), a lavorare costruttivamente, con queste difficoltà tecniche che hanno reso molto avvincente questo decreto-legge. Siamo passati da alcune migliaia di emendamenti a poche decine di emendamenti, su cui ci siamo messi d'accordo. Quindi, pensavamo di poter andare ad una lavorazione ordinaria del provvedimento in Aula ed a una conversione con delle votazioni: quell'atto che, a quanto pare, a questo Governo, o a pezzi rilevanti di esso, risulta abbastanza allergico e antipatico. Invece, improvvisamente, a sorpresa di fiducia. Allora, la riflessione che uno fa è questa: se si deve mettere la fiducia su un decreto la cui conversione comporta 40 votazioni, questo cosa significa? che i primi a non fidarvi di voi stessi siete voi. Partendo dal presupposto che voi vi conosciate meglio di quanto vi conosciamo noi, perché, allora, dovremmo darvi la fiducia, se voi stessi non vi fidate? *(Applausi)*. Non vi fidate al punto da blindare, con una fiducia, un provvedimento su cui, sostanzialmente, esisteva un accordo,

fuori. La discussione sulla fiducia, quindi, è presto chiusa. Non sta a me fare la dichiarazione di voto, ma la dichiarazione di voto è nelle cose. Visto, però, che qualcuno prima aveva voglia di contenuti, approfitto per dare qualche dato, così ragioniamo di che cosa stiamo parlando.

e dà, per quest'anno, un risultato del meno 9 per cento. Goldman Sachs è ancora più ottimista: ci dà un meno 8,7 per cento. In Germania tutte le previsioni danno un meno 5,8 oltre 3 punti più in basso della Germania in questa classifica. Ma che cosa succederà l'anno prossimo? Questo è interessante, perché Goldman Sachs, estremamente ottimista, nel 2021 ci dà al 6 Le previsioni di consenso ci danno al 5,5 per cento. Bankitalia, a luglio, ci dava al 4,8 per cento. Sempre Bankitalia, nelle previsioni di dicembre, dopo aver visto l'importante potenza di fuoco dispiegata da questo Governo, ci ripensa e ci dà al 3,5 per cento. A fine anno, con le informazioni sulle misure prese durante il 2020, rivede di meno 1,3 punti la crescita per il 2021. Ancora Banca d'Italia ci informa che ci vorranno tre anni per tornare al livello del PIL del 2019. Quando saremo tornati al livello del PIL del 2019, sarà il 2023; e nel 2023 saremo dov'eravamo nel 2019, cioè circa cinque punti sotto il reddito del 2007, che, nel frattempo, sarà diventato il reddito di sedici anni prima. Parliamo, allora, degli occupati. Sempre la Banca d'Italia dice che quest'anno andremo a meno 1,8. Quindi, l'anno prossimo ci sarà il rimbalzo? No, ci sarà il trascinamento a meno 1. Da quando si rimbalza? Dal 2022. Sì, ma per il 2022 serve la palla di vetro. Pare che si farà un 1,6 e poi un 1,2. Quindi, forse nel 2023 avremo un po' quasi gli stessi occupati del 2019. Tutto questo di fronte a una macchina dello Stato in cui l'unica cosa che funziona a pieno regime è il fisco. Non so se avete visto i titoli di «Italia oggi», che parlava di 31 milioni di atti: va bene, hanno un po' inflazionato il numero, mettendo

Rinviare le scadenze fiscali, senza voler prendere una decisione di qualsiasi tipo sulla loro gestione. A un certo punto, però, bisognerà tirare una linea e allora che succederà? Rinviare poi con le garanzie: la famosa potenza di fuoco non erano soldi che metteva lo Stato, ma che avrebbe dovuto mettere il sistema bancario (con un atto d'amore, che poi non è stato così travolgente) e rispetto al quale lo Stato metteva la garanzia. Sapete e sappiamo benissimo che molti imprenditori, piccoli, medi e grandi, non saranno in condizione di restituire Non si è voluto intervenire in modo diverso e si è voluto lasciare a chi verrà dopo l'onere di coprire le garanzie, quando verranno escusse. Rinviare con tutte le varie misure di credito di imposta, che sono un semplice differimento di gettito, che apre un altro buco insidioso, dai contorni non facilmente quantificabili, nel bilancio dello Stato. Rinviare, infine, anche col patrimonio destinato, perché alla fine bisogna vedere come sarà gestita questa misura. Stiamo cercando di studiare il regolamento, in Commissione finanze e tesoro,

i quali comunque, poverini, si sa che non potranno governare, perché il dottor signor De Benedetti ha detto in televisione che, quando arriveremo noi, l'Unione europea ci schianterà. Se non ci schianterà lei, colleghi, ci schianteranno i debiti che ci avete lasciato, ma siamo pronti ad affrontare con coraggio questo destino e anche a dire cosa avremo fatto e cosa è stato fatto in altri Paesi. Il risultato dell'Italia, infatti, non nasce, come questa sinistra insistentemente cerca di dimostrare, da un'inferiorità antropologica degli italiani, ma da errori fatti da questo Governo. Intanto vorrei ricordare il tema della pace fiscale. Dobbiamo pure porci il problema di cosa fare, quando non sarà più possibile rinviare e una proposta ce l'abbiamo: riaprire i termini della rottamazione-*ter*, intervenire con una definizione agevolata del contenzioso e fare uno stralcio delle mini-cartelle. *(Applausi)*. Sono tutte cose che allevierebbero di molto anche i costi di gestione

e uno da 130 miliardi di euro, e un vero fondo perduto, prima con il *Soforthilfe* e poi con l'*Überbrückungshilfe,* e alle aziende sono arrivati i soldi (prima 18 miliardi di euro) e il primo fondo perduto è più di tutti i pezzettini di fondo perduto che abbiamo visto arrivare da

La BCE avrebbe coperto e sta coprendo. Allora come volete giustificare questi ritardi? È subalternità rispetto a Bruxelles o paura che, avendo troppi soldi a disposizione, le contraddizioni interne della maggioranza esplodano nell'assalto alla diligenza? Ditecelo, però risolvete questo problema, perché il Paese non può più permettersi di aspettare.

Possiamo definirlo, in ordine di grado, il più importante dopo il decreto rilancio, che ha attutito gli effetti del primo duro *lockdown* della scorsa primavera. Lo considero il più importante in quanto a rapidità, efficienza e capacità di sostenere a tutti i livelli il tessuto sociale del nostro Paese. Ci siamo fatti trovare pronti, quando le condizioni dello stato pandemico si sono improvvisamente e nuovamente aggravate, perché tutte le ulteriori necessarie restrizioni, se non sorrette da un adeguato supporto, avrebbero potuto minare la tenuta di tante imprese in pericolo, già provate, che fin dall'inizio dell'estate sono ripartite, hanno investito per poter riaprire, hanno sostenuto l'offerta di posti di lavoro e poi purtroppo hanno dovuto abbassare di nuovo le serrande, a causa di questa perdurante pandemia. L'economia, nonostante il duro colpo, tiene e i risultati ottenuti che man mano tocchiamo sono il frutto di un intenso lavoro di studio e analisi del Governo e nostro (del Parlamento) sugli strumenti e sui dati socio-economici e finanziari che abbiamo a disposizione adesso. L'esperienza del primo *lockdown* di marzo ci ha mostrato infatti un dato inequivocabile: il miglior strumento per ristorare celermente le nostre imprese è stato l'accredito diretto sul conto. I dati in nostro possesso, relativi alla prima *tranche* di marzo, hanno permesso a chi aveva già usufruito del fondo perduto un accredito rapidissimo. Proprio perché la rapidità era l'elemento prioritario, noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo chiesto espressamente al Governo di assicurare rapidità e automatismo negli indennizzi alle imprese coinvolte in questa grave questa grave crisi pandemica. Il positivo lavoro dell'Agenzia delle entrate ha consentito di assicurare, nei primi dieci giorni, l'erogazione di un miliardo di euro a livello nazionale, per un totale di circa 200.000 aziende in crisi colpite dalla seconda ondata pandemica. I dati ci dicono anche che sono stati rispettati i vincoli per assicurare un maggior gettito alle Regioni inserite subito in zona rossa, rispetto alle altre. Anche su questo, l'obiettivo di arrivare a risultati concreti in poco tempo si è realizzato. Il decreto ristori è stato solo il punto di inizio, a cui sono seguiti altri provvedimenti. È stata la prima dimostrazione che lo Stato c'è e che ha saputo dare una risposta concreta in tempi brevissimi. Sottolineo ancora una volta l'importanza di quanto appena descritto, perché è importante evidenziare che, all'inizio della seconda ondata di infezione, la maggioranza ha risposto prontamente, intervenendo nuovamente e con la massima rapidità. Non appena sono scattate le nuove restrizioni, il 24 ottobre, nel giro di pochissime ore, è stato scritto ed emanato un decreto importantissimo per la tenuta del Paese. È per questo che in premessa ho sottolineato la massima importanza del decreto ristori sin dall'inizio della pandemia. Non intervenire presto avrebbe significato emergenza sociale diffusa, crisi totale del settore impresa e serio rischio di una depressione economica, anche decennale. Per scendere maggiormente nel dettaglio, parliamo di numeri. Ne parlo anch'io, ma i miei sono diversi. Alla data del 10 dicembre, sono stati completati i pagamenti di tutti i contributi automatici previsti dai quattro decreti ristori (quindi parliamo di cose già avvenute), per un importo complessivo che supera i 2,3 miliardi di euro. Gli accrediti sono stati effettuati da un minimo di quattro giorni a un massimo di quindici, rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti. A questi bonifici si aggiungono i 6,6 miliardi di euro erogati dall'Agenzia delle entrate, relativi al decreto rilancio. Sono partiti inoltre prima 28.000 contributi a fondo perduto per gli esercizi aperti al pubblico nei centri storici delle città italiane, più turistiche, che hanno fatto domanda sul sito dell'Agenzia. Dunque, in totale, al 7 dicembre 2020, i contributi a fondo perduto e i ristori erogati dall'Agenzia delle entrate ammontano a più di 9 miliardi di euro, mentre la platea dei beneficiari è rappresentata da 2,4 milioni di partite IVA. Di questo monte complessivo, 1,8 miliardi hanno raggiunto il settore della ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie); più di 2 miliardi di euro sono stati destinati al commercio al dettaglio (supermercati, *discount*, farmacie, edicole ed altri) e quello all'ingrosso; più di mezzo miliardo di euro al settore dell'edilizia. Il decreto-legge oggetto dell'odierna discussione, però, non è soltanto fondo perduto. Parliamo anche di sostegno allo spettacolo, al cinema, alle agenzie di viaggio, all'*export* e alle fiere. Parliamo di proroga della cassa integrazione, del blocco dei licenziamenti, della cancellazione della seconda rata IMU, dell'esonero e sospensione dei contributi, dell'incentivo allo *smart working* di altre due mensilità di reddito di emergenza, su cui tornerò. Parliamo anche di altre novità, apparentemente piccole, ma significative, come l'estensione del microcredito, la riduzione delle bollette energetiche, lo sconto dello Stato da applicare ai proprietari di abitazioni che ridurranno i canoni di locazione ai nostri cittadini che vivono in affitto. Abbiamo cercato di farlo con la dovuta attenzione, proponendo di restituire ai proprietari degli immobili una parte, fino alla metà, dell'importo scontato agli inquilini, proprio per permettere che la crisi non vada a gravare eccessivamente sui proprietari e che, nel contempo, porti un concreto vantaggio agli inquilini in difficoltà e alle famiglie, che potranno vedersi ridotto concretamente l'affitto di casa. Tante cose come questa sono le risposte concrete a chi ci accusa di aver distribuito fondi a pioggia e null'altro. Aggiungo che gli interventi appena elencati sono solo una parte minima del grande e organico lavoro effettuato dal Governo, prima, e dal Parlamento, poi. E tutto sembra tranne una mera distribuzione di risorse senza interventi complementari. C'è da dire anche che, in un momento di crisi che non ha alcun precedente nella storia della Repubblica italiana, appena emanato il primo decreto, la maggioranza ha lavorato nell'immediatezza sui passi successivi da compiere per non lasciare indietro nessuno. Da questo moto nascono i decreti-legge ristori *bis*, *ter* e *quater*, tramite i quali uno dopo l'altro, abbiamo allargato la platea dei beneficiari e introdotto novità importantissime. Mi preme sottolineare un aspetto, caro a me, ma anche a tutto il MoVimento 5 Stelle. Nel decreto ristori-*ter* abbiamo rinnovato quest'anno, con altri 400 milioni di euro, il fondo per consentire ai Comuni di adottare misure urgenti di solidarietà solidarietà alimentare, per dare sostegno a chi è maggiormente in difficoltà. Parlo di difficoltà alimentare, una cosa molto seria. Nessun'altra forza politica è stata così vicina ai fragili e agli ultimi in questo Paese. E se, accanto a questo provvedimento, inseriamo il reddito di cittadinanza, che autorevoli fonti riferiscono essere uno strumento decisivo, importante e fondamentale per una fascia di popolazione che si è ritrovata catapultata senza difesa in questa pandemia, e il reddito di emergenza, che abbiamo fortemente voluto e oggi prorogato, possiamo affermare come il circolo virtuoso di buoni spesa, reddito di cittadinanza e reddito di emergenza abbia permesso alla fascia più fragile della popolazione di questo Paese di non cedere all'incuria, al degrado e alla disperazione. Abbiamo conservato intatta la dignità delle famiglie e dei cittadini italiani. Questo è il MoVimento 5 Stelle e da questi valori siamo nati. Siamo la difesa degli ultimi, degli esclusi, e stiamo attenti alle richieste di aiuto di tutti i cittadini, delle imprese e delle partite IVA, come abbiamo dimostrato durante questi ultimi duri mesi. Mi avvio a concludere, signor Presidente, sottolineando il lavoro e l'impegno che il Governo, questa maggioranza e il MoVimento 5 Stelle hanno posto durante l'*iter* di questi decreti-legge ristori. Il nostro miglior modo di rispondere alle necessità del Paese è fatto di provvedimenti immediati e concreti, non di elenchi di parole vuote, sentiti purtroppo in quest'Aula; provvedimenti concreti, che vanno in aiuto e a sostegno della nostra comunità; provvedimenti legati al progetto di ripresa e alla visione del domani; provvedimenti proprio come questo che stiamo approvando oggi in quest'Aula.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, come stralciato a seguito del vaglio di ammissibilità. «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato 1'emendamento 1.900 del Governo, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, acquisita la relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, all'articolo 15, delle parole «il comma 9 è soppresso», nonché alla soppressione del comma 5-*quater* dell'articolo 19-*ter*. Il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: - il comma 14-*quater* dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente: «14-*quater*. «14-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede quanto a 2.930 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13»; all'articolo 6-*bis*, il comma 7 sia sostituito dal seguente: «7. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, e 6 del presente articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34»; dopo l'articolo 7, siano inseriti i seguenti capoversi: "All'articolo 8, al comma 4, le parole «in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «in «in 274,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni di euro per l'anno 2021»; All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni: "al comma 4, le parole: «121,3» sono sostituite dalle seguenti: «137»; all'articolo 9-*bis*.2 siano apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 sia sostituito dal seguente; «1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.»; b) il comma 3 sia sostituito dal seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo e la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.»; all'articolo 13-*ter*.9, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto- legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi, anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.»; all'articolo 15-*bis*, il comma 11-*ter* sia sostituito dal seguente: «11-*ter*. All'onere derivante dal comma 11-*bis*, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 3,3 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede: 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto; quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 190 del 23 dicembre 2014; *c*) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1 milione di euro per l'anno 2023, 1,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 11-*bis*"; - all'articolo 23-*quater*, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del "Fondo unico giustizia" da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, 7, lettere *a)* e *b)*, del decreto legge 16 settembre 2008, n.143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato."; l'articolo 32-*bis*.l sia sostituito dal seguente: n. 273 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza. 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."; all'articolo 32-*ter*, siano apportate le seguenti modificazioni: a) al comma l-*bis* le parole "e le province autonome" nonché le parole "e dalle province autonome" siano soppresse; la rubrica sia sostituita dalla seguente: *"(Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19)";* *(Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori)*, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.";

Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di personale con contratto di lavoro atipico bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, in essere o scaduti nell'anno 2020, Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai presenti commi con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

32-*bis*, 32-*ter* e 33, e dai commi 1, 2, 3, 5, 9 e 10 del presente articolo, determinati complessivamente in 19.021,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021, 161,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini

per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: "; al medesimo comma-6, la lettera *p)* sia sostituita dalla seguente: quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, di 69,331 milioni di euro per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti

Grazie, Presidente.

hanno garantito il buon clima di lavoro. *(Applausi).* Le risorse messe a disposizione con i quattro provvedimenti, che sono sicuramente importanti per alcuni settori, di certo non basteranno. Siamo in un passaggio delicatissimo in cui ogni nuova restrizione ha inflitto, martoriato dei nostri lavoratori e delle nostre imprese, ferite sempre più profonde. Una terza ondata avrebbe ripercussioni drammatiche e a quel punto non basterebbe di sicuro uno scostamento di bilancio di 20 miliardi e neanche uno di 30. Mi piacerebbe che in quest'Aula si avesse massima consapevolezza su questo punto, e cioè che non possiamo farci guidare dalle emozioni: quelle che un giorno fanno iscrivere tutti al partito degli aperturisti, e il giorno dopo - perché vediamo le foto di quartiere dello *shopping* - passare tutti di colpo a quello dei rigoristi. È un'altalena inutile e pericolosa che dimostra che gli ultimi mesi non ci hanno insegnato molto. Bisogna costruire percorsi guidati in ogni momento dalla razionalità e dal buonsenso, questo vale anche per gli esperti, gli scienziati, che non possono limitarsi a dire che quando crescono i contagi bisogna chiudere, ma sono chiamati a fornire un contributo più fattivo, di costruzione di una prospettiva. Devono aiutare la politica a costruire una strategia di medio e lungo termine, adesso che conosciamo meglio questo virus. *(Applausi).* E bisogna subito iniziare con le vaccinazioni: la Gran Bretagna gli Stati Uniti hanno già incominciato; la Germania inizierà il 23 dicembre. Anche noi dobbiamo dare avvio alle vaccinazioni, perché così salveremo vite ogni giorno. ogni giorno di ritardo fa crescere il numero dei morti. Iniziamo, e subito! Ho detto che ci vuole una strategia, perché la conseguenza di un approccio dettato dal momento è che si producono vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini e categorie economiche. I fatti legati al turismo estivo (le discoteche, le spiagge affollate) hanno fatto scattare un vero e proprio pregiudizio il turismo, la montagna e le attività invernali. Eppure, è evidente a tutti che non sono la stessa cosa e mi sembra

operatori del turismo di montagna e dei settori legati avevano lavorato a protocolli di sicurezza, presentati dalle Regioni interessate alla Conferenza Stato-Regioni. A distanza di un mese, non hanno neppure ricevuto uno straccio di risposta dal comitato tecnico scientifico (CTS). Questo non è un comportamento rispettoso, perché sono istituzioni che sanno cosa serve ai loro territori. Questo perché tutto quello che può ricordare il turismo è diventato un tabù, senza rendersi conto, ad esempio, che con la chiusura degli impianti viene meno la gestione del territorio. E poi davvero lo sci è più pericoloso di una passeggiata in un parco di Roma? Davvero un pranzo in baita è più pericoloso di uno in un ristorante di città? Davvero una funivia e una seggiovia sono più pericolose di una metropolitana o di un autobus? Davvero la fila a un impianto di risalita non è meglio organizzabile di un assembramento in una piazza cittadina? *(Applausi)*. Sta in domande come queste il motivo per cui diventa sempre più difficile introdurre nuove restrizioni e garantirne fino in fondo il rispetto. I cittadini devono capire che le regole vanno rispettate, ma queste devono apparire logiche ed eque, il che vuol dire sempre proporzionate rispetto al potenziale di rischio dei vari contesti. Ne parleremo domani, ma le proteste sugli spostamenti a Natale nascono esattamente per motivi di questo tipo. Per passare al provvedimento, signor Presidente, salutiamo positivamente tutte le norme sulle scadenze fiscali, le rateizzazioni, le proroghe, le sospensioni e le moratorie, così come l'intero pacchetto per il turismo, con gli aiuti per gli stagionali del settore termale e con quelli per commercio al dettaglio, l'artigianato e le imprese edili. Tuttavia, sappiamo che qui bisognerà continuare a intervenire, perché c'è una questione di filiera e di indotto che richiede un'attenzione e un sostegno costante, anche per far passare l'appetito a qualche investitore straniero che ha già messo gli occhi sui pezzi pregiati di questo settore (e ce ne sono tanti, credetemi).

estremamente grande: il commercio al dettaglio, l'agricoltura, l'artigianato, i servizi e l'edilizia.

Grazie a un emendamento del nostro Gruppo, 2 milioni di euro verranno destinati a favorire l'accesso alla didattica a distanza per gli alunni in situazioni di fragilità nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e in Valle D'Aosta. Poi, con la norma sulla A22, il Governo ha dimostrato la volontà di mantenere pubblica l'infrastruttura: non è ancora risolutiva, ma costituisce un buon punto di partenza di quel percorso, per garantire gli investimenti ed esprimere fino in fondo il suo valore strategico; speriamo, tutti assieme, di poterla migliorare. Mi dispiace invece che altre proposte emendative, volte a rendere più efficace la distribuzione degli aiuti, non siano state accolte: penso a quella per sostituire i codici Ateco con il criterio dalla perdita di fatturato su base plurimensile *(Applausi)* e a quello sull'accesso alla cassa integrazione per i lavoratori stagionali dei settori colpiti da provvedimenti sospensivi, come i lavoratori del turismo, delle funivie, del commercio e delle scuole di sci. Questo mi appare oggi come uno dei limiti del provvedimento, perché, com'è stato detto da più parti, rischia di non esserci il principio di congruità sull'importo e sulle platee interessate. Presenteremo nuovamente queste proposte, mentre è giusto sottolineare che, rispetto a precedenti provvedimenti, la velocità di erogazione delle risorse è stata adeguata caso, sappiamo che i tempi non sono una variabile secondaria, ma anzi un elemento di sostanza. Per concludere, signor Presidente, come ha detto la Banca d'Italia, le misure di questi mesi sono riuscite ad attenuare la gravità della situazione, tuttavia le imprese hanno visto aumentare la loro esposizione bancaria e questo grazie anche alle misure che hanno favorito l'accesso al credito. Questo è, in prospettiva, un elemento di rischio e un mancato rimbalzo economico avrebbe pesanti conseguenze anche per le banche. banche. Ancora una volta, quindi, emerge la necessità, per non dire l'urgenza, di concentrarsi sulle politiche per la crescita, a cominciare dal *recovery plan*. Oggi 9 miliardi di euro possono essere liberati dalla sanità per consolidare gli altri ambiti di intervento, se si supereranno, una volta per tutte, le resistenze su MES sanitario sì o MES sanitario no. Per i ritardi e i limiti del nostro sistema sanitario per il progressivo smantellamento della medicina territoriale di base, l'incidenza del virus in termini di mortalità purtroppo non ha paragoni al mondo. Quei 36 miliardi di euro, o almeno una parte di loro, si possono prendere subito e sono fondamentali, se davvero, come dicono alcuni esperti, la terza ondata sarà inevitabile. Oggi siamo ancora in tempo per dare un colpo di reni, a cominciare dalle cose più semplici, come garantire la presenza di personale medico-infermieristico. Anche a tal proposito sono contento che sia passato un nostro emendamento, che prevede la proroga di un anno per il personale a contratto, che non possiede l'attestato di bilinguismo, perché consente la continuità di personale nelle nostre strutture. È vero che molto è stato fatto, ma adesso occorre un altro salto di qualità in avanti, su tutti i fronti. Ci vogliono strategie intelligenti, perché siamo ancora dentro la pandemia e la battaglia contro il Covid non è ancora finita.

del Governo, ci apprestiamo a convertire i decreti ristori, un panetto di provvedimenti che cerca di tamponare il *lockdown* differenziato il Governo ha deciso di applicare a questa seconda ondata del Covid-19. Si tratta di un panetto di decreti che tenta di dare risposte tempestive alle attività che sono state chiuse con i DPCM e con le ordinanze.

sapendo che l'equilibrio tra salute ed economia è sempre molto difficile e che, ancora una volta, ha dovuto avere la priorità la salute. Sappiamo benissimo, però, che coloro che hanno chiuso le attività non possono essere né contenti, né soddisfatti, né sentirsi ristorati dai pochi

molto e con grandissima pazienza sul provvedimento in esame. Nonostante però il clima umano e relazionale molto buono, qua dobbiamo anche dirci una cosa molto vera: questa procedura di conversione

Forse negli ultimi anni, ma ancora di più in quello corrente ci siamo trasformati in un magazzino che riceve i decreti-legge come pacchi e li manda in *Gazzetta Ufficiale* quasi come li ha ricevuti. per quanto il periodo sia difficile, il Parlamento non possa cedere così la propria potestà legislativa, né rinunciare alla propria vocazione, a dare gli indirizzi al Governo e a confermare di volta in volta, come faremo stasera, la fiducia È una questione istituzionale importantissima e nemmeno in una fase grave di Covid come questa possiamo trasformarci in un governatorato; non lo possiamo fare. Dal 2021 questo rapporto sbilanciato tra Governo e Parlamento deve cambiare, come pure l'approccio politico del Parlamento, che vuole scegliere i progetti del *recovery plan* e del Next generation Italia,

è l'indirizzo che il Parlamento vuole dare al Governo rispetto al piano vaccinale. Questo diventa veramente dirimente. Abbiamo sentito ieri le parole chiarissime di Draghi, il quale ha detto la sostenibilità dell'enorme debito che abbiamo fatto quest'anno passa per la crescita e per la realizzazione dei progetti del Next generation. Questo vuol dire che dobbiamo istantaneamente

e ristori; non possiamo più permettercelo, assolutamente. In Gran Bretagna stanno vaccinando 5.000 persone al giorno. L'altro giorno Biden negli Stati Uniti ha annunciato 100 milioni di vaccinazioni in cento giorni. La Germania il 23 dicembre, dopo l'ok della European medicines agency

alcuni suggerimenti che sono stati trasformati in norma e che erano molto attesi, soprattutto dal mondo imprenditoriale. Tra questi voglio ricordare il rinvio dei versamenti delle imposte, cercando di mettere a fuoco una cosa. L'altro giorno ho sentito un intervento piuttosto interessante circa la complessità di approvazione. Sembra un po' un cubo di Rubik: a seconda dei colori, i professionisti devono capire chi paga, quando e come. E qui voglio parlare del ruolo dei professionisti, in particolare dei commercialisti. Abbiamo una classe dirigente altamente titolata, che quest'anno ha visto svilire il proprio ruolo a facchino fiscale. E ha visto questo *downgrade* nonostante non abbia ricevuto alcun ristoro e senza nemmeno il diritto di ammalarsi. Abbiamo proposto un emendamento per tutti i professionisti,

Ci è stato risposto di no, naturalmente dai tecnici ministeriali, che lavorano in *smart working* e sono super garantiti. A me queste risposte preoccupano molto, perché dimostrano l'incapacità di conoscere le difficoltà del Paese e la mancata riconoscenza del reciproco valore e della sinergia che può portare l'Italia fuori

Questa complessità del cubo di Rubik si è ripetuta però anche nel provvedimento in esame. Voglio dirlo come monito *pro futuro*; non vorrei che quest'attitudine alla complessità venisse poi applicata anche alla futura riforma fiscale. Questo nome di riforma alla tedesca, tanto puntuale quanto astrusa, non vorrei prendesse le mosse anch'esso da un nuovo cubo di Rubik, avremmo idee un po' diverse. Nonostante tutte queste difficoltà e questo momento così drammatico, rispetto al quale bisogna fare un passo avanti, abbiamo investito in questo decreto 18 miliardi, cinque dei quali serviranno

prima di ripartire, per rafforzare le misure esistenti, colmare gli Ateco delle attività che sono state escluse e introdurre formule perequative. Ci sono attività stagionali che nel fondo perduto aprile su aprile ovviamente non possono essere soddisfatte. Ci sono moltissime attività in filiera che hanno perso

Al di là del fatto tecnico, sono molto preoccupata, perché, quando in norma si introduce un riscatto forzoso, come Stato e come modello Paese stiamo dando un messaggio a tutti gli investitori: stiamo dicendo che in Italia, qualora serva, facciamo norme per riscattare le azioni degli investitori. Questo è un messaggio che non può essere veicolato molto a lungo e al di fuori di quest'Aula. Le difficoltà e le contraddizioni - è inutile negarlo - ci sono, ma Italia Viva ha scelto di continuare a lavorare per chi lavora, per chi ha voglia di lavorare per rimettere l'Italia in pista, per chi soffre e per chi ha voglia di correre.

Crediamo che in questo momento sia importante invece proteggere gli italiani dalla pandemia con moltissimo coraggio e moltissima lungimiranza.

ma anche all'intero arco del Parlamento, ai colleghi della Lega, di Forza Italia, del MoVimento 5 Stelle, del Partito Democratico, alla maggioranza. Mi rivolgo a voi perché avete sentito, come me e come gli italiani che hanno avuto la pazienza di ascoltarci anche sui canali satellitari, canali satellitari, che oggi probabilmente, dimenticando gli ultimi venti secondi dell'intervento della collega Conzatti e del collega Steger,

Non c'è parola e non c'è considerazione che abbiano fatto il collega Steger e la collega Conzatti che non trovino il centrodestra unito pienamente d'accordo. Avete di fatto demolito la politica sanitaria del Governo. L'ha demolita il collega Steger. Avete demolito il rapporto con il mondo delle professioni. Eppure, i due colleghi che mi hanno preceduto sono parte della vostra maggioranza. Credo che abbiate da riflettere su quello che oggi rappresentate nel Paese, cioè molto poco, molto vicino allo zero. E non basta, perché, prima di entrare nel merito del provvedimento al nostro esame, ribadisco che gran parte dei contenuti del mio intervento l'hanno svolta i colleghi di maggioranza che mi hanno preceduto.

Vorrei vedere qualche Ministro presente qui, durante una dichiarazione di fiducia, visto che noi parlamentari abbiamo lavorato per giorni e anche nottate nelle Commissioni per arrivare a questo momento. Purtroppo, vedo solo

che il 1° gennaio, cioè tra poco più di quindici giorni, entreranno in vigore le norme sul credito, il *calendar provisioning*. Tali norme possono minare in modo drammatico il nostro sistema economico.

né un estremista della Lega o di Fratelli d'Italia, come talvolta li definite, che ha detto nei giorni scorsi che siamo di fronte a una bomba atomica per il credito italiano. Quel signore, tanto per chiarirci, è l'amministratore di Mediobanca. però, in Commissione d'inchiesta sul sistema bancario, il direttore dell'ABI Sabatini ha usato parole molto, molto dure e sferzanti nei confronti della situazione attuale, parlando di desertificazione del sistema produttivo italiano per effetto delle norme di quell'Europa che non perdete mai l'occasione di esaltare, anche quando distrugge - e l'ha distrutto - il sistema finanziario del credito italiano. Il 1° gennaio, amici del Partito Democratico, entrano in vigore quelle norme europee per le quali - ricordiamolo agli italiani - basteranno novanta giorni di ritardo nel pagamento di soli 100 euro per gli individui e 500 per le imprese per diventare

È una vergogna e voi sarete chiamati a rispondere di questo davanti alle piccole e medie imprese italiane, un terzo

sede. Ho voluto utilizzare questo tempo per rivolgere un appello accorato, di cuore, che viene da quelle imprese che stanno soffrendo e alle quali non state dando risposta. Per quanto riguarda il decreto-legge, dopo aver condiviso contenuti e parole di coloro che mi hanno preceduto, non voglio esacerbare né evidenziare ulteriormente il mostro giuridico che avete creato con quattro decreti mescolati l'uno all'altro, ma voglio esporvi una considerazione, anche *pro futuro.* Cari colleghi, quel poco di buono che c'è in questo decreto è frutto del lavoro che abbiamo fatto tutti insieme, maggioranza e opposizione, nelle Commissioni parlamentari. Quei miseri 600 milioni su quasi 20 miliardi, cioè quel misero 3 per che è stato dato in dotazione alle Aule parlamentari, hanno prodotto le uniche note positive che sono state giudicate così non da me, ma dalla stampa. Leggete gli articoli de «Il Sole 24 Ore», di «Italia oggi» della principale stampa specializzata e vedrete che i tre quarti dei loro commenti non riguardano i 20 miliardi che avete utilizzato, ma per lo più gli emendamenti di maggioranza e di opposizione che il Parlamento nelle Commissioni ha saputo approvare. Questo dovrebbe far riflettere ulteriormente una maggioranza - o, meglio, un Governo che si sta dimostrando sempre più lontano dagli italiani e che, come magistralmente ha detto il mio collega senatore Urso poche ore fa, è forse molto più interessato a vicende personali e a lotte sul potere nelle banche che non agli interessi degli italiani, delle nostre imprese e dei nostri artigiani. artigiani. Vogliamo parlare dei professionisti? Vogliamo ricordare, come ha detto la mia collega senatrice Conzatti, quella categoria

contributo a fondo perduto? Ricordiamo che i professionisti sono stati esclusi anche dai ristori, oltre che dai contributi del decreto estivo, senza motivo; anzi, il lavoro encomiabile dei miei colleghi commercialisti, ma di tutti i professionisti italiani, avrebbe dovuto essere premiato in un momento così difficile, invece non li avete neppure considerati alla pari degli altri lavoratori. questi professionisti, però, non avete voluto neanche riconoscere ciò che non costa, perché sono di queste ore non le mie lamentele quale primo firmatario, insieme alla consulta dei parlamentari commercialisti, del disegno di legge sulla malattia e l'infortunio dei professionisti, ma le agenzie di tutte le categorie professionali, lo sottolineo. Voglio citarne una

i quali hanno detto chiaramente che è una vergogna che non si proceda in tempi celeri, dopo che la Presidenza ha dato la possibilità al Senato di lavorare su questa materia. Vi state arrampicando davvero sugli specchi non dare nulla ai professionisti, anzi, per togliere loro anche quel diritto alla salute e all'infortunio al quale avrebbero pieno titolo. Visto che il tempo mi pare che stia terminando, vi chiedo ancora un minuto per poter concludere su due passaggi. Condivido in pieno la posizione sull'autostrada del Brennero, una delle migliori concessioni autostradali europee, che state cercando di espropriare, con un concetto giuridico degno di un passato comunista che non dovrebbe avere niente a che vedere con la cultura liberale. State espropriando espropriando una proprietà privata, senza che ciò abbia la benché minima funzione di utilità sociale, che sarebbe l'unico elemento che lo potrebbe giustificare. Voglio concludere quindi

all'inverno, non c'è nulla per la ripresa, tutto è fondato sulla logica dell'assistenzialismo, del reddito di cittadinanza e di emergenza, sempre sulle passività.

legati all'emergenza. Lo ricordo perché è difficile discutere se, quando facciamo interventi sui ristori, si chiede di discutere della strategia. Se andassi a leggere gli innumerevoli emendamenti

infatti migliaia di emendamenti dell'opposizione che vanno esattamente nella direzione dei ristori. Tuttavia cari colleghi dell'opposizione, abbiamo fatto meritoriamente uno sforzo insieme. Ciò

e voglio interpretarlo come il primo passo di un ragionamento che va fatto poi anche sui prossimi provvedimenti. Quando parlate di briciole, vorrei ricordare che nel provvedimento al nostro sono misure che giustamente avete richiesto a gran voce, come per esempio il rinvio di tutte le scadenze fiscali, che vale diversi miliardi. Attenzione, non vorrei che metteste in discussione anche le battaglie che avete fatto in questi mesi e che hanno trovato una risposta positiva da parte del Governo.

questioni rilevanti, che riguardano il sistema delle imprese e i problemi sociali, e lo avete condiviso anche voi, per una serie di proposte che ha fatto la maggioranza.

baseremo finalmente sul fatturato e sulla conseguente riduzione delle tasse. Questa è una scelta politica che il Governo ha già fatto e presentato, su cui mi aspetto, ristori, un grande apprezzamento dell'opposizione, perché questa è la strategia che ci avete più volte evocato.

Vorrei dire una cosa, prima di tutto a noi della maggioranza: siamo tutti consapevoli che il *recovery fund* è un'occasione storica, storica, forse unica; per corrispondere bisogna avere il coraggio di cambiare il Paese. A me francamente della discussione su cabina di regia, *staff* dirigenziale e tecnici interessa fino a un certo

perché non la pensiamo tutti allo stesso modo, altrimenti non saremmo a sedere in posizioni diverse. Ben venga questa discussione. Sapete qual è la mia paura? Ve lo dico con sincerità

Certo, è banale dire che 9 miliardi per la sanità sono una scelta assolutamente inadeguata. Ma io voglio capire cosa facciamo sulla sanità, quale strategia assumiamo, quale rinnovamento del sistema del rapporto tra sanità territoriale e ospedaliera. Voglio capire e non mi accontento più, a seconda dei momenti, di dire che le Regioni devono contare di più e di meno. Quale idea abbiamo di Paese? Chi fa che cosa? Quale responsabilità ci assumiamo? Queste sono le vere discussioni. Colleghi, davvero volete il rimpasto o il rimpastino? Ma dove pensiamo di poter andare? *(Commenti).* State calmi. Fuori di qua i cittadini italiani ci chiedono di svolgere la nostra funzione. La nostra funzione, ci piaccia o non ci piaccia, è avere il coraggio, la forza e la determinazione di cambiare questo Paese, in modo tale che fra qualche anno la discussione classica, per esempio, sul prelievo fiscale non si faccia più, perché avremo costruito più giustizia, più equità, più libertà.

parole e chiacchiere. Il Paese, se vogliamo riprendere e ricostruire, ha bisogno di una svolta, prima di tutto culturale. E questa svolta noi, colleghi della maggioranza, ci piaccia o meno, siamo obbligati a farla, perché non c'è alternativa in questo Parlamento che non sia il fatto di riuscire a realizzare questa svolta.

nei decreti-legge e che questa Camera ha contribuito a rafforzare. Molti di voi hanno parlato delle misure nel merito mi permetto di ricordarne solo una, una piccola misura che riguarda l'esonero dal versamento TOSAP e COSAP fino a marzo 2021; una piccola misura che dà un segnale in questa fase difficile ai bar e ai ristoranti, che danno maggiore vivacità e vitalità alle nostre città, oggi rabbuiate dalla pandemia. Nel mio intervento vorrei esprimere due apprezzamenti e un auspicio: il primo apprezzamento riguarda il lavoro svolto dalla maggioranza e dalle opposizioni. Lo dico senza ipocrisia: alcuni toni esacerbati di questa sera non attenuano il valore del lavoro fatto insieme ed è un bene averlo fatto perché aver lavorato insieme ha migliorato l'impianto originario. Spero che questo metodo possa continuare anche nel futuro perché questo ci chiede il Paese, di lavorare insieme prescindendo dai ruoli che oggi abbiamo e che penso avremo anche nel futuro. Il secondo apprezzamento riguarda il rapporto con il Governo. Sono presenti due Sottosegretari che ci hanno seguito passo per passo e anche il Ministro per i rapporti con il Parlamento. È stata una collaborazione utile, costruttiva, preziosa e leale, ma voglio aggiungere una cosa: questa procedura legislativa andrebbe ripensata andrebbe ripensata perché, se analizziamo bene, tra pareri, bollinature, pareri successivi e altro e altro l'ampiezza dell'esercizio del nostro ruolo di legislatori eletti democraticamente dai cittadini è molto ridotto.

L'auspicio è di passare dalla filosofia dei ristori alla filosofia del sostegno alle filiere produttive, alle famiglie, ai professionisti, ai settori economici più vessati dalla pandemia perché non è vero che tutti

nell'incendio e dobbiamo spegnerlo anche con misure assistenziali, anche con i ristori, con ciò che allevia, ma non crea condizioni di ripresa e di resilienza. Adesso deve arrivare il momento della transizione, dall'emergenza (la casa che brucia) al Paese che va ricostruito e anche un po' ripensato.

Next generation EU o *recovery plan*, è perché c'è un'Unione europea che mette a disposizione 209 miliardi tra sovvenzioni e prestiti per l'Italia. Questa grande opportunità non va sprecata, non va sciupata ma va utilizzata per dare fiato e respiro alle grandi potenzialità di questo Paese. Questa è una fase di transizione cui dobbiamo andare sapendo che c'è una realtà forse ancora più grave di quella che avvertiamo. Non sottovaluto l'allarme che ieri il gruppo di lavoro del G30 ha lanciato sulla dimensione della sofferenza che c'è nel mondo, lenita dalle

ma è dall'analisi dura della realtà che può e deve partire la rinascita. «È di notte che è bello credere nella luce» scriveva Edmond Rostand e noi ci crediamo e lavoriamo perché torni a splendere il sole sul nostro amato Paese. forse non tutti i colleghi della maggioranza ricordano che l'*incipit* dell'articolo 41 della Costituzione italiana che abbiamo sotto il banco e dovremmo tutti aver presente - recita che l'attività economica è libera. Quindi, l'approvazione di un provvedimento di ristoro non si configura, come ho sentito da parte di qualche collega della maggioranza, come una gentile concessione alla libera impresa. Una norma di ristoro è un atto dovuto e necessario nel momento in cui lo Stato - attraverso il Governo, prima, e il Parlamento, decide di limitare e di chiudere la libera iniziativa economica sancita dalla Costituzione italiana, seppure in modo temporaneo e modulato. Non è la prima volta, in epoca moderna, che l'Occidente si trova ad affrontare eventi come quello che stiamo vivendo. Ci sono stati grandi eventi pandemici: penso alle pestilenze del 1340 e del 1630, alla Prima guerra mondiale (dal 1914 al 1918), all'epidemia di influenza spagnola nel 1919, alla grande influenza asiatica del 1957. Eppure, è la prima volta che l'Occidente ha scelto e ha deciso di limitare le libertà personali, la mobilità delle persone, la dimensione della socialità - tanto preziosa, per esempio, per i nostri ragazzi e per i nostri anziani - e di limitare soprattutto le libertà economiche, che sono l'elemento di certezza e di sicurezza attraverso cui ciascuno costruisce la propria esistenza. Questa decisione è stata assunta perché oggi viviamo sicuramente in un mondo interdipendente, dove le libertà non sono solo scontate, ma rappresentano il fondamento della vita civile e democratica, e i Governi europei, in modo particolare - ha ragione, collega - hanno scelto di privilegiare la strada di anteporre la vita e la salute all'economia e alla socialità. a ciascun Governo - anche a quello italiano - tocca singolarmente il compito di pensare non soltanto al rischio sanitario, ma anche alle prospettive economiche che ne derivano, perché la salvaguardia del tessuto economico, delle imprese e del lavoro delle persone sono obiettivi e valori per noi irrinunciabili.

perché nel dizionario della lingua italiana «emergenza» significa un evento improvviso, inaspettato e circoscritto nel tempo. Ora, sfido ciascuno in quest'Aula a definire il Covid, dopo un anno in cui non abbiamo elementi scientifici *(Applausi)* né elementi sanitari, conosciamo il tempo di durata né abbiamo certezza dei vaccini, ripeto, sfido chiunque a definire il Covid un'emergenza. Il Covid è un evento con cui ci dobbiamo confrontare, che ci pone di fronte alla necessità di dare risposte a un'emergenza sanitaria, a un tema economico ed è un evento nefasto destinato, purtroppo, a durare nel tempo. Un evento che non si può affrontare con decreti a singhiozzo, come avete fatto voi ma che richiede, come giustamente ha detto Errani - ma mi stupisco che lo dica lui, che non dovrebbe fare domande ma dare risposte, visto che è maggioranza un impegno che dovrebbe implicare da parte della maggioranza la capacità di mettere in piedi una prospettiva, un piano, una capacità di avere una visione

Provo a tradurlo in termini ancora più semplici. Secondo voi, davvero una cifra che va dal 40 al 60 per cento del fatturato di aprile 2019, alla traslazione delle imposte, che poi dovranno essere pagate nel 2021 (insieme alle imposte del 2020 traslate al 2021, ma anche quelle del 2021),

Se oggi molte attività sono ancora aperte, non è grazie alla gentile concessione dei vostri ristori, ma è grazie alla capacità e alla volontà dei risparmiatori di mettere mano alla propria tasca e di mettere i propri soldi nell'impresa, per salvare l'impresa stessa e per salvare il lavoro. Ma questa cosa, chiaramente, non può durare per sempre, perché, come si dice dalle mie parti, anche gli *schei* a un certo punto finiscono e bisogna avere delle idee, bisogna avere un progetto, bisogna avere la capacità, soprattutto da parte vostra, che avete la responsabilità di spiegare quali politiche di sviluppo avete in mente per questo Paese. Anche se, come centrodestra, siamo riusciti ad ottenere qualche risultato, anche grazie alla disponibilità che vi abbiamo dato sullo scostamento del bilancio, denunciamo questa mancanza di visione della maggioranza,

i teatrini che state facendo sul rimpasto e le discussioni sulla cabina di regia. Le nostre imprese vogliono sapere quali saranno le misure strategiche che consentiranno di contare su un tessuto sociale economico in grado di garantire una possibilità di ripresa.

ma anche in termini fiscali, perché se non c'è chi produce la fiscalità lo Stato non si regge in piedi. *(Applausi)*. Se non c'è chi paga le tasse nel Paese, come mandiamo avanti la macchina pubblica? Come paghiamo gli stipendi dei medici? Come paghiamo gli stipendi degli operatori della pubblica sicurezza? Come paghiamo le pubbliche amministrazioni, i Comuni e anche le pensioni (perché ci può essere una ricaduta anche in termini pensionistici)? Se voi siete rassegnati, cari colleghi della maggioranza, al fatto che sia normale rinunciare alle libertà personali, alla socialità e che sia normale limitare la libertà di impresa, noi non siamo rassegnati a questo. Pensiamo che non sia normale e che, quando lo si fa, bisogna assumersi la responsabilità di mettere in campo immediatamente delle risposte, per poter dare un futuro al Paese e, soprattutto, ai nostri giovani. Penso che l'unica soluzione sia mettere in campo un grande progetto di investimento e di rilancio dell'economia. Una visione di futuro di questo Paese che voi, in tutta evidenza, avete dimostrato, in queste settimane e in questi mesi, di non avere; una visione che vi manca e che non apparirà d'incanto a seguito di *summit*, riunioni o tentativi di rimpasto. Per queste ragioni, annuncio il voto contrario alla fiducia da parte del Gruppo Forza Italia.

Dopo il secondo *lockdown* avete emanato il primo decreto ristori, dopo dieci giorni è arrivato il secondo, poi vi siete accorti che le Regioni cambiavano colore e avete dovuto emanare il terzo, poi avete capito che molte attività non sarebbero state in grado di pagare le tasse e avete fatto il quarto, adesso vi siete accorti che le risorse non sono sufficienti e ne avete previsto un quinto, a testimonianza del fatto che non si può pensare di andare avanti a tentoni, come fa il Governo, per risolvere davvero i problemi delle tante attività e dei tanti cittadini che hanno sofferto per questa pandemia.

di usare il termine e di prevedere indennizzi e non ristori, perché il termine giuridico indennizzi significa che il beneficiario ottiene né più né meno di quello che ha perso, mentre col termine ristori, artifizio di questo Governo, la persona che ha subito il danno si deve accontentare di quello che lo Stato fondamentalmente le può dare e quindi delle elemosine *(Applausi)*, perché stiamo parlando di questo. una collega ha citato le 73.000 imprese chiuse, di cui 17.000 probabilmente non riapriranno più: stiamo quindi parlando di danni drammatici. terzo luogo, abbiamo detto che le risorse non sono sufficienti e che molte categorie sono rimaste escluse, non si è riusciti ad andare oltre la questione dei codici Ateco, non si è guardato alla logica del fatturato e addirittura state escluse tantissime filiere, *in primis* quella dell'agricoltura, di cui vi siete assolutamente dimenticati, e poi quella del turismo, un altro settore che avrebbe bisogno di maggiore sostegno, visto quanto è

È sbagliato prendere a riferimento solo un mese, perché i danni della pandemia hanno causato problemi in tutti i mesi dell'anno e non solo nel mese di aprile. Lo stesso sindaco di Milano,

Penso ai tanti ambulanti che potevano organizzare fiere nei Comuni; ma i Comuni non si prendevano la responsabilità di fargli organizzare le fiere, nonostante lo si potesse fare. Alla fine questa gente, anche se poteva lavorare, non ha lavorato; e nei loro confronti cosa avete previsto? Zero, questo è il punto.

dopo le 23 dello stesso giorno in cui scadevano i termini per presentare gli adempimenti alla dichiarazione dei redditi. Il cittadino avrebbe dovuto immaginarlo prima

Qualcuno dice che l'avete fatto apposta, così molti non hanno avuto probabilmente il tempo di organizzarsi in questa direzione. Inoltre (settimo motivo) il decreto ristori-*quater* rinvia al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate sulla rottamazione-*ter* in scadenza nel 2020. Chi beneficia di questa sospensione dovrà pagare tutto il 1° marzo e dovrà pagare anche la prima rata del 2021. Ma davvero potete pensare che chi era in difficoltà prima della pandemia dopo la pandemia possa pagare tutto in un'unica rata, con l'anno nuovo,

tra gli emendamenti che avete approvato in maggioranza, la cosa più scandalosa è che, di fronte a un tema così importante come quello dei ristori, abbiamo visto degli emendamenti, che per fortuna il Presidente del Senato ha dichiarato inammissibili,

Parliamo di interventi che si fanno normalmente in una legge di bilancio, non in un provvedimento che deve aiutare le aziende che sono in grave difficoltà. Come si fa a presentare emendamenti che vanno in questa direzione?

sulle bollette elettriche, portato avanti dal collega Arrigoni, sicuramente è un passo in avanti, come i maggiori trasferimenti alle Regioni e le maggiori risorse per il trasporto pubblico locale e per fare le convenzioni con i taxi, gli NCC e quant'altro. parliamoci chiaro: è veramente un primo passo. Di questo vi va dato atto; però, da qua a pensare che questi tre emendamenti potessero farci cambiare idea, davvero ce ne vuole tanto. Alla faccia della collaborazione! *(Applausi)*. Il decimo e

doverne intrecciare quattro. Chissà che cosa viene fuori: scadenze, adempimenti, posso fare quello, posso fare quell'altro. Si tratta davvero di una confusione normativa che non aiuta i beneficiari, che rischiano di non prendere poi

propagandato? Utilissimo nelle sue finalità iniziali, però purtroppo tutti ne parlano, ma nessuno sa come farlo. Tanto è vero che il ministro Patuanelli a un'interrogazione ha risposto che gli interventi da maggio ad oggi

Queste norme scritte male vanno in questa direzione. La morale qual è? È che purtroppo - lo dico portando stima nei confronti di molti colleghi che sono in maggioranza -, nel momento più difficile per l'Italia dal dopoguerra ad oggi, purtroppo ci troviamo di fronte al Governo più imbarazzante della storia d'Italia. Presidente, è per me un onore intervenire oggi, in un momento così difficile e delicato per il Paese, quando portiamo a compimento un'opera: siamo riusciti ad approvare quattro decreti-legge in uno con questo clima, quindi direi che siamo riusciti veramente a fare qualcosa di grande. *(Applausi)*. Sono veramente orgoglioso di questo e ringrazio tutta la maggioranza, tutta l'opposizione

Causin; è un'emergenza evolutasi nel tempo toccando in modo diverso Regioni diverse. Quindi abbiamo dovuto intervenire in modo diverso: mi sembra molto, molto semplice. Ora siamo riusciti a mettere a sistema queste norme e le approviamo tutte insieme: una cosa veramente fatta bene. Molti ci accusano del fatto che le norme sono frammentarie. Ma siamo consapevoli a quante categorie di cittadini e di imprese dobbiamo rendere conto e dare dei ristori e degli aiuti? Ebbene, per questo motivo le norme sono frammentarie: sono veramente tante le categorie alle quali dobbiamo riferirci. Insomma, abbiamo speso 100 miliardi quest'anno e probabilmente ne serviranno molti anche l'anno prossimo, perché i numeri li vediamo tutti. I numeri sono gravi e la situazione è ancora grave: se a marzo avevamo come picco 6.000 casi al giorno, adesso continuiamo ad averne 12.000, e non sono pochi. Dobbiamo renderci conto di questo: la situazione è ancora difficile. Ma guardiamo avanti. Siamo riusciti ad avere sicuramente un buon passo. Siamo riusciti a collaborare con l'opposizione, e non è stato facile. Però devo dire che anche l'opposizione è riuscita a a portare a casa - direi a portare nelle case degli italiani - tre cose molto importanti. Direi quindi grazie per le cose che ci avete suggerito *(Applausi)*. Probabilmente le avremmo fatte anche noi, ma ho visto che voi voi sponsorizzate poco le cose che avete fatto, come se vi vergognaste che la maggioranza ha dato l'opportunità anche a voi di fare qualcosa di concreto per i cittadini italiani. Signor Presidente, noi siamo davvero orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, però abbiamo visto che dall'altra parte si è lavorato, sì, ma c'è sempre stato qualcuno che voleva fare lo sgambetto, qualcuno che voleva lo sgomitamento *(Applausi)*, qualcuno che sempre in modo strumentale ha messo un po' il bastone tra le ruote. Ma va bene così, va bene lo stesso, perché noi abbiamo un obiettivo: quello di far del bene ai cittadini che più hanno bisogno. Quindi, se vuoi continuerete con le ingiurie, noi andremo avanti lo stesso. Se voi andrete avanti con gli schiaffoni al posto degli abbracci, a noi va bene lo stesso, perché abbiamo solo quell'obiettivo e continueremo a porgere l'altra guancia, perché vogliamo fare del bene ai cittadini che hanno bisogno. E continueremo a fare del bene. Presidente, il momento è difficile. Ci stiamo avvicinando al Natale, un momento in cui tutti vogliamo stare vicini alle nostre famiglie, alle famiglie che stanno lontano, ai familiari che stanno lontano. la distanza e la solitudine; molte famiglie hanno sopportato il dolore, quindi è un momento in cui vogliamo stare più vicini. Purtroppo però le condizioni non ci lasciano la possibilità di farlo. So che ora sono in discussione le misure per il Natale, e mi vieni da fare questa preghiera: innanzitutto a tutti noi e a tutti i cittadini italiani, di fare il possibile per rispettare queste regole. Ma soprattutto, se vi fosse l'idea di mettere in discussione queste idee, chiedo di farlo con grandissima attenzione,

e sono italiani i ricercatori che vincono più concorsi per realizzare progetti interessanti. Purtroppo in Italia non abbiamo gli strumenti. Dobbiamo fare il possibile per trattenerli e quindi abbiamo rinnovato quantomeno per tre mesi le borse di studio alle dottorande e ai dottorandi. È un minimo, però quantomeno gettiamo le basi per una riforma che deve

seguire l'insegnamento da casa. Andiamo avanti e pensiamo ai problemi di tutti i giorni. Pensiamo a quelle famiglie che devono pagare un affitto troppo alto. Sappiamo benissimo che purtroppo il reddito per molte persone è sceso. Per il problema della casa ci siamo inventati un premio per i proprietari di immobili che decideranno di abbassare l'affitto ai loro inquilini. È una misura unica, sperimentale, che abbiamo provato, l'abbiamo scritta e siamo riusciti a realizzarla. *(Applausi)*. I proprietari potranno ricevere fino al 50 per cento dello sconto del canone che faranno ai propri inquilini. Proviamoci, magari non sarà la soluzione ottimale, ma vediamo come va e al massimo ci metteremo anche altre risorse oltre ai 50 milioni già stanziati. stanziati. Colleghi, vi devo ringraziare col cuore perché per sei mesi abbiamo lavorato tutti insieme ad una misura che adesso ha preso concretezza, cioè il sovraindebitamento. L'ho ripetuto diverse volte in quest'Aula. Purtroppo non ci siamo mai riusciti ma adesso ce l'abbiamo fatta. Abbiamo migliorato le norme sul sovraindebitamento per dare una mano alle persone che più hanno bisogno e che non riescono a pagare i loro debiti.

Migliorando le norme sul sovraindebitamento, le famiglie potranno accedere tutte insieme alla procedura, spendendo meno. Potrà essere più facile accedere alle procedure anche per i piccoli imprenditori. Ma soprattutto abbiamo reso possibile la famosa esdebitazione grazie alla quale chi non ha nulla non darà nulla, ed è la cosa più importante perché è un concetto che dovremmo imparare anche a livello internazionale, visto che purtroppo molti Paesi sono veramente molto in difficoltà. *(Applausi)*. Non aggiungo altro, se non che è necessaria molta creatività. Nelle cose che facciamo, colleghi, dobbiamo metterci creatività, altrimenti le leggi rimangono grigie e scure, mentre dovremmo fare qualcosa in più per renderle effettivamente utili ai nostri cittadini. Quindi mettiamoci creatività. Tra l'altro siamo in un periodo ricco di nuove risorse e di nuove opportunità. Servono nuove idee. Secondo me siamo sulla strada giusta. Continuiamo su questa strada, con forza e decisione ma anche ascolto e condivisione. *(Applausi)*.

Il presidente Romeo le sta chiedendo la parola sull'ordine dei lavori che precede l'intervento del senatore Paragone. PRESIDENTE. No, non può precedere, perché devono finire le dichiarazioni di voto. l'intervento sull'ordine dei lavori va fatto immediatamente. Lei lo può rifiutare, ma lo deve accogliere.

*(Applausi)*. Più che decreto ristori lo avreste dovuto chiamare decreto "spera in Dio" perché ormai la vicenda dei ristori sta diventando una lotteria:

fare il predicozzo ai cittadini quando noi siamo i primi a stare lì riuniti in capannello. Più che decreto ristori lo avreste dovuto chiamare decreto "spera in Dio" perché ormai la vicenda dei ristori sta diventando una lotteria: se la fortuna ti assiste, allora pigli qualcosa. Quando eravamo piccoli al bar dell'oratorio prendevamo i boeri, e non il Boeri dei vaccini petalosi, no: prendevamo i boeri del bar nella speranza di vincere altri boeri o altri premi. Anche con voi si scarta il decreto e si spera nella fortuna: chissà se piglio qualcosa? Chi intanto piglia è il suocero di Giuseppe Conte con la norma salva furbetti tassa di soggiorno *(Applausi)*, nota anche come norma salva suocero, della quale il suocero del *Premier* si è subito avvalso con effetto retroattivo. Per uno che piglia, tanti invece non pigliano, perché non hanno un conto in famiglia, perché sono figli di nessuno o perché impigliati nella riffa dei codici Ateco. Mi scrive la signora Rosy, una ristoratrice: «Mi ritrovo senza ristori, con una stagione turistica inesistente, con costi fissi mai sospesi. Qui si continua a prendersi gioco di tutti noi giocando con i codici Ateco, non tenendo conto che dietro al numerino di appartenenza ci sono famiglie e dipendenti esasperati». Stamattina i ristoratori sono scesi a Roma, hanno protestato davanti a Montecitorio. «Fermi noi fermi tutti» era scritto sul volantino che hanno distribuito, un volantino pieno di proposte per rilanciare il settore dell'ospitalità, uno dei settori che voi state distruggendo lentamente. I settori delle agenzie di viaggio, dell'agricoltura, del *wedding*, delle palestre sono letteralmente piegati. Signori del Governo, avete capito o no che gli operatori economici hanno il fiato sul collo delle banche e che una segnalazione alla centrale rischi significa morire definitivamente? Lo avete capito che i fornitori devono essere pagati, che la merce è in deposito? A chi già paga gli abbonamenti del *software* di gestione per le fatture elettroniche avete caricato altri costi gestionali per la vigliaccata del *cashback* o per la trappola della lotteria degli scontrini. Avete diviso l'Italia in zone rossa, arancione e gialla; poi, quando scatta il colore giallo, ve la prendete con i cittadini e con i commercianti perché non si sono imposti l'auto *lockdown* e dopo avere spinto per il super *cashback*. Il Governo, che quindi non ha predisposto il piano pandemico, esponendo cittadini e operatori sanitari anche al pericolo di morte, si permette di fare la morale. Voto no a questo Governo amico dei suoceri, delle banche e delle multinazionali, cui è permesso tutto, anche pagare un po' di tasse. Italexit vuole superare il falso mito del *deficit.* Chi ha moneta sovrana non fallisce e soprattutto non permette che fuori dai centri d'aiuto ci siano centinaia e centinaia di persone in fila per un pasto caldo.

Sappiamo che di solito, passando alla votazione del maxiemendamento, quando c'è la chiama ci sono alcuni impegni istituzionali, per cui alcuni senatori possono accedere e votare per primi rispetto ad altri. però l'orario e dubitando, essendoci il coprifuoco, anche del fatto che ci siano a mezzanotte alcuni impegni istituzionali, mi auguro che nella seduta di questa sera si segua normalmente il corso dell'estrazione.

Come deciso dal Consiglio di Presidenza, noi dovremmo rispondere ciascuno dal proprio posto. Abbiamo altresì stabilito un certo numero di presenze all'interno dell'Aula e negli spalti soprastanti. Se uno prende visione dell'Aula in questo momento, si rende conto immediatamente che c'è il doppio delle presenze rispetto alle previsioni fatte dai nostri questori, non ultime le presenze in piedi tra i banchi e nell'emiciclo. Le chiedo quindi che i numeri vengano fatti rispettare perché, nel momento in cui ciascuno di noi sarà chiamato ad esprimere il proprio voto, non sarà a una distanza di sicurezza rispetto a quelle che sono le previsioni. È inutile poi fare il ricambio d'aria, se poi ci sputiamo addosso. Quindi, tutti coloro che sono in più devono uscire dall'Aula e votare da altri spazi. il richiamo del senatore Calderoli mi pare appropriato. Vedo un assembramento nell'emiciclo. Prego ciascuno

nel senso di occupare i posti per quella che sarà la chiamata anche nelle tribune. Siccome stiamo tribune. Siccome stiamo parlando continuamente di emergenza, di misure di sicurezza, di mascherine e di restrizioni, ciascuno di noi si restringa. Non

io aspetto, tanto stiamo qua e passiamo la serata assieme.

come stralciato a seguito del vaglio di ammissibilità e corretto secondo le indicazioni della Commissione bilancio, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.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

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. senatore Caliendo).*

Coltorti,

interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sull'approvazione del quale

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 137.